Di Taranto e di Ilva si parla praticamente da sempre in Parlamento, a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso. Taranto è stato un simbolo positivo e vanto dell'industrializzazione del Mezzogiorno d'Italia, ma è nel 2012 che comincia quella che potremmo definire la sua travagliata storia moderna. In quell'anno la procura di Taranto ordinò il sequestro degli altiforni, giudicati altamente inquinanti. Nonostante quei sequestri, però, fino ad oggi, di fatto, quegli altiforni non hanno mai smesso di funzionare. Con l'affidamento dell'acciaieria al commissariamento, però, la loro capacità produttiva si è progressivamente ridotta. Nel 2018 l'intero impianto è stato acquistato, con bando pubblico, dal colosso mondiale d'acciaio ArcelorMittal, che aveva il compito di rimettere in piedi l'azienda tentando di risanarla. Ma anche questo tentativo è fallito, anche perché - bisogna ricordarlo - il Governo Conte ha stracciato gli accordi contrattuali precedentemente sottoscritti. Lo Stato italiano ha deciso quindi di diventare direttamente proprietario della società. Per mezzo di Invitalia oggi lo Stato possiede il 32 per cento del capitale, in attesa che la quota superi la maggioranza a maggio del 2024, così come previsto dagli accordi. Con questo decreto-legge la stessa Invitalia viene autorizzata a effettuare ulteriori rafforzamenti patrimoniali sino a un importo di un miliardo. Un ulteriore finanziamento in conto soci, nel limite massimo di 705 milioni di euro, servirà a risollevare l'azienda, a oggi a corto di liquidità principalmente per via dell'aumento dei prezzi del gas, e dovrà essere impiegato *in primis* per pagare i debiti contratti con le società energetiche ENI e Snam. Qualcuno ieri nel dibattito ha parlato semplicisticamente di pagamento delle bollette. Fin qui potremmo dire che va tutto bene. Si tratta di garantire la sopravvivenza del colosso industriale della siderurgia italiana e dell'occupazione, coniugandola al meglio possibile con la tutela ambientale e della salute dei cittadini di Taranto. La questione più spinosa del provvedimento in esame riguarda, invece, sicuramente le disposizioni normative relative al cosiddetto scudo penale, che ieri è stato oggetto di particolari critiche in alcuni interventi - mi riferisco in particolare a quelli di ieri - tra i quali quelli del senatore Misiani e soprattutto della senatrice Aurora Floridia. Vorrei tranquillizzare chi ci ascolta: al Governo al Governo non ci sono degli irresponsabili e neppure - addirittura peggio - dei concorrenti nel reato di omicidio. Sarebbe davvero ingiusto che da questo dibattito passasse all'opinione pubblica e ai cittadini di Taranto siffatto messaggio. Per questo dedicherò il mio intervento soprattutto a esaminare e commentare le norme sullo scudo penale. Partiamo dall'articolo 5 del decreto-legge, che ha l'obiettivo di garantire la continuità aziendale tramite il commissario anche nel caso di sanzioni. L'articolo prevede che le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o in parti di essi dichiarate di interesse strategico nazionale, sempre che l'ente elimini le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. È del tutto evidente che si vuole preservare l'attività industriale, coniugandola però con la prevenzione delle fattispecie di reato. L'articolo 6 detta una specifica disciplina in materia di sequestro per la prosecuzione delle attività. In particolare prevede che, ove necessario per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo del lavoro, della salute dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detti le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità. La Commissione giustizia, di cui faccio parte, ha posto in evidenza come la norma in esame non specifichi nel dettaglio su quali provvedimenti amministrativi si deve basare in effetti il giudice nel dettare le prescrizioni. Potrebbe apparire una norma troppo generica, che attribuisce al giudice poteri troppo discrezionali e meriterebbe forse in fase meditativa di essere maggiormente dettagliata per garantire meglio il principio della tassatività penale. con le sentenze nn. 85 del 2013 e 58 del 2018, ha definito imprescindibile un intervento diretto del legislatore per coordinare l'interesse nazionale alla prosecuzione delle attività e l'applicazione di alcuni istituti processuali, quali nella fattispecie il sequestro. L'articolo 7 è sicuramente quello più delicato sotto il profilo normativo. Esso disciplina la responsabilità penale e stabilisce in effetti quello che viene chiamato, in modo più o meno appropriato, scudo penale. Il testo stabilisce che chiunque agisce al fine di dare esecuzione a un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o di parte di esso dichiarato di interesse strategico non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento diretto a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici o se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni. La norma comunque chiarisce che la responsabilità penale è esclusa solo - sottolineo: solo - per fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento diretto a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici e solo quando l'autore abbia agito in conformità alle medesime prescrizioni. Queste due previsioni, peraltro piuttosto generiche nel loro portato normativo, delimitano fortemente la operatività dello scudo. Non possono essere certamente scriminati i comportamenti dolosi, anche se come giurista non posso non cogliere la singolarità e l'asistematicità di questo disposto normativo. Ci si affida sostanzialmente ai princìpi di buona fede e affidamento. Si tratta, comunque, con tutta evidenza, di norme eccezionali che derogano a dei princìpi generali dell'ordinamento penale e come tali non potranno essere estese ad altre fattispecie diverse da quella del tutto peculiare in esame e neppure fatte oggetto di interpretazione analogica. signor Presidente, sono a nostro giudizio giustificate dalla necessità: la prosecuzione delle attività del sito industriale di Taranto è strategica per il nostro Paese; viviamo tempi eccezionali, l'Italia e anche l'Europa hanno necessità di presidiare, oltre alle fonti di approvvigionamento energetico e delle materie prime, anche le produzioni industriali, come nel caso di specie quella dell'acciaio. Purtroppo, il conflitto russo-ucraino ha cambiato completamente i paradigmi e le priorità. Questa guerra sciagurata, che nessuno di noi ha voluto e che si spera possa cessare in fretta, impone all'Italia, ma credo a tutto l'Occidente, di ridisegnare le ragioni di scambio del commercio internazionale. In questo ambito vanno rafforzate e difese a denti stretti le produzioni nazionali di beni strategici. Non a caso, alcune delle norme contenute nel decreto riguardano anche le industrie aeronautiche. Per questo, per garantire agli amministratori delle Acciaierie d'Italia di operare in un contesto di sufficiente serenità normativa, che - ahimè - in precedenza troppo spesso è mancata, una norma come lo scudo penale in esame può trovare giustificazione. Si tratta di un punto di equilibrio certamente complicato, difficile e di non facile individuazione, tra le ragioni della produzione, della tutela dell'ambiente della salute pubblica e dell'occupazione, ma è la soluzione migliore possibile nel contesto dato. Concludo il mio intervento, signor Presidente, sperando che comunque questo decreto possa costituire un passo in avanti decisivo per il risanamento anche ambientale del sito produttivo di Taranto. Forza Italia se lo augura davvero con tutte le proprie forze. *(Applausi).*

ma forse sarebbe più onesto chiamarlo decreto forse salva Ilva. Di certo, esso condanna tutti gli altri, perché è quello che fa. È questa l'ipocrisia di fondo di un decreto che, per salvare un'azienda, un *asset* fondamentale del nostro sistema industriale, ma pur sempre un'azienda, un'azienda, che cosa fa? Abbandona i cittadini di Taranto, calpesta il loro diritto alla salute, condanna i creditori dell'acciaieria, le aziende fornitrici, prende letteralmente a schiaffi l'ordinamento giuridico. Come? con uno scudo penale, un vergognoso scudo penale, trasferendo su Roma tutti i procedimenti che riguardano Ilva, togliendo di fatto ai giudici che lavorano a Taranto la possibilità di fare il loro lavoro, sollevando i giudici tarantini dalla legittima giurisdizione. Signor Presidente, mi assumo la responsabilità di quello che dico. Se questa maggioranza avesse un minimo di onestà intellettuale, utilizzando il registro linguistico che più le appartiene, avrebbe definito questo provvedimento quantomeno anti patriottico. Invece no, nulla di tutto ciò. Del resto, se foste stati capaci di onestà intellettuale, non vi sareste dovuti nascondere e inventare un fantomatico buco di bilancio per distogliere l'attenzione dal pasticcio che state combinando sul super bonus: pasticcio di cui un intero settore industriale vi sta chiedendo conto in queste ore. Ma torniamo al decreto e vediamo le vostre contraddizioni patriottiche. Per ragioni di tempo, signor Presidente, mi limiterò alle due più belle, le più significative. concerne lo scudo penale e la salute dei cittadini. Il decreto ripropone lo scudo penale per gli amministratori. Ebbene, quando parliamo di scudo è normale pensare a qualcosa che ci protegge da una minaccia. Quindi, associarlo a termini quali penale e fiscale, significa che consideriamo o, meglio, considerate giustizia e fisco delle minacce. In audizione in Commissione industria qualcuno è andato anche oltre, vedendo nello scudo penale una misura utile per incentivare gli investimenti esteri in Italia. Certo, è così che dovrebbe funzionare: garantiamo l'impunità, così siamo certi di attrarre investimenti esteri; o comunque, così facendo, evitiamo che scappino. Alla faccia del sovranismo! Del resto, signor Presidente, anche questo depenalizzare per ridurre i tempi della giustizia è un vostro *evergreen*. Logico: come bruciare mezza vigna per ridurre i tempi della vendemmia. Geniale. *(Applausi)*. perché uno scudo penale in questo momento? Stando ai dati, sembrerebbe che sia tutto a posto. Lo stabilimento Ilva rispetta addirittura il 95 per cento delle prescrizioni contenute contenute nella autorizzazione integrata ambientale. Forse non è così e c'è qualcosa che ci sfugge. No, in realtà - e aggiungo - purtroppo, non ci sfugge proprio niente. Il perché è forte e chiaro. Il perché ce lo dice uno studio dell'Istituto superiore di sanità, che ha documentato - non lo ha ipotizzato o nei corridoi - la riduzione del quoziente intellettivo e l'incidenza di disturbi del neuro sviluppo in bambini che vivono a ridosso dell'area industriale di Taranto. La riduzione intellettiva è chiaramente correlata - e anche su questo c'è ampia documentazione - alle sostanze neurotossiche emanate dall'impianto siderurgico di Taranto. *(Applausi)*. Il perché - un altro, l'ennesimo perché - ce lo dice l'Agenzia regionale di protezione ambientale della Regione Puglia, secondo cui le emissioni di benzene dello stabilimento hanno superato di gran lunga il limite consentito per legge. E ancora: il perché ce lo dice addirittura

produce cinque morti all'anno; lo sottolineo: cinque morti all'anno. Ce lo dice la Corte europea per i diritti dell'uomo, che solo nel 2019 ha condannato non una, neanche due, ma ben quattro volte l'Italia per non aver tutelato i diritti dei cittadini di Taranto. Cos'altro deve succedere? Presidente, questa maggioranza, consapevole della situazione, è comunque tranquilla quando garantisce l'impunità penale sui reati ambientali. Salviamo Ilva: questa è la cosa più importante? Questa è la cosa più importante. A salvare i tarantini ci penserà qualcun altro. Per rendere la cosa ancora più deplorevole e grottesca il Governo ha anche previsto che il tribunale competente per le controversie penali sia Roma e non più Taranto; ma sì, in effetti i giudici tarantini potrebbero essere forse troppo di parte? C'è il rischio che non possano giudicare con la giusta lucidità? Insomma, come si dice: lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Acciaierie d'Italia, che evidentemente ci ha visto bene, ha riconosciuto un vento favorevole, il famoso vento da capitalismo occidentesco, piacevole come il maestrale a luglio nella nostra Sardegna. Ha visto bene. Infatti, ha chiesto che l'esautorazione del foro di Taranto in favore di quello romano fosse estesa anche alla controversie amministrative, così, per essere sicuri sicuri. C'è stato anche chi - in preda a un delirio di onnipotenza - ha proposto un'aggiustatina al testo unico degli enti locali, per eliminare la fastidiosissima e irriverente prerogativa del sindaco di Taranto di emanare ordinanze per motivi sanitari. Questo, per fortuna, era troppo anche per voi. Veniamo alla seconda contraddizione patriottica: la gestione dei debiti di Acciaierie d'Italia e la situazione di Sanac, in particolare.

Da qualche tempo, però, Acciaierie d'Italia ha bloccato tutti gli ordini di materiale da Sanac, e non solo: ha anche accumulato nei suoi confronti debiti per oltre 20 milioni di euro. Presidente, qui la situazione è davvero paradossale: abbiamo Acciaierie d'Italia, una società partecipata dallo Stato - la cui quota azionaria è destinata ad aumentare a dismisura, in ragione di questo decreto-legge - che vanta debiti nei confronti di tutti i fornitori, compresa Sanac, anch'essa sotto controllo statale essendo in amministrazione straordinaria. Insomma, lo Stato non paga lo Stato. Per questo abbiamo chiesto che l'erogazione dei fondi pubblici in favore di Acciaierie d'Italia fosse subordinata quantomeno alla garanzia del pagamento dei debiti nei confronti delle società che sono in difficoltà a causa dei ritardi di Acciaierie d'Italia, come Sanac. Il Governo ha bocciato l'emendamento. Acciaierie d'Italia finora non solo non ha previsto un piano di rientro nei confronti di Sanac, ma ha anche bloccato le commesse nei confronti del suo principale fornitore di refrattari e ha cominciato ad acquistare il materiale dai fornitori esteri. Ma perché? perché? Praticamente concediamo a una società a controllo statale un aumento di capitale ingente senza nemmeno chiedere che paghi i fornitori italiani e senza nemmeno pretendere che continui a ordinare i materiali dalle nostre aziende. Veramente per voi tutto questo è normale? Il risultato della vostra illuminata politica industriale è che l'ex Ilva è ben lontana dall'essere salva; le agenzie di questi giorni infatti parlano di fabbrica al collasso, di forni spenti per carenza di materie prime, tra cui - guarda caso - anche il refrattario. Ma allora a che gioco stiamo giocando? E nel frattempo Sanac muore. I rappresentanti sindacali parlano di due o quattro mesi di autonomia. Urgono provvedimenti per ridare liquidità alle aziende; le commesse devono riprendere immediatamente. Parliamo di 350 lavoratori e 350 famiglie, di un'azienda italiana che avrebbe davvero tutte le caratteristiche per essere inclusa tra gli impianti di interesse strategico. Lo abbiamo chiesto e - indovinate? - lo avete negato. Tutto questo per tutelare chi? Un'azienda, Acciaierie d'Italia, in cui lo Stato, in assenza di qualsiasi strategia, continua ancora a iniettare liquidità, mentre la controparte privata - è evidente e chiaro - non ha alcun interesse a vederla prosperare. a vederla prosperare. In sintesi, questo decreto-legge, nella sua formulazione, lo riteniamo vergognoso e lo sarà ancora di più nelle sue conseguenze. Immaginate voi di salvare Acciaierie d'Italia avendo come unica strategia quella di piegarvi a ogni loro richiesta, calpestando il diritto alla salute, alla giustizia, le istanze degli amministratori locali, la sopravvivenza di aziende fornitrici, i lavoratori? Mi chiedo e vi chiedo chi difenderà l'Italia dal vostro ambiguo patriottismo. *(Applausi)*.

colleghi, il provvedimento che oggi approda in quest'Aula è stato contestato da una parte della comunità tarantina e pugliese. Ma io credo che sia indispensabile considerare che il mantenimento in esercizio dello stabilimento ex Ilva di Taranto sia condizione essenziale per alimentare tutti gli altri stabilimenti del gruppo. È per questo, oltre che per il fatto che si tratta del maggior sito produttivo siderurgico italiano, sia per capacità produttiva, sia per dipendenti impiegati, che è considerato sito di interesse nazionale strategico per il nostro Paese. I lavori di ammodernamento tecnologico e gli interventi di riduzione dell'impatto ambientale scontano purtroppo grandi ritardi e così il personale direttamente occupato è in forte contrazione. È necessario tenere sempre a mente che per le attività di esercizio, di manutenzione e di servizio, nonché per le forniture a servizio dello stabilimento tarantino, sono utilizzate in larghissima parte imprese che hanno sede nella Provincia ionica e nella Regione Puglia. Parliamo di aziende del settore metalmeccanico, edile, di trasporto e di servizi che occupano oltre 4.000 lavoratori. d'Italia ha però accumulato pesanti ritardi nei pagamenti di forniture e prestazioni regolarmente erogate che hanno generato gravissime ripercussioni sulla gestione di quelle imprese. Alcune hanno cessato l'attività, altre hanno ridotto drasticamente l'occupazione, altre ancora hanno potuto utilizzare gli ammortizzatori sociali. Ma il risultato è che circa 4.000 famiglie sono in grave difficoltà. È davvero inammissibile che il più grosso gruppo mondiale di produzione siderurgica sia incapace e incapiente nei confronti delle imprese dell'indotto. Il Governo è dovuto intervenire nuovamente per garantire la continuità produttiva dello stabilimento, evitando che l'attuale sequestro degli impianti si protragga pregiudicando definitivamente l'economia della Regione Puglia, e ha trovato un punto di equilibrio tra la tutela dell'ambiente, del diritto alla salute e del diritto al lavoro. Ora - da un lato - bisogna incentivare e rafforzare i processi di riconversione tecnologica mirati alla chiusura delle fonti inquinanti dell'ex Ilva per garantire l'avvio della produzione dell'acciaio pulito e - dall'altro lato - è necessario - come previsto dall'ordine del giorno presentato dai colleghi della Lega Bergesio, Bizzotto e Cantalamessa tutelare le 145 imprese dell'indotto. Le risorse messe a disposizione non devono essere polverizzate dal pagamento dei debiti verso i fornitori energetici, Presidente. Sono le aziende dell'indotto a reclamare il ristoro dei crediti. Almeno una parte di questi fondi deve essere impiegata per tutelare le imprese dell'appalto che hanno garantito la prosecuzione dell'attività produttiva del siderurgico, anche a fronte dei sistematici ritardi nel pagamento delle fatture da parte del committente. Queste ditte ora messe alla porta attendono la ripresa dei cantieri e degli ordini per salvare i propri lavoratori.

impone a tutti noi una riflessione, soprattutto in discussione generale, sul perché siamo arrivati sin qui. Nella discussione generale che si è aperta ieri sera è emerso un tema, soprattutto dai banchi della maggioranza; una maggioranza articolata che ha al suo interno forze politiche che hanno partecipato all'approvazione di altri provvedimenti su Ilva; una forza politica che orgogliosamente rivendica di non averlo fatto nell'ultima legislatura, dimenticando però di averlo fatto nelle legislature precedenti. Ai colleghi della maggioranza vorremmo ricordare un po' di storia di Ilva,

di costruire l'uguaglianza tra due diritti, il diritto al lavoro e il diritto alla salute. Io penso che non ci sia lavoro se non c'è salute e che la storia di Ilva degli ultimi diciassette anni, partendo non casualmente dal 2005, dimostra che, quando si calpesta il diritto alla salute, inevitabilmente non c'è più il diritto al lavoro o esso viene compromesso. Nel 2005, signor Presidente, una mobilitazione civile, senza precedenti, portò all'apertura di una discussione nel nostro Paese sui livelli di diossina prodotti dallo stabilimento di Ilva. ricorderanno i colleghi dell'attuale maggioranza, che lo erano anche allora in Regione Puglia - non c'erano meccanismi di misurazione della diossina. I composti cancerogeni non erano misurabili. Quella mobilitazione portò all'apertura di una prima inchiesta. Fu archiviato tutto dopo un anno. Ricordo questo momento perché io, per una coincidenza della storia, ero commissario liquidatore della città di Taranto alla fine del 2006.

alla quale chiesi banalmente di pagare l'ICI che pagavano i tarantini. Forse molti colleghi non ricordano o non sanno che Ilva insiste su un territorio di Taranto pari a due volte la superficie del territorio in cui vivono 200.000 persone; un terzo della città di Taranto vive in uno spazio che è pari alla metà del territorio della stessa azienda. Quella richiesta che era legittima, perché Ilva pagava un centesimo di ICI di quello che pagava tutta la città, portò allora a una reazione delle forze politiche e anche di alcune forze sociali. La faccio breve: nel 2008 partì l'inchiesta che poi ha caratterizzato in qualche modo la storia non solo giudiziaria, ma anche industriale di questo stabilimento. Lo dico perché noi oggi, colleghi della maggioranza, dobbiamo decidere se rimpallarci le responsabilità o assumerci fino in fondo l'onere di guidare il processo di salvataggio di uno stabilimento che non produce acciaio come dovrebbe. Nel 2012 il gip Todisco diede il via a un percorso che inevitabilmente poi ha caratterizzato alcune inchieste che non sono oggetto di questo confronto. Il primo decreto Ilva lo varò il Governo Monti nel 2012 e diede a quell'impianto lo *status* di impianto strategico nazionale; nel 2015 l'amministrazione straordinaria, nel 2016 fu pubblicato il bando di vendita dell'Ilva. Nel 2017 Mittal vinse una gara; una gara discussa, una gara discutibile in quel momento, una gara per la quale in Parlamento alcuni di noi si alzarono e dissero che non erano d'accordo, nonostante la vicinanza del Governo di allora. Ma il tema era e resta lo stesso: la strategia industriale. Cosa fa l'Italia sull'acciaio? Quali sono i nodi da affrontare? L'acciaio torna a essere quasi di Stato nel 2020. Intanto nel 2021 arrivano le sentenze, per le quali inviterei tutti a guardare i dettagli connessi al legame tra la produzione industriale e l'inquinamento. E arriviamo a oggi.

molti di noi avevano chiesto certezze sull'impatto occupazionale. C'era stato l'impegno per garantire quest'anno un impatto occupazionale pari a 5.000 unità. Come sapete, in questo momento ci lavorano 3.000 unità. In ogni caso, l'aspetto che ha caratterizzato in qualche modo il dibattito e che ci ha portato a presentare gli emendamenti che il mio collega Misiani ieri ha rivendicato è stato cestinato da parte della maggioranza. In questo momento - lo dico al mio collega Melchiorre, che ieri è intervenuto con tanta enfasi e passione - si dovrebbe sapere che l'Afo2 è fermo da luglio; che oggi ci sono solo un'acciaieria e un convertitore; che lo stato impiantistico della struttura è catastrofico; che si cambiano i direttori più di quanto si cambino i Presidenti del Consiglio. Ovviamente auguro al presidente Meloni di non durare quanto i direttori degli stabilimenti di Ilva. Insomma, siamo in una condizione in cui produciamo 3 milioni di euro l'anno e abbiamo 3.000 persone in cassa integrazione, 2.500 solo a Taranto. E gli investimenti paralleli allo stabilimento di Taranto - lo voglio ricordare - sono stati varati dal Governo Conte 2 e riguardano gli investimenti Ferretti, l'ex Yard Belleli, il potenziamento di Grottaglie, gli investimenti di Leonardo, l'Arsenale sul piano Brin, le opere portuali, il Molo polisettoriale. Perché avevamo presentato quegli emendamenti e, sia in sia in Commissione che ieri con Misiani, abbiamo contestato il no del Governo e della maggioranza? L'accordo di programma, sul quale ritorneremo in sede emendativa, Presidente, serviva per riscrivere un piano industriale che tenesse conto delle caratteristiche della città di Taranto. E quella proposta emendativa, che è stata bocciata, ci consentiva di rimettere insieme quel tavolo che ha portato lentamente Taranto a essere una città che ha investito sul passaggio all'acciaio *green* - siamo però ancora fermi - ma nello stesso tempo ha creato le condizioni affinché il funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico avesse un senso rispetto alle finalità che ci eravamo proposti. Così come sul cambio della *governance* abbiamo presentato emendamenti che sono stati respinti, ma ci aspettavamo un sostegno sugli emendamenti che hanno caratterizzato in qualche modo l'idea di una boccata d'ossigeno per le imprese fornitrici di Acciaierie d'Italia; così come per quelli legati alla valutazione di impatto sulla salute. Insomma, presidente La Russa, abbiamo avuto la sensazione che questo provvedimento sia stato fatto per comprare tempo, per prendere tempo, esso non affronti alcuno dei temi che purtroppo hanno caratterizzato la storia dolorosa della città e dello stabilimento, che si lega a doppio filo alla città. Ci auguriamo che, nella discussione che sta per iniziare sugli emendamenti, la maggioranza abbia l'attenzione, la sensibilità e l'umiltà di aprire un dibattito e magari di cambiare idea sugli emendamenti presentati dal Partito Democratico e dalle opposizioni.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, quella del rilancio dell'Ilva, la più grande acciaieria d'Europa, è una delle questioni più delicate e da tenere maggiormente in conto nel nostro Paese, sia dal punto di vista dello sviluppo strategico industriale, sia della tutela e del recupero ambientale, che della salvaguardia dell'enorme capacità occupazionale che l'impianto sviluppa e può ancora sviluppare. Sono state prese molte misure per rilanciare il polo produttivo, fiore all'occhiello mondiale della nostra industria pesante per decenni, su cui ruotano migliaia di lavoratori tra dipendenti diretti e dell'indotto e la cui vendita di acciaio nel 2021 si è comunque attestata oltre i 3 miliardi di euro. L'obiettivo del provvedimento sugli impianti strategici è tutelare tutte quelle imprese ritenute strategiche per il nostro sistema economico nazionale, tra cui quello dell'Ilva, ora Acciaierie d'Italia. L'impianto Ilva è stato, suo malgrado, protagonista negativo negli ultimi undici anni di una storia tanto travagliata quanto ora ingarbugliata. Nel corso del tempo i Governi che si sono succeduti hanno iniettato fondi e dotazioni importanti per evitare che l'impianto più grande d'Europa fallisse. L'intera struttura è stata nel frattempo acquistata dal colosso dell'acciaio ArcelorMittal. Lo Stato italiano per mezzo di Invitalia, l'agenzia governativa italiana che si occupa degli investimenti dello Stato, entra in gioco e ad oggi possiede il 38 per cento del capitale. Stante la complessità del *dossier* sull'Ilva, il presente provvedimento non sarà quello che metterà fine a questa annosa questione e lo sappiamo, ma rappresenta un primo impegno del Governo in quella direzione. In questo momento la principale urgenza e necessità è la stabilità dell'occupazione, al fine di garantire la produzione, evitando di compromettere irrimediabilmente l'attività di Taranto per poi poter pianificare un serio e definitivo piano di riconversione ambientale. A chi accusa il Governo di avere iniettato l'ennesimo fondo per salvare Mittal, rispondo che purtroppo i debiti ci sono e la situazione si è ulteriormente aggravata a causa dello *shock* dei prezzi dovuto alla crisi russo-ucraina e alla pandemia. Ciò che si va a salvare è l'intero sistema di produzione. Invitalia, infatti, è autorizzata a sottoscrivere e a erogare finanziamenti in conto soci da convertire in aumento di capitale sociale, in modo da permettere allo Stato italiano di avere più voce in capitolo. La riconversione di un'azienda, però, la si fa se l'azienda è ancora in piedi. Altro obiettivo prioritario in questo momento è snellire l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, fornendo la possibilità di richiesta, anche in caso di inerzia degli amministratori, al fine di garantire una maggiore tutela. Allo stesso modo, è una misura di buon senso prevedere un parametro per calibrare il compenso remunerativo per l'attività di gestione, al fine di promuovere una maggiore efficacia, efficienza ed economicità. È stato pertanto doveroso prevedere il tanto discusso strumento cosiddetto di immunità penale, un sistema che garantisce la prosecuzione delle attività del sito, adottando un bilanciamento tra le esigenze di continuità produttiva e la tutela della salute e dell'ambiente. Per questo è stato ripristinato lo scudo penale, una misura introdotta dal Governo Renzi e poi temporaneamente congelata per dare attuazione al principio che chi ha in gestione l'attività non deve incorrere in eventuali azioni penali, in virtù del fatto che il loro operato è indissolubilmente legato all'attuazione di prescrizioni stabilite prima della loro nomina. Il provvedimento quindi recepisce le urgenze attuali, le principali criticità e le traduce in misure concrete. Viene poi il miglioramento della sostenibilità, così come le misure che più nel dettaglio andranno a definire il ripristino e il recupero dell'impianto dal punto di vista della riconversione ambientale, con il fine ultimo di accompagnare l'impianto verso una riqualificazione, che vedrà l'ex Ilva alimentata solo da idrogeno verde. Bisogna utilizzare le risorse e le energie guardando all'ambiente, all'economia circolare, alla trasparenza, alle comunità locali, e per fare questo servono una pianificazione, un cambio di passo e una gestione che sia il frutto di una visione a lungo termine; in due parole, serve una pianificazione strategica. Quello che il Governo auspica è poter intavolare una seria discussione, al fine di trovare insieme una soluzione a uno dei *dossier* più importanti e delicati del nostro Paese. Il fatto che, nel corso del tempo, i vari Governi si siano alternati nel tentativo di porre rimedio e tutelare l'impianto, i lavoratori e le famiglie è un segnale che la questione è ampiamente e largamente ritenuta come delicata, e pertanto va risolta al più presto. L'attuale Governo ha dato prova di sensibilità all'ascolto e disponibilità al dialogo, e per quello che ci riguarda non ha precedenti. L'opposizione in tutto questo ha un ruolo importantissimo: non si deve limitare a fare un'opposizione di tipo conflittuale, perché ha un chiaro mandato democratico, ossia quello non solo di fornire rappresentanza a tutti a beneficio del pluralismo, ma anche di contribuire alla realizzazione dei provvedimenti a vantaggio della collettività intera. L'occasione che si presenta in questo momento è forse quella giusta per tentare insieme, al di là del colore politico e delle ottuse logiche legate agli steccati di partito, di mettere la parola fine a questa matassa. Concediamo finalmente ai lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto una certezza occupazionale intangibile. Assicuriamo ai tarantini a tutti i miei corregionali che ivi lavorano, che frequentano e vivono la splendida Taranto, il diritto non ammalarsi di tumore più che in ogni altro luogo d'Italia. Garantiamo che un lavoratore dell'area non debba mai più essere esposto ad infortuni mortali maggiormente che in ogni altro luogo di lavoro della civile Europa. *(Applausi)*. Solo battendoci nel senso indicato Solo battendoci nel senso indicato dalla Costituzione e dal giudice delle leggi, cioè contemperando un equilibrato bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, perseguiremo l'obiettivo del rilancio della nostra industria pesante, anche attraverso la qualità del *made in Italy*, con il ritorno a quello che era definito il migliore acciaio del mondo, la stabilità occupazionale e, non per ultimo, la serenità che Taranto aspetta ormai da troppo tempo.

Il 22 febbraio 2021, vicino alla città di Goma, in Congo, mentre viaggiavano su un convoglio delle Nazioni Unite, vennero barbaramente assassinati l'ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista del World food programme Mustapha Milambo. Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci erano due giovani italiani che, con coraggio, generosità e passione, rappresentavano l'anima migliore della nostra Nazione all'estero. Luca era stato insignito del Premio internazionale Nassiriya per la pace nel 2020, mentre Vittorio è stato insignito della Medaglia d'oro al valor militare alla memoria. La loro missione, così come quella di tanti altri rappresentanti della diplomazia e delle Forze armate, appare ancora oggi fondamentale per garantire alle popolazioni civili di diversi luoghi del Pianeta - in quel caso era l'Africa - quei diritti che dovrebbero essere alla base di qualsiasi civiltà e di qualsiasi società. Un impegno, il loro, svolto nella loro vita con una dedizione al sostegno degli ultimi, che rimane un vero e proprio insegnamento civile. Li ricordiamo oggi con l'ammirazione che si deve agli eroi morti nel nome della Nazione, o più semplicemente a chi ha dato la vita per adempiere al proprio dovere e per contribuire a portare la pace nel mondo. A loro, alle loro famiglie, al corpo diplomatico, all'Arma dei carabinieri va il nostro commosso ricordo. Vi invito ad osservare un minuto di silenzio in loro memoria.

La Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento,

Grazie,

decreto-legge, che abbiamo definito pessimo. Con riferimento a Sanac, le cui sorti sono direttamente legate a quelle di Acciaierie d'Italia, abbiamo chiesto sostanzialmente due cose: in primo luogo, come ho detto poco fa nel mio intervento, abbiamo richiesto che Sanac venisse ricompresa tra gli stabilimenti dichiarati di interesse strategico, insieme ad Acciaierie d'Italia. Gli impianti produttivi di Sanac, infatti, danno lavoro a circa 350 persone, escluso l'indotto. Sanac aveva e dovrebbe avere come suo principale cliente l'ex Ilva di Taranto. In aggiunta, i territori interessati dai siti produttivi Sanac vivono situazioni di difficoltà strutturale che richiedono tutte le attenzioni di un Governo veramente votato al mondo delle imprese, se così è. Fate finta di avere a che fare con le squadre di calcio e provate a mettere su Sanac, Assemini, Gattinara, Vado Ligure e Massa Carrara lo stesso impegno che avete messo nel trovare le risorse per rateizzare i debiti della serie A. luogo, Sanac rappresenta il 35 per cento del mercato nazionale dei materiali refrattari, materiali indispensabili, essendo una produzione legata al processo produttivo dell'acciaio. Il nesso logico tra le due filiere è lampante: Sanac è parte integrante della filiera dell'acciaio e, quindi, andrebbe considerata La seconda cosa che abbiamo provato a richiedere è che i nuovi apporti di capitale di Invitalia nei confronti di Acciaierie venisse subordinata al pagamento dei debiti di ADI nei confronti di Sanac: una richiesta di assoluto buon senso, che avrebbe dovuto essere superflua, ma evidentemente non lo è. Infatti avete bocciato tutti i nostri emendamenti tranne uno; un emendamento speculare al nostro, ma presentato da un membro della vostra maggioranza, il senatore Bergesio, che evidentemente è sensibile al buon senso, infatti in Commissione lo avete invitato a ritirare l'emendamento. Quindi delle due l'una: o non capite nulla di filiere industriali (lo dico con umiltà e rispetto) e proponete decreti-legge tirando fuori dal cilindro idee fantasiose di politica economica, o siete semplicemente asserviti ad ArcelorMittal, tanto da preferire che questo colosso dell'acciaio continui a rifornirsi di materiale refrattario sul mercato internazionale, a discapito delle imprese italiane. Vorrei ricordare che il *made in Italy* in Italy* si diffonde con le norme, non con gli slogan. Capiamo che vi risulti difficile ascoltare le opposizioni: appena ne avete il sentore vi opponete con un riflesso condizionato, tanto che scambiate anche i vostri membri. A proposito, signor Presidente, se il senatore Bergesio vuole, tra le nostre file c'è spazio per chi comprende la situazione di difficoltà delle imprese, solo per loro. Tuttavia, se questa maggioranza non vuole ascoltare le opposizioni, quantomeno ascolti i lavoratori. A tal riguardo, signor Presidente, faccio un appello ai colleghi senatori ai colleghi senatori sardi, toscani, piemontesi e liguri. Colleghi, andate a spiegare il decreto-legge salva Ilva davanti ai cancelli degli stabilimenti Sanac del vostro territorio che chiuderanno tra aprile e giugno; andate a spiegare perché avete bocciato gli emendamenti che avrebbero salvato il loro gruppo. Se avete deciso di condannare i lavoratori di Sanac, non dovete dirlo a me, Sabrina Licheri del MoVimento 5 Stelle, ma alle famiglie che state condannando alla cassa integrazione quando andrete ad elemosinare qualche voto per le prossime elezioni. Ripensateci. *(Applausi.

Presidente, entriamo nel merito delle questioni. Abbiamo proposto di eliminare la reintroduzione dello scudo penale, ma ci avete detto di no; abbiamo proposto di reintrodurre il vincolo del dissequestro, ma ci avete detto no, per cui adesso state finanziando degli impianti posti sotto sequestro, con il rischio di confisca e che ancora oggi producono danni alla salute e all'ambiente. Avete detto di no anche ad una riconversione *green* di quegli impianti, per cui oggi esiste il rischio che questi due miliardi vadano in un mare senza fondi, senza una garanzia di ottenere

Abbiamo anche proposto di inserire e qualificare le imprese dell'indotto come strategiche, ma ci avete detto di no. Nel 2015 quelle stesse imprese hanno subito un danno di oltre 100 milioni di euro.

un'impresa che ha prodotto sempre perdite, cassa integrazione, danni all'ambiente e morte dei cittadini di Taranto. Vi state assumendo una responsabilità senza fine. *(Applausi).* Comunico che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo

Signor Presidente, nel primo emendamento che come Partito Democratico poniamo all'attenzione c'è molto dell'impostazione che riteniamo doverosa per uscire da una condizione assolutamente negativa della produzione di acciaio nel nostro Paese. Anche in questi ultimi anni, in tutto il mondo occidentale e non solo tutte le aziende che producono acciaio hanno avuto grandi guadagni, noi siamo riusciti, attraverso Acciaierie d'Italia, a essere in perdita. Abbiamo diminuito di circa un terzo la produzione di acciaio - tra l'altro, parliamo di acciaio che si è sempre caratterizzato per essere di alta qualità nella più grossa acciaieria d'Europa, che ha sede nel nostro Paese, che coinvolge Taranto come sito industriale, ma non solo perché ha diversi siti industriali. I dati sconcertanti dal punto di vista ambientale - ma non ridiamo, né sorridiamo nemmeno per i dati occupazionali, espressi prima nell'intervento del collega senatore Boccia - ci - ci dicono che, in questi ultimi dieci anni, quando molto spesso ci siamo dovuti occupare di produzione di acciaio nel nostro Paese, e in modo particolare di Ilva, siamo riusciti a non fare passi avanti né per quanto riguarda il risanamento ambientale, né per quanto concerne la qualità dell'occupazione e purtroppo nemmeno per quanto attiene alla produzione di acciaio in Italia.

Cosa è mancato? È mancato un piano industriale degno di questo nome - e ancora oggi non lo abbiamo, drammaticamente che è l'unico strumento per garantire produzione di qualità e anche occupazione di qualità. Non è un caso che in Acciaierie d'Italia, come peraltro in molte imprese italiane, siano notevoli - per numero, per consistenza, per drammaticità anche gli infortuni e le morti sul lavoro. Siamo riusciti in questi anni ad avere una continua litigiosità, uno scontro terribile, anche tra le istituzioni. Abbiamo bisogno che con questo decreto-legge si cambi rotta, che davvero la nostra produzione torni a essere degna di questo nome, con qualità; che il lavoro sia di qualità e che il tema di dover scegliere tra salute e lavoro non si debba più porre come un'alternativa; anzi, al contrario, attraverso il contributo di tutti si sciolga questo nodo. E c'è un unico strumento che garantisce questo: l'accordo di programma. Non mi so dare spiegazione di contrarietà. Se c'è uno strumento di partecipazione e di responsabilità tra le parti sociali, l'impresa, le rappresentanze dei lavoratori, ma anche tutti i livelli istituzionali, dal Governo ai Ministeri, al Comune alle Regioni a tutti gli interlocutori, è proprio l'accordo di programma. Non volere questo significa non volere fare passi avanti insieme nel rispetto del lavoro, dell'economia del Paese, della salute dei cittadini e anche della dignità di un territorio. Allora io faccio un appello a tutti quelli che ritengono, come me, che la produzione di acciaio sia importante, che la qualità dell'occupazione sia valore aggiunto e la salute sia garantita. Facciamo il patto...

**Il Senato non approva**.

Avevo già fatto un intervento in quest'Aula invitando tutti i colleghi a porre la massima attenzione perché parliamo di aree di crisi industriale della Sicilia, suol dire, a gravi crisi dovute al mercato nazionale ed internazionale. Per Termini Imerese parliamo di Fiat, per l'area di Gela parliamo di Petrolchimico, un altro stabilimento di interesse nazionale strategico che ora è diventato il primo polo nazionale per la produzione di carburanti verdi. Pertanto, Presidente, come Gruppo MoVimento 5 Stelle, voteremo a favore degli emendamenti in questione, auspicando che il Governo possa continuare a porre la massima attenzione anche ai tanti emendamenti dell'"opposizione" perché noi lavoriamo per il bene della Nazione. Le questioni di parte le lasciamo ad altri lidi. Grazie, Presidente, confermo il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

non si tratta di ravvedimento operoso. Avevamo preso come Governo e come maggioranza un impegno e al primo provvedimento utile abbiamo risolto la questione,

Grazie aver dimostrato questa volta oggettivamente amore per questa Nazione. Lo stesso amore che abbiamo dimostrato noi e anche il Governo, come giustamente anticipava il senatore Damiani, relativamente al tentativo

i membri del Governo che hanno lavorato con noi in Commissione, la sottosegretario Bergamotto e la sottosegretario Siracusano che si è da subito spesa perché su questo emendamento

usati da alcuni rappresentanti, che qui stiamo parlando di 992.000 euro per tutte le aree di crisi complessa. *(Applausi)*. Non stiamo facendo un intervento di politica industriale capace di migliorare la situazione complessa di molte aree di crisi del nostro Paese.

un accordo di programma, che preveda innanzitutto la chiusura delle fonti inquinanti e la destinazione delle ingenti risorse pubbliche alla realizzazione di impianti ecosostenibili, unitamente a una serie di tutele a favore dei lavoratori e delle imprese dell'indotto, nonché l'introduzione

l'emendamento che ho proposto fa riferimento all'articolo 6 del decreto.

fra l'autonomia dell'attività dell'autorità giudiziaria e l'autonomia dell'intervento di politica, del Governo. Quello che qui avviene è che si disegna un percorso paradossale perché, se da una parte sembra aumentare l'autonomia della magistratura, dall'altra trasforma l'autorità giudiziaria in un decisore politico, in un decisore di *policy*, in qualcuno che non deve soltanto valutare

di disincagliare il sequestro e nominare un commissario, c'è un ricorso che può essere fatto dal Governo. Pertanto tutta questa vicenda si risolve in una *litigation* di carattere giudiziario. Nell'emendamento che proponiamo, invece, in pieno rispetto della decisione della Corte costituzionale, noi separiamo la parte che riguarda l'autonomia del Governo da quella riguardante l'autonomia della magistratura e del giudice. Sostanzialmente, prevediamo che ci siano dei commissari nominati dai Ministeri competenti e dei commissari nominati dall'autorità giudiziaria e che di concerto definiscano le prescrizioni e quell'equilibrio tra tutela dell'ambiente e tutela dell'occupazione e dell'interesse nazionale che è di rilievo.

Il problema che si pone con questa formulazione del Governo è che si sta introducendo una normativa di carattere generale, per cui sostanzialmente di fronte a qualunque sequestro c'è una discrezionalità del Governo a definire *ex post* cosa sia un impianto di interesse strategico nazionale. Quindi non c'è prima una definizione di interesse strategico nazionale e poi un'attività di indagine e di sequestro, ma il processo contrario, generando un'incertezza rispetto alla quale si confondono gli ambiti dell'autorità giudiziaria e quelli dell'autorità politica. Questo è già avvenuto perché,

Non è il caso Ilva. Noi stiamo applicando questa norma molto forte che riguardava il caso Ilva a casi molto più piccoli rispetto ai quali qualunque cosa può essere interesse strategico nazionale. Si crea un *vulnus* tra due piani di autonomie e si fa politica industriale attraverso questo meccanismo, generando incertezza.

Signor Presidente, in merito al principio introdotto dal Governo sul bilanciamento tra diritti costituzionali,

cui noi dobbiamo decidere cosa sacrificare della salute umana e di un altro diritto costituzionale, che è la tutela ambientale, per garantire la continuità produttiva. Per noi, Presidente, la vita umana

già trovato risposta in diverse sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione a sezioni unite.

intervengo in merito ad una norma assurda, che sicuramente sarà oggetto di attenzione da parte della Corte costituzionale. Noi chiediamo l'eliminazione della previsione per cui la Presidenza del Consiglio possa impugnare il provvedimento del giudice in cui si procede a non autorizzare la continuità dell'attività produttiva dannosa per l'ambiente e per la salute. Si rischia, infatti, un conflitto tra poteri dello Stato, nel senso che il Governo, tramite la Presidenza del Consiglio, va ad impugnare un provvedimento della magistratura, peraltro trasferendo al foro di Roma la decisione. Un vero e proprio disastro giuridico quello che state compiendo, che sarà oggetto sicuramente di attenzione da parte della Corte costituzionale.

Presidente, noi chiediamo innanzitutto di sopprimere l'articolo 7, che in particolar modo introduce lo scudo penale, norma che era stata eliminata dal Governo Conte 2 e che adesso viene ripristinata. Quindi, viene ripristinata una zona franca di impunità giuridica. Si ripristina, in sostanza, il cosiddetto diritto di uccidere, che sicuramente sarà oggetto anch'esso di attenzione della Corte costituzionale, così come era già avvenuto ante 2019, allorquando la Corte costituzionale si stava pronunciando su questo scudo penale. Voi oggi, a distanza di anni, lo state reintroducendo per un'azienda che crea danni all'ambiente e alla salute. Chiediamo, dunque, ancora una volta, di ravvedervi su questo provvedimento.

Ce ne sono state molte, rispetto all'Ilva, di occasioni difficili rispetto alle quali trovare le soluzioni: questa è una di quelle. Credo che dovremmo tutti provare a ragionare sul fatto che continuare a finanziare - così come si sta facendo un attore privato, senza che questo determini risultati positivi, forse non è la soluzione migliore. Soprattutto, non è la soluzione migliore creare le condizioni per cui si determinano precedenti che poi varranno anche per altre occasioni, oltre che per quell'azienda. Il settore siderurgico non brilla per essere un comparto a grande sicurezza del lavoro; è purtroppo uno di quei settori dove gli incidenti si ripetono, e spesso sono mortali. Lo stabilimento di Taranto non fa eccezione da questo punto di vista: ha una storia molto difficile, anche durante tutte le situazioni che si sono determinate dopo i sequestri, le amministrazioni straordinarie e così via. Allora, davvero stupisce l'idea che si reintroduca uno scudo penale che prevede anche lo scudo, l'impunibilità rispetto alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Non va bene dire che un'azienda può ricevere prescrizioni differenti da quelle che già la legge prevede rispetto alla salute e alla sicurezza sul lavoro, alla salute e alla sicurezza sul lavoro, che non è solo la norma generale, ma è l'insieme dei provvedimenti che si prendono e che si devono determinare in qualunque situazione di ristrutturazione, riorganizzazione e avviamento degli impianti. Peraltro, come già veniva citato e ricordato dai miei colleghi, la Corte costituzionale e la Corte europea ci hanno già detto che la salute e la sicurezza del lavoro non possono essere sottoposte a scudo penale. E vorrei dire a quest'Assemblea che noi saremo un Paese normale quando un'azienda non chiederà mai lo scudo penale per la salute e la sicurezza sul lavoro *(Applausi)*, perché quell'azienda dovrebbe sapere che garantire la salute e la sicurezza sul lavoro è una delle condizioni per la qualità della sua produzione e per la risposta agli impegni. Capisco davvero che questa maggioranza ha una grande difficoltà a mettere mano a qualunque provvedimento come se i suoi equilibri venissero meno ogni volta che si prova a migliorare un testo che viene presentato, in un Paese che continua ad avere 1000 morti all'anno sul lavoro, che ogni volta che c'è un morto sul lavoro si impegna a dire che farà chissà quali cose e poi non succede niente, il regalo che fa al Paese, rispetto ai grandi impianti strategici, è la moratoria e lo scudo penale sulla sicurezza sul lavoro? certi che è questa la risposta che stanno chiedendo i lavoratori che si domandano cosa vogliamo fare rispetto a una strage continua? Non capisco cosa vi costi dire seriamente che, se ci possono essere ragioni di scudo penale rispetto ai provvedimenti che la magistratura propone, siano escluse la salute e la sicurezza sul lavoro, perché escluderle vuol dire dare un segnale a quei lavoratori che hanno una prospettiva, perché escluderle vuol dire che l'insieme di questo Paese vuole porre fine alla strage sul lavoro, e che la salute delle persone viene sempre prima delle ragioni del profitto di una riorganizzazione o di qualunque altra ragione. Non farlo è il peggior messaggio che oggi questo Parlamento potrebbe dare al Paese, che pure ha un gravissimo problema di salute e di sicurezza sul lavoro; ma è anche un gravissimo segnale rispetto al futuro di uno stabilimento strategico come l'Ilva, perché diciamo che potrà continuare a operare senza alcuna attenzione alla salute e alla sicurezza di chi in quello stabilimento opera.

Con riferimento all'articolo 8, facendo riferimento non a una nostra posizione ideologica,

a tutela dell'ambiente e della salute, che si collegano anche con l'obiettivo della transizione ecologica per l'energia e della sostenibilità.

a produrre e si inserisce solo la valutazione del danno sanitario *ex post.* Quello che chiediamo è di passare da una valutazione *ex post* ad una valutazione *ex ante*. Non possiamo prima andare a calcolare i morti e le malattie per poi intervenire: cerchiamo di prevenire i danni all'ambiente e alla salute. Chiediamo quindi da una parte l'introduzione della in sede di autorizzazione integrata ambientale, modificando il codice dell'ambiente, e dall'altra parte di modificare e rettificare i limiti degli inquinanti previsti dal decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010. L'OMS li ha dichiarati elevati rispetto a quelli tollerabili dall'essere umano.

su indicazione ben precisa, relativa ad Acciaierie d'Italia, ma il resto è molto importante. Qui stiamo parlando di aziende strategiche per il loro *core business* e per la loro attività, che hanno avuto un problema enorme dal punto di vista dei consumi energetici. Avere la possibilità, entrando nel sistema strategico, di essere considerate energivore

dei prezzi dei prodotti che vendono nei confronti dei consumatori. La misura era inserita in un emendamento presentato in Commissione, che poi abbiamo trasformato in ordine del giorno, in quanto non è stato possibile reperirne la copertura, e qui ringrazio la sottosegretaria Bergamotto per la sua attività. Siamo riusciti comunque a contemplare questo questo particolare momento di presa d'atto perché diventi importante anche nei provvedimenti futuri che andremo ad approvare.

soprattutto forme di tutela a favore del quartiere dei Tamburi di Taranto, dove vivono, Presidente, oltre 40.000 persone. Invito pertanto la maggioranza, ma soprattutto il Governo e il ministro Urso (che è qui presente in Aula), a venire a fare una passeggiata al quartiere Tamburi e a vedere tutte le targhe che i cittadini di quel quartiere affiggono di fianco

che il Ministero vorrebbe lavorare con le istituzioni, innanzitutto con il Comune di Taranto, alla definizione di un accordo di programma. Come mai lei parla di questa svolta? E perché oggi non è stato espresso parere favorevole sugli emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 1 e all'articolo 8, volti proprio alla definizione di una cabina di regia istituzionale, della quale devono far parte le amministrazioni centrali e locali e le organizzazioni economiche e sindacali del territorio? Vede, Ministro, c'è una differenza tra voler proporre qualcosa, magari annunciarla e poi esprimere un parere contrario sugli emendamenti che abbiamo presentato. bastava dare un parere favorevole all'emendamento del Partito Democratico. Vede, c'è anche una seconda differenza. Con questi emendamenti abbiamo voluto dare un riconoscimento pubblico abbiamo voluto dare un riconoscimento pubblico e legislativo a un'area che ha già pagato un prezzo così alto e di cui adesso andava garantita la specialità, inserendo per legge l'accordo di programma.

di questo Governo e dal nostro punto di vista - cosa ancora più grave - di un ennesimo provvedimento che, con la modalità della decretazione d'urgenza, interviene sull'Ilva di Taranto, ancora una volta omettendo di affrontare il problema alla radice ed evitando di ricercare soluzioni strutturali per quello che ormai può essere considerato a tutti gli effetti un contrasto irrisolvibile. Da una parte, c'è l'interesse della produttività, con le evidenti ricadute economiche sul nostro Paese e, dall'altra, la salute delle persone e il diritto di una comunità a vivere a vivere in un ambiente sano. Questo decreto-legge purtroppo è un'ennesima pezza, com'è stato detto anche in diversi autorevoli interventi in discussione generale, e posso dire di condividere questo tipo di impostazione. Esso introduce, peraltro, norme poco chiare e assai generiche, ambigue nella formulazione, carenti sotto il profilo della coerenza sistemica credo, da questo punto di vista, anche a rischio di illegittimità costituzionale, come peraltro proprio a proposito dell'Ilva è già accaduto in passato. Quello che si è cercato di fare - male - è facilitare la produzione, restringendo l'ambito di applicazione delle sanzioni interdittive e del sequestro conservativo. L'intento del Governo appare assai chiaro: garantire la continuità produttiva dell'Ilva, evitando che l'attuale sequestro degli impianti ritenuti pericolosi per la salute e per l'ambiente si protragga, pregiudicando l'acquisto degli impianti. esclude l'applicazione delle sanzioni interdittive nel caso di stabilimenti di interesse strategico nazionale sulla base di una vera e propria condizione presuntiva, come se bastasse cioè la scelta di un modello organizzativo astrattamente idoneo per prevenire la possibile violazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. Come ben si comprende, la norma crea una precondizione in base alla quale il modello organizzativo scelto risulta essere idoneo per definizione e quindi, adottato il modello, decadranno tutte le forme di responsabilità per la lesione della salute e per la sicurezza dei lavoratori. Signor Presidente, a me pare molto grave, cosa che il successivo articolo 6 peraltro conferma, anteporre l'interesse nazionale alla prosecuzione dell'attività dell'impresa oggetto del sequestro, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, mentre i successivi articoli 7 e 8 reintroducono lo scudo penale, sancendo una sorta di presunzione assoluta di diligenza e quindi di non punibilità delle condotte che autorizzano l'attività produttiva, eludendo in questo modo le pronunce della Corte costituzionale. Proprio la Corte, come sappiamo, ha ritenuto più volte che non possano essere oggetto di bilanciamento l'attività industriale, da una parte, e la sicurezza dell'ambiente e della salute dei lavoratori, dall'altra, come peraltro ci dicono in maniera molto evidente gli articoli 2 e 32 della Costituzione italiana. Credo che non sia davvero accettabile oggi, dopo dieci anni dal sequestro degli impianti,

coinvolti non siano inconciliabili, ma debbano all'opposto andare di pari passo: il lavoro dovrebbe sempre avvenire in condizioni di sicurezza per la salute del lavoratore stesso

Non c'è alcuna traccia di progetti di riconversione e non ci sono risorse per le bonifiche, né interventi concreti per un territorio che aspetta risposte reali. Non c'è nulla su un piano industriale che possa dare garanzie sul fronte ambientale, né su quello sanitario e lavorativo, men che mai un piano concreto che consenta il reintegro dei lavoratori ex Ilva in cassa straordinaria o che garantisca per lo meno di lavorare con dignità. La vicenda industriale e ambientale, lo sappiamo bene, è assai assai complessa e anche onerosa, ma a maggior ragione sarebbe stata necessaria una maggiore complessità, ad esempio - lo dico ancora una volta rammaricandomene molto entrando nel merito degli emendamenti dell'opposizione, che spesso erano semplicemente e soltanto di buon senso, ma che, ciononostante, sono stati sistematicamente ignorati, esattamente come non sono state ascoltate le osservazioni proposte dalle parti sociali in audizione nelle scorse settimane. Non è stata tenuta in nessuna considerazione la richiesta dei sindacati, ad esempio circa il cambio della *governance* e l'introduzione di un vincolo di destinazione sui soldi pubblici, in modo che possano essere utilizzati per un chiaro processo di transizione ecologica e sociale. Non c'è niente sul futuro dei lavoratori, come accennavo. Il Governo sembra essersi dimenticato di di quelli rimasti in Ilva in amministrazione straordinaria, per i quali si chiede il rispetto dell'accordo del 2018.

che peraltro nella nostra ottica non possono che essere la stessa cosa. Mi pare di poter dire che il vostro e quello del Governo sia null'altro che un via libera per continuare ad ignorare i disastri ambientali e ad inquinare. Per tutte queste ragioni, noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra voteremo convintamente contro questo decreto-legge sbagliato.

Signor Presidente, ancora una volta ci troviamo a trattare un provvedimento che il Governo è stato costretto ad adottare in via d'urgenza per far fronte alle gravi conseguenze della crisi energetica che, investendo duramente le imprese operanti nel nostro Paese, Paese, ha generato una significativa riduzione della liquidità, che non può essere sottovalutata, con riguardo ai contesti industriali di rilievo strategico nazionale. Come già il precedente decreto-legge n. 187 del 2022, il Governo è riuscito ad agire tempestivamente, perseguendo, attraverso una proficua allocazione delle risorse, il massimo bilanciamento tra le esigenze di protezione della salute e dell'ambiente e quelle di tutela dell'occupazione e della produzione. parametri, questi, che costituiscono il metro di giudizio dell'azione amministrativa di un Governo efficiente ed efficace. Anche questa volta, questo Esecutivo e questa maggioranza hanno voluto mettere al centro della propria azione l'interesse nazionale, garantendo la tutela dei lavoratori,

con cui si sono messe in sicurezza aziende operanti nei settori strategici del nostro Paese, fornendo allo Stato strumenti più celeri per intervenire a fronte di gestioni disfunzionali rispetto all'interesse nazionale. Venendo al merito del provvedimento in esame e proprio in relazione all'impianto siderurgico di Taranto, grazie a questo intervento potranno essere finalmente approntate le misure di rafforzamento patrimoniale necessarie a garantire la permanenza dell'azienda e la sua competitività sul mercato. Voglio cogliere l'occasione per apprezzare pubblicamente le prospettive indicate dal ministro delle imprese e del *made in Italy* Adolfo Urso per il lancio industriale e la riconversione ambientale del sito siderurgico pugliese, anche in considerazione dell'ottima proposta di perseguire un accordo di programma per reindustrializzare quell'area di Taranto. Realizzare il polo siderurgico *green* più grande d'Europa renderà queste acciaierie un modello per tutto il mondo. Tornando alle misure contenute nel decreto, voglio citare anche altri interventi a nostro avviso meritevoli di plauso in questa sede. Il rafforzamento del ruolo del socio pubblico, anche in minoranza, nelle grandi imprese di interesse strategico nazionale, soprattutto nel caso di inerzia degli amministratori, è fondamentale e prioritario. Condividiamo in tal senso le disposizioni che consentono l'accesso all'amministrazione controllata direttamente su istanza del socio pubblico, perché semplificano una procedura in cui la tempestività gioca un ruolo di primo piano nella salvaguardia delle strutture aziendali. Consentire di fatto allo Stato di intervenire anche di fronte all'inerzia degli amministratori, sussistendo un fondato pericolo, eviterà infatti l'aggravarsi di situazioni di dissesto o di danno. Voglio anche evidenziare la delicatezza e l'attenzione con cui si è deciso di intervenire sul tema del delicato bilanciamento tra gli strumenti giuridici collegati all'esistenza di un procedimento giudiziario e la tutela della continuità dell'attività di un'impresa di interesse strategico nazionale. Non può infatti sottacersi come le risultanze delle attività giudiziarie o i vincoli posti alla disponibilità dei beni strumentali, come il sequestro, possano determinare danni significativi e talvolta irreparabili alle imprese coinvolte, che nel caso in cui agiscano in determinati settori possono però riverberarsi anche sul sistema economico nazionale, pregiudicando coesione sociale e soprattutto occupazione. Ebbene, pur garantendo lo svolgimento dell'eventuale giudizio, si è giustamente voluta salvaguardare la prosecuzione dell'attività dell'impresa, limitando, da un lato, l'applicabilità delle sanzioni interdittive e delle misure cautelari previste dal decreto legislativo n. 231 del 2001 e, dall'altro, temperando gli effetti del sequestro, valorizzando il principio della continuità aziendale. Concludo, auspicando che su questo provvedimento, contenente prima di tutto norme di buon senso, possa esservi la massima convergenza di quest'Assemblea. Per questi motivi, il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia esprimerà con convinzione il voto favorevole a questo provvedimento. Signor Presidente, con il voto di oggi ci accingiamo a scrivere l'ennesimo capitolo legislativo della vicenda ex Ilva. Ho provato a contare il numero dei decreti-legge che hanno riguardato questo tema e devo dire che è stato un esercizio complicato: credo che siano circa una dozzina e già questo è indice di una seria difficoltà, direi di una malattia che affligge il nostro Paese, che non riesce a dotarsi di una vera e propria politica industriale e procede di emergenza in emergenza, di decreto in decreto, lasciando sullo sfondo giudizi ideologici che ci allontanano dalla difesa degli interessi nazionali. Devo dire che anche il precedente Governo, nella consapevolezza che questo stabilimento ha una valenza strategica che l'Italia è la seconda manifattura d'Europa e che soprattutto non si può e non si deve fermare la produzione dell'acciaio in questo Paese, ha fatto una serie di cose: la prima è l'autorizzazione a Sace a rilasciare garanzie su finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore degli impianti siderurgici. È stata destinata la cifra di 150 milioni di euro dei fondi confiscati alla precedente gestione per progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio. È stata autorizzata Invitalia a sottoscrivere aumenti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci per un valore di 705 milioni di euro. È chiaro che anche il Governo attuale deve affrontare le gravi esigenze di liquidità e l'esplosione dei costi energetici e ha il dovere di definire un piano industriale adeguato. Quel che è certo, però, è che questa vicenda non sarà risolta sul piano giudiziario e dico con franchezza a chi ha applaudito a sentenze come quelle del maggio 2021, che hanno irrogato pene esemplari alla precedente proprietà, chi se ne vanta che dovrebbe ricordare che alcune responsabilità le ha anche lo Stato, perché negli oltre sessant'anni di storia di questo complesso industriale soltanto diciassette sono stati a conduzione privata; a conduzione privata; nei restanti, Ilva era sotto il controllo pubblico e una cosa che per qualcuno in questo Paese è di per sé migliore, cioè il fatto che fosse lo Stato a occuparsene, in realtà ha visto molte lacune e criticità anche quando lo Stato ha avuto responsabilità di gestione.

sono noti e che non vogliono assolutamente dire che chi guida l'ex Ilva è autorizzato a sversare in atmosfera qualsiasi inquinante o a compiere atti illeciti. Serva da monito a chi ha un'impronta giustizialista la storia dell'ex prefetto di Milano Bruno Ferrante, per il quale i pubblici ministeri avevano chiesto una condanna a diciassette anni di carcere e che poi è stato assolto dopo un processo durato un decennio. Siamo favorevoli allo scudo penale perché siamo convinti che, se vogliamo disegnare un futuro industriale per questo Paese, occorre uscire da una logica binaria che prevede che l'industria sia sempre e comunque sinonimo di inquinamento e che la protezione dell'ambiente si possa realizzare solo e soltanto bloccando le produzioni, fermando lo sviluppo e condannando migliaia di persone alla perdita del posto di lavoro. Non è così. Pensiamo che non sia così ed è un fatto che solo in Italia acciaio e ambiente sono considerati incompatibili. Grazie alle moderne tecnologie, le due cose non solo non sono più alternative,

per una volta sono d'accordo con lui, ma questa cosa dobbiamo tenerla a mente mentre siamo costretti ad acquistare acciaio all'estero, magari anche da Paesi che non hanno i nostri vincoli ambientali e che non pagano le loro emissioni quanto le fanno le nostre aziende. alle elezioni politiche, il MoVimento 5 Stelle ottenne a Taranto il 47 per cento dei voti, promettendo che avrebbe chiuso lo stabilimento e bonificato tutto. Non è andata così, tuttavia quella battaglia un esito lo ha prodotto: sotto il Governo Conte fu infatti cancellato lo scudo penale, che era una delle architravi della gara predisposta dal Governo Gentiloni, quando ministro dello sviluppo economico era Carlo Calenda Cancellando lo scudo penale con un tratto di penna, si è consentito ad ArcelorMittal di sottrarsi ai suoi impegni - ebbene sì - e si è provocato l'ingresso dello Stato nel capitale sociale. Potevamo forse vedere dunque un altro film, con un esito diverso, ma oggi siamo di fronte ad un copione già scritto, che è frutto di quell'errore del 2019. Ne prendiamo atto. Il decreto-legge in votazione votazione è abbastanza modesto. Non sposta più di tanto i termini della questione; consente l'immissione di liquidità che era già stata prevista, con la flessibilità necessaria a far fronte all'esplosione dei costi energetici. La bolletta dell'Ilva, infatti, è passata da 200 milioni a 1,5 miliardi e questo, per un'azienda che ha un fatturato di 3,5 miliardi, evidentemente non è sostenibile. Ugualmente, sarebbe impensabile immaginare una conduzione dell'Ilva nei prossimi anni senza la reintroduzione dello scudo penale. Tutto ciò non ci entusiasma, perché la soluzione avrebbe potuto essere diversa. Tuttavia, la politica non si fa con i se e con i ma e bocciare questo decreto oggi non ci darebbe la possibilità di tornare indietro nel tempo e di evitare gli errori che sono stati commessi. Prendiamo per buone le affermazioni della Presidente del Consiglio, che ha affermato che il consolidamento della partecipazione in Acciaierie d'Italia non prelude alla stabile nazionalizzazione dell'Ilva, anche se certe previsioni di questo decreto ci lasciano molto La partita decisiva, adesso, è nell'attuazione di quel piano di sviluppo che è stato illustrato dall'azienda anche nel corso delle audizioni che si sono svolte in Commissione industria e che punta, in un decennio, alla completa decarbonizzazione della produzione. Lo diciamo francamente: non siamo ottimisti, anche perché par di capire che quel piano si fondi sul pieno utilizzo di una modalità di produzione a idrogeno ancora lontanissima dalla maturità. Ci piacerebbe poterci fidare di questo Governo e del *partner* industriale che ha al suo fianco, che in questi ultimi anni ha mostrato una certa dose di opportunismo. Nell'uno e nell'altro caso, abbiamo motivate riserve anche sul piano industriale. Tuttavia, per favorire la produzione dell'acciaio in questo Paese, per il bene dell'Italia e della sua politica industriale, sperando di essere smentiti nei dubbi che abbiamo, annunciamo un voto di astensione al provvedimento. la questione dell'acciaieria di Taranto si trascina ormai da molti, forse troppi anni. Sono ormai decine gli interventi normativi in tema di Ilva:

di un problema che si trascina da molto tempo e che il decreto-legge in esame tenta di portare a soluzione. Tra le questioni da mettere insieme, rispetto a uno dei siti industriali più inquinati e pericolosi d'Italia, vi è quella di coniugare lo sviluppo industriale con la salvaguardia dei posti di lavoro e il rispetto della salute e del lavoro. La tematica è stata affrontata nelle sedi parlamentari e in quella regionale e comunale e, per le implicazioni che comporta, ha interessato anche alcune sentenze della Corte costituzionale e persino della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il decreto si inquadra appunto all'interno di una cornice di provvedimenti assunti negli anni dall'autorità giudiziaria. Le norme puntano proprio a risolvere le questioni annesse alle problematiche ambientali, coniugandole con il rispetto massimo del diritto alla salute della comunità locale e con la tutela dell'occupazione. Il provvedimento è quindi anche il prodotto di un confronto tra il Governo, le amministrazioni e i soggetti privati coinvolti, che ha portato alla decisione di mantenere la produzione di acciaio nel rispetto dell'ambiente e della salute. Dopo il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), da parte del Ministero dell'ambiente, sono stati fissati termini per il rispetto dei tempi e delle procedure di risanamento. La società Ilva ha quindi la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti ed è autorizzata proseguire la produzione e la vendita per tutto il periodo di validità dell'AIA.

necessari. Si sono registrate critiche, ma soprattutto proposte, da parte degli auditi, che hanno portato la Commissione a migliorare e integrare il testo uscito dal Consiglio dei ministri. In particolare, vengono modificate le misure di rafforzamento patrimoniale previste nel 2019, volte ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico dell'Ilva di Taranto. Inoltre, viene specificato che gli interventi sono autorizzati anche in costanza di provvedimenti di sequestro e confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico e viene eliminato il riferimento al fatto che gli stessi debbano essere effettuati nell'anno 2022. Cambia inoltre la definizione degli strumenti d'intervento, chiarendo che Invitalia è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale sociale e a erogare finanziamenti in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato. La Commissione ha poi introdotto un comma che prevede la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali nell'area di Taranto anche per l'industria aeronautica. Con nuove disposizioni si entra sulla procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, prevedendo che questa possa avvenire su istanza del socio pubblico detentore di almeno il 30 per cento delle quote societarie. Oltre a ciò, si cambiano i criteri per la determinazione e le modalità di compenso ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato d'insolvenza. Un'altra modifica introdotta in Commissione prevede premi e penalizzazioni ulteriori per i commissari straordinari. Inoltre, una modifica pure introdotta in Commissione riferisce la previsione agli incarichi di amministratori giudiziari conferiti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. La Commissione ha introdotto anche un articolo aggiuntivo, che contiene modifiche alla disciplina del comitato di sorveglianza, con termine di tre anni per la durata del mandato e il limite al cumulo degli incarichi. quindi di norme che introducono modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, in materia di sanzione interdittiva, misure cautelari e sequestro preventivo, al fine di limitare l'applicazione alle imprese d'interesse strategico nazionale di misure che impediscono la prosecuzione della loro attività. Vengono integrate le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale con due nuovi commi, i quali specificano gli effetti del provvedimento di sequestro che abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarate d'interesse strategico nazionale. Si prevede la non punibilità della condotta dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione ai provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato d'interesse strategico nazionale. prorogata per tutto il periodo di vigenza del Piano ambiente, approvato nel 2014, l'esclusione sia della responsabilità amministrativa a carico della persona giuridica società Ilva SpA sia della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati. Insomma, si tratta di una serie di modifiche che possiamo considerare molto tecniche, ma tanto serviranno ora per provare a uscire da questo pantano e tornare a produrre in sicurezza, nel rispetto delle disposizioni che chiedono la tutela dell'ambiente. È un percorso non facile, attraverso il quale Governo e Parlamento intendono continuare a sostenere Taranto e il suo maggiore polo produttivo. Ecco perché al provvedimento va il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, nella speranza che queste norme raggiungano gli scopi prefissati. rappresentante del Governo, colleghi, a nome del MoVimento 5 Stelle esprimo da subito il nostro voto contrario al provvedimento in esame, che antepone gli interessi economici all'esigenza di tutelare i valori fondamentali dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro. È un provvedimento pericoloso, innanzi tutto perché, con il ripristino dello scudo penale, già eliminato con il Governo Conte II, si reintroduce l'autorizzazione a mettere a rischio la salute dei cittadini, in violazione del diritto alla vita e alla sicurezza sociale. Si priva infatti la magistratura, ma anche le stesse istituzioni, di quegli strumenti necessari per impedire che impianti dannosi per la salute dei cittadini e dei lavoratori possano continuare ad inquinare, sollevando gli amministratori di quelle aziende da ogni tipo di responsabilità. La norma si pone in palese contrasto con la Costituzione, in particolare con i novellati articoli cui la Repubblica tutela l'ambiente, e 41 della Costituzione, secondo cui l'attività economica non può svolgersi in modo da creare danni alla salute e all'ambiente, ma anche con le norme europee sui diritti dell'uomo e la giurisprudenza. Con questo provvedimento state perpetuando il sostegno di un antiquato e superato paradigma economico-produttivo senza prospettiva, contrario agli obiettivi europei della transizione ecologica, basato ancora su inquinamento e impunità, che provocherà ulteriori danni alla salute e all'ambiente e in alcuni casi, come per l'ex Ilva, condannando anche a morte altri cittadini. Per scongiurare la chiusura di impianti strategici come l'ex Ilva di Taranto, avete persino stabilito che gli stessi non possano essere oggetto di sequestro e di misure interdittive, perché basterà impegnarsi ad adottare un semplice e indefinito modello organizzativo idoneo a garantire uno pseudo-bilanciamento tra continuità produttiva e tutela della salute, come se il diritto fondamentale alla vita potesse essere bilanciato per garantire l'attività economica. Sull'ex Ilva di Taranto, poi, dimostrate di non conoscere la realtà e le sentenze di condanna della corte di assise del tribunale di Taranto e della Corte europea dei diritti dell'uomo: quest'ultima solo il 5 maggio 2022 ha condannato ancora una volta lo Stato italiano per non aver soprattutto tutelato la salute dei cittadini e per non avere introdotto misure predittive contro le emissioni nocive del siderurgico. Per cui vi chiedo: come è possibile, di fronte al permanere di questo disastro ambientale, peraltro ancora in corso, parlare di bilanciamento di interessi? Nel concepire questa assurda norma, per caso vi siete chiesti come realizzare il bilanciamento per tutelare il diritto alla salute? Saremo curiosi, insieme ai cittadini di Taranto, di conoscere il numero di decessi o di malattie tollerabili: avete fatto questo calcolo? Vorremmo sapere se nel computo siano inclusi anche tutti quei cittadini e quei bambini che hanno già pagato il bilanciamento con il prezzo della vita o delle malattie. Non può esistere un interesse superiore, anche se siamo di fronte a un impianto che ritenete strategico per il Paese, a quello del diritto alla vita, specialmente quando a Taranto c'è non un rischio di inquinamento, ma la certezza dell'inquinamento.

prima si scriveva che il bene della salute è assicurato all'uomo come uno e anzi come il primo dei diritti fondamentali. La stessa Suprema corte, inoltre, afferma anche che nessun organo di collettività potrebbe disporre, per qualsiasi motivo di pubblico interesse, della vita e della salute di un uomo. Vi chiediamo pertanto se la tutela ambientale e della salute è un principio che vale per tutti tranne che per quelli di Taranto e attendiamo una risposta su questo. La posizione del MoVimento 5 Stelle sul tema rimane quella di sempre: chiusura delle fonti inquinanti e riconversione economica, sociale e culturale nella prospettiva della transizione energetica ed ecologica. Per noi la vita umana è un valore da preservare a ogni costo e non può essere merce di scambio. Per assicurare il diritto di uccidere vi siete perfino spinti oltre, eliminando anche il vincolo del dissequestro degli impianti quale condizione necessaria per sbloccare i finanziamenti pubblici e garantire la continuità produttiva. In questo modo vi state assumendo una grande responsabilità: state finanziando, con altro denaro pubblico, impianti che ancora oggi continuano a inquinare, così come è stato affermato recentemente dalla corte d'assise di Taranto sul rigetto della domanda di dissequestro. Inoltre, a sostegno del vostro disegno banditesco, avete persino blindato il testo, senza permettere al Parlamento di migliorarlo e di eliminare le storture giuridiche in esso Diverse erano le proposte emendative del MoVimento 5 Stelle - caro ministro Urso, mi potrebbe anche ascoltare invece di andar via

abbiamo proposto di vincolare le ingenti risorse pubbliche, pari ad oltre due miliardi, a finanziare investimenti ecosostenibili in conformità agli obiettivi del *green deal*. Abbiamo anche chiesto tutele a favore dei nuovi poveri ossia i lavoratori ex Ilva, quasi 5.000 persone in perenne cassa integrazione, di cui 1.500 in amministrazione straordinaria in attesa di ricollocamento. Sono nostre le proposte di riconoscere indennità per il lavoro usurante, per l'esposizione all'amianto, piani di riqualificazione per il loro reinserimento anche in altre attività produttive. E questo perché Taranto non vuole più vivere solo di produzione di acciaio: attende la riconversione industriale orientata all'ecosostenibilità. Abbiamo anche chiesto e suggerito forme di tutela alle imprese dell'indotto per riconoscerle imprese strategiche in modo tale da preservare il loro diritto di credito alle prestazioni. Voglio ricordarvi che già le imprese dell'indotto hanno avuto una perdita di oltre 100 milioni per l'amministrazione straordinaria nel 2015. Abbiamo altresì suggerito forme di tutele sanitarie e ambientali con le proposte di legge volte a introdurre la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario e la revisione dei limiti degli inquinanti, di cui al decreto legislativo n. 155 del 2010, considerati troppo elevati dall'OMS. Abbiamo infine proposto un accordo di programma per favorire il reinserimento dei lavoratori, salvaguardare le imprese dell'indotto, riqualificare l'ambiente, garantire la riconversione economica, sociale e culturale del territorio. Nulla di tutto questo è stato accolto. Siete stati sordi alle istanze di cambiamento del territorio. Anzi, avete avuto il coraggio, dopo due anni di immobilismo assoluto del ministro Giorgetti, nell'ultimo incontro con le parti sociali, con il ministro Urso, di paventare la possibilità di un piano industriale che prevedesse la produzione a carbone ancora per altri dieci anni, l'aumento di volumi produttivi sino a 6 milioni di tonnellate, la costruzione di un rigassificatore, la costruzione di forni elettrici

sono stati eseguiti esperimenti di combustione di materiale plastico negli altiforni, come se gli impianti fossero degli inceneritori, senza alcun preavviso alla cittadinanza. È questa la riconversione *green* che il Governo intende perseguire? Ma non era Giorgia Meloni che, in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite a Sharm el Sheikh, si era impegnata a ridurre le emissioni? O era una sua controfigura? In definitiva, Presidente, state arrestando quel processo di riconversione economico-sociale e culturale, iniziato nel corso del Governo Conte 2 con il cantiere Taranto, con il rischio che esploda una bomba sociale, economica e ambientale nel territorio di Taranto. Concludo, Presidente. I cittadini di Taranto sono stanchi, ma stanchi stanchi, di mangiare solo pane e veleno, anzi, negli ultimi anni solo veleno. *(Applausi)*.

potrebbe mettere a repentaglio il funzionamento ordinario di produzioni industriali considerate di interesse strategico nazionale. Per tale motivo risulta urgente intervenire, sia per salvaguardare determinati contesti industriali di rilievo strategico nazionale, sia per fornire allo Stato strumenti più rapidi per intervenire laddove la gestione di tali imprese dovesse ritenersi disfunzionale rispetto all'interesse nazionale, specialmente in una fase in cui il contesto internazionale richiede particolare rapidità al fine di consentire la permanenza e la competitività nel mercato. Risulta tuttavia però evidente che, se oggi c'è una crisi, questa non dipende soltanto dal caro energia. Andrebbe anche ricordato come il piano industriale del 2017 non ha mai praticamente visto la sua attuazione. Solo poco più di due anni fa il Paese viveva un disagio socio-economico crescente dovuto all'incertezza politica e all'atteggiamento troppo attendista degli Esecutivi precedenti, che hanno puntato sulla tecnica del rinvio, lasciando che i nodi si aggrovigliassero fino a diventare quasi del tutto inestricabili; un Esecutivo che pensava solo a trattare in modo serrato con l'Europa per ottenere un po' di mancette. Ma si sa che le aziende che sono sull'orlo del fallimento e rischiano di finire nella spirale dell'usura o di diventare preda dei circuiti malavitosi non hanno il tempo di attendere le decisioni europee. Si aspettano invece con ansia dal Governo scelte coraggiose e immediate, cosa a cui questo Esecutivo sta finalmente pensando. L'Italia in questi mesi ha dimostrato di saper crescere, di saper affrontare l'inflazione e di avere imprese e più in generale attività produttive capaci non solo di resistere agli urti, ma anche di fare molto meglio degli altri. A chi conviene che l'Italia viva dei momenti di ambasce? Basterebbe tirar giù un elenco di tutte le aziende italiane che negli ultimi anni hanno cambiato bandiera e proprietà e contemporaneamente osservare chi ha comprato quelle aziende e da quali nazioni. A quel punto la risposta risulterebbe molto semplice. Oggi l'Italia e soprattutto la sua impresa sta invece dimostrando di sapere molto bene il fatto suo; la crescita registrata negli ultimi mesi ne è una delle tante testimonianze. La sensazione è che la forza delle imprese italiane possa creare un certo disagio alle nostre opposizioni, quasi come se l'obiettivo della crescita del Paese non fosse comune, ma valido, eventualmente, solo se a governare è la sinistra. Con il provvedimento in esame si vuole lavorare perché Acciaierie d'Italia SpA (ex Ilva) torni a essere la più grande fabbrica siderurgica d'Europa. *(Applausi).* I due eventi straordinari I due eventi straordinari degli ultimi anni (la pandemia e il conflitto russo-ucraino) hanno causato effetti *shock* sia sulla produzione che sui prezzi. Nella fattispecie, a seguito degli aumenti di prezzo, il costo dell'energia - come già ricordato da altri colleghi è passato per l'azienda da 200 milioni circa in un anno normale (come il 2019) a un miliardo e 550 milioni in termini finanziari, che, compensati con il meccanismo del *tax credit*, sono diventati 1.100 miliardi; si tratta comunque di un onere insostenibile, abbastanza

per proseguire l'attività e garantire il risanamento ambientale. Nel 2017 il ministro dello sviluppo Calenda diede il via libera all'offerta ArcelorMittal, scartando quella della cordata Arvedi-Jindal. Furono sufficienti neanche due anni per accertare l'indisponibilità indiana a farsi carico delle incombenze che il Governo Conte accollò a Invitalia, all'epoca di Domenico Arcuri. Secondo il punto di vista di una sinistra ormai fin troppo franata in considerazioni che sanno veramente di vecchio, quando c'è una crisi lo Stato deve fare economia. Noi viaggiamo su tutt'altra lunghezza d'onda: quando c'è una crisi, lo Stato ha il dovere di mettere in condizione le imprese di fare economia. Il contrario non può mai valere: sarebbe una visione folle, che ci riporta a un'ideologia del secolo scorso che è morta fortunatamente con la caduta del muro di Berlino. I 680 milioni deliberati dal Governo all'ex Ilva serviranno a riprendere fiato e ad alleggerire l'enorme indebitamento che la schiaccia: parliamo di 600-700 milioni di debiti solo nei confronti di Eni e Snam per le forniture di gas e di altri 100 milioni da corrispondere all'indotto di Taranto. Alla luce di ciò condividiamo certamente il rafforzamento patrimoniale di AdI. Tuttavia, siamo consapevoli che non vi potrà essere crescita duratura, se questo non viene ancorato a un piano industriale di rilancio che miri a restituire una prospettiva di sviluppo alle imprese dell'indotto e, di conseguenza, all'intero territorio. Cari colleghi, stupisce poi che, dopo un silenzio durato anni e dopo che persino in campagna elettorale il PD non ha detto una parola - dico una - sull'ex Ilva, il *dossier* industriale più importante del Paese, oggi ci troviamo con un'opposizione che tuona contro il Governo e con un decreto che finalmente - aggiungo - pone tutte le condizioni affinché l'azienda possa tornare a produrre e, quindi, a guadagnare, mantenendo l'occupazione. Sarà forse complice la campagna per le primarie congressuali, ma persino i due candidati segretari del Partito Democratico sono diventati improvvisamente esperti siderurgici. Così, dopo mesi di silenzio sulla vertenza, entrambi si stanno improvvisando in grosse dichiarazioni sull'acciaio, partendo ovviamente dal loro pallino, vale a dire dal cambio della *governance* *governance* e, non per un efficientamento delle strutture, ma per una mera occupazione di potere. La proposta di Bonaccini prevedeva come grande novità i forni elettrici. Forse gli è sfuggito che il piano per aggiungere un forno elettrico e un impianto DRI già esiste ed è stato finanziato dal Governo Meloni nel decreto aiuti, mentre Emiliano e sindaco di Taranto che sostengono Bonaccini chiedono la chiusura dell'area a caldo e, quindi, di tutta la fabbrica: dunque l'esatto opposto di quanto dichiarato dal candidato segretario. In altre parole, mentre loro litigano, noi pensiamo ai fatti e al bene del Paese. Per anni poi, rispetto alla questione ex Ilva, abbiamo dovuto subire un'ideologia perbenista e fintamente al servizio dell'uomo, che non fa nient'altro che tendere ad alimentare l'antinomia tra la protezione dell'ecosistema e lo sviluppo della proprietà industriale. Per fortuna, però, a volte la magistratura smonta questi teoremi e ristabilisce un corretto ordine delle cose, dimostrando che si può produrre in sicurezza, evitando devastazioni ambientali e proteggendo la salute delle comunità senza alimentare contrapposizioni di natura ideologica. Questo ragionamento è particolarmente valido per quello che si può definire la telenovela infinita dell'IVA. Quanto ai colleghi del MoVimento 5 Stelle - prima sentivo le accuse mosse al Governo - hanno sempre detto che non volevano quel mostro d'acciaio in Puglia, offrendo come alternativa per gli oltre 10.000 dipendenti gli allevamenti di cozze pelose, come detto da personaggi del Governo dei 5 Stelle. Se all'opposizione dà fastidio la tutela dell'interesse nazionale e dell'Italia, se ne facciano una ragione, perché questo invece è il nostro unico obiettivo: vale a dire evitare la paralisi delle aziende di interesse strategico nazionale e su questo infatti lavoriamo alacremente. In tale prospettiva, il decreto-legge nella seconda parte inserisce due nuovi commi all'articolo 104-*bis* in materia di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari, nonché in materia di tutela dei terzi nel relativo giudizio. Nella stessa logica si è introdotta una disciplina processuale volta a valorizzare non soltanto la posizione dell'indagato o del soggetto che avrebbe diritto alla restituzione del bene, ma anche l'interesse dello Stato alla continuità dell'attività tramite la legittimazione processuale dei soggetti preposti alla tutela dell'interesse strategico nazionale dello stabilimento e alla tutela dell'ambiente. L'articolo 7 prevede poi la non punibilità della condotta dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale.

È evidente al contempo che, sia per le aziende di interesse strategico dell'Italia, sia per tutta la vicenda legata all'ex Ilva, niente è destinato a concludersi con l'approvazione del decreto-legge in esame. Ci auguriamo, tuttavia, di restituire alle aziende la solidità necessaria per raggiungere la ripresa produttiva, che è una priorità da perseguire, anche a sostegno di tutto l'indotto. Nessuno deve dimenticare in quest'Aula che l'ex Ilva rappresenta un *asset* produttivo di primaria importanza per il Paese ed è semplicemente folle anche solo pensare che possa essere andato perso. Sappiamo che in quest'Aula c'è ancora qualcuno che si commuove alla retorica comunista. Tutta la storia dell'industria moderna mostra che il capitale lavora senza scrupoli per far precipitare tutta la classe operaia al livello della più profonda degradazione: questa frase di Karl Marx fa emozionare addirittura qualcuno in quest'Aula. «La difficoltà non risiede nelle idee nuove, ma nello sfuggire a quelle vecchie»: così diceva Keynes, uno dei più influenti economisti del XX secolo. Si riferiva a questo genere di idee, ma sfuggiremo alla visione di un'economia sempre e solamente socialista. D'altronde, come riteneva sempre Keynes: «Il socialismo marxista deve

Presidente, noi dobbiamo correre, perché chi c'era prima di noi ha perso troppo tempo. Corriamo perché il mercato globale non aspetta le contorsioni della politica. Corriamo perché l'Italia non può rinunciare alla propria vocazione industriale e tecnologica. tecnologica. Sappiamo che questo è il destino dell'attuale Esecutivo sui principali *dossier* che riguardano l'industria italiana, ma accettiamo l'onere con estremo orgoglio. Corriamo, intanto andiamo avanti, certi di avere una sola preoccupazione, ossia la tutela degli interessi degli italiani e nient'altro. Per questo votiamo in modo favorevole, come Gruppo Lega Salvini Premier, su questo decreto-legge.

la vicenda dell'ex Ilva si trascina di fatto da ormai oltre undici anni e ha assunto le dimensioni di una enorme matassa di fronte alla quale tutta la classe dirigente del Paese, istituzionale e politica, nazionale e locale, economica e sindacale, è chiamata ad assumersi piene e precise responsabilità. La gravissima situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda è ormai tale che a essere sempre più in forse è la stessa continuità produttiva del più grande polo siderurgico d'Europa. Questo è il punto, né più né meno. Il problema è che, di fronte a questa disastrosa prospettiva, ci troviamo a discutere di un provvedimento che è del tutto inadeguato, incapace com'è di incidere sulla realtà e e di centrare alcuno degli obiettivi necessari. Questo perché non muove dalla comprensione di una realtà, quella di Taranto, che da anni vive una situazione drammatica e sta rischiando di sprofondare in una crisi occupazionale e sociale gravissima; inoltre, perché è privo di una strategia nazionale per il nostro Paese che, se vuole continuare a essere competitivo dal punto di vista economico, ha bisogno di una vera e rinnovata politica industriale dotata di una visione. Ma in questo decreto-legge, francamente, di visione non c'è traccia. D'altra parte, non è una novità. Poche settimane fa abbiamo affrontato il decreto Lukoil e anche in quella circostanza abbiamo visto affermarsi una logica da pronto soccorso, senza la capacità di proporre una terapia adeguata, proprio come oggi rispetto al provvedimento Si sta giocando la più importante partita di politica industriale per l'Italia con visione zero e in totale assenza di un piano nazionale della siderurgia. in tutta la discussione, non è venuta una parola su come si intende affrontare la difficile situazione del mercato dell'acciaio, sia per quanto riguarda la produzione, sia per quanto riguarda i prezzi. Inoltre il Governo, durante tutta la fase di discussione, ha dimostrato di essere completamente sordo alle istanze e alle voci che sono giunte dalle istituzioni locali e dal territorio e che abbiamo ascoltato nel corso di tutte le audizioni. *(Applausi)*. Questo è un decreto-legge miope, di cortissimo respiro, che si limita a stanziare risorse per cercare di far fronte alla situazione debitoria pregressa, con il rischio però - colleghe e colleghi - di di bruciarne altre di risorse, anche per via di una gestione piuttosto discutibile, quando invece sarebbe necessario un piano di investimenti calibrato sulle politiche ambientali e industriali per il sito. È la ragione per cui abbiamo chiesto, con i nostri emendamenti, un programma pluriennale per vincolare le misure di rafforzamento patrimoniale; un tavolo istituzionale composto dalle amministrazioni centrali e locali aperto al territorio, alle organizzazioni sindacali e ai rappresentanti degli operatori economici e delle imprese. Era questo il modo per dare un riconoscimento pubblico e legislativo a Taranto, una realtà che ha già pagato un tributo altissimo, e arrivare finalmente a una vera e propria svolta per realizzare gli obiettivi fondamentali: bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica, tutela della salute, salvaguardia dei livelli occupazionali e formazione dei lavoratori per prepararli ai nuovi processi produttivi. Mi rendo conto c'è qualcosa di molto diverso in questo decreto e non c'è quello che sarebbe stato necessario: un piano industriale ambizioso, che avrebbe richiesto ben altra attenzione e programmazione da parte del Governo. Infatti, in una situazione in cui ci sono 3 milioni milioni di tonnellate di acciaio prodotti e 7.000 addetti in cassa integrazione, è evidente che questo diventa un tema cruciale e il Governo avrebbe dovuto affrontarlo in modo diverso. E ciò anche perché non sfugge a nessuno, certamente non sfugge a noi che, mentre Taranto rallenta fino a quasi fermarsi, condizionando anche gli altri siti presenti in Italia, ArcelorMittal corre in altri stabilimenti e nel resto d'Europa. È evidente, quindi, che qualcosa, anzi molto non torna e non funziona. Ma è il motivo per cui, a fronte di nuove risorse pubbliche,

maggioritaria al socio pubblico, anticipandolo al 31 dicembre 2023. Voglio dire con molta chiarezza - anche questo è stato detto nel corso di tutte le audizioni - che, senza un assetto diverso, senza una nuova *governance* e una guida capace e sicura, non si riuscirà ad affrontare il tornante decisivo che abbiamo davanti. È vero che dal punto di vista ambientale non c'è paragone rispetto a dieci anni fa, ma questo non può bastare. E quel che si è fatto non è sufficiente: troppo grande e cruciale è la sfida ambientale per non vedere che l'indispensabile piano di decarbonizzazione da portare avanti non può essere solo uno *slogan*, ma deve essere anche un preciso obiettivo per arrivare alla completa eliminazione delle emissioni climalteranti. E la produzione di acciaio *green* di cui tanto si parla non è solo possibile, ma è la carta su cui Taranto deve puntare per tornare a essere competitiva. Allo stesso modo, non si può non tenere costantemente presente che l'ex Ilva è anche l'indotto: di questo ci siamo occupati, cercando di tutelare le imprese fornitrici, consapevoli che il livello di sofferenza del contesto industriale che gravita gravita attorno ad Acciaierie d'Italia è arrivato ormai a un punto limite. Per questo è indispensabile ripartire con gli ordini e le attività delle imprese appaltatrici dell'indotto devono ripartire. È per questo che abbiamo previsto di stanziare 50 milioni di euro per le fatture non saldate e garantire l'accesso al credito per i fornitori creditori di Acciaierie d'Italia. Come se tutto questo non bastasse non bastasse ancora, a sconcertare di più è la totale assenza di attenzione da parte del Governo ai temi dell'ambiente e della salute dei cittadini. Da parte nostra abbiamo chiesto che si effettui la valutazione di impatto sanitario, prevedendo, in caso di rischi per l'ambiente, il riesame degli atti autorizzativi per la prosecuzione di attività produttive.

applicabilità per fatti riguardanti la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Per tutto questo serve un cronoprogramma degli investimenti, perché elettrificazione e decarbonizzazione sono le strade che possono consentire a Taranto di ritornare centrale nella produzione di acciaio in Europa. Tutto questo manca nel decreto-legge, perché non nasce da uno sguardo portato avanti e lontano. Colleghi, i piani Mattei che tanto vengono evocati parlando di immigrazione dovrebbero servire innanzitutto a fare delle politiche industriali nazionali, cosa che non troviamo né in questo né nei decreti-legge precedenti. Per fare tutto questo ci vorrebbe una visione. Del resto, è dall'inizio di questo cammino che il Governo procede così a tentoni, alternando operazioni di cinico e rozzo *marketing* politico, portate avanti su un piano identitario e ideologico, a provvedimenti improvvisati e confusi come questo; provvedimenti sui quali il più delle volte ha dovuto fare imbarazzate retromarce, fino al presente decreto-legge e per stare all'attualità - alla vicenda di queste ore del superbonus e della cessione dei crediti fiscali, su cui ci si è mossi senza alcun preavviso, senza un progetto chiaro, mettendo in pericolo la sopravvivenza di 25.000 aziende e rischiando di provocare un vero e proprio terremoto sociale. sociale. A guidare ogni passo del Governo sembrano esserci davvero due parole: improvvisazione e approssimazione. Come principale forza dell'opposizione, se anche noi pensassimo solo al nostro esclusivo interesse, dovremmo esserne lieti, perché con il passare del tempo e il moltiplicarsi di provvedimenti che creano problemi o addirittura dannosi, gli italiani che hanno dato fiducia a questa maggioranza si accorgeranno di averla malriposta. però siamo abituati a fare diversamente, a ragionare pensando al bene del Paese e, se oggi esprimiamo critiche approfondite e molto argomentate, teniamo a questo Paese. Con il decreto-legge in esame non si raggiungono gli obiettivi che si dovrebbero ottenere e lo giudichiamo insufficiente, incapace di affrontare una partita decisiva per un settore fondamentale della nostra industria. E questa insufficienza e questa incapacità davvero non possiamo permetterle. Per questo il Partito Democratico esprimerà un voto contrario. Signor presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, rappresentanti del Governo, sono contenta di poter intervenire in dichiarazione di voto su un provvedimento così importante che riguarda la terra che amo: la mia Puglia, la nostra Puglia. Sono altresì felice di poter soddisfare qualcuno che, come da tradizione del partito al quale appartiene - la solita sinistra demagogica e populista - aveva così forte la necessità di sentire la mia voce. È giusto, senatrice Aurora Floridia? In quest'Aula negli ultimi dieci anni si è discusso e soprattutto taciuto - ahimè - su svariati decreti-legge

casi sì che c'erano elementi errati assurdi, e non in un testo come questo che ha necessitato solo di alcune piccolissime limature tecniche. Il decreto-legge che ci accingiamo a convertire punta all'efficientamento di settori strategici per il nostro interesse nazionale, perché è rivolto a quelle realtà in grado di incidere positivamente sul PIL italiano che dunque creano ricchezza economica e benessere. Il provvedimento è stato elaborato dal Governo mentre era all'esame del Parlamento il decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici; una circostanza che scandisce in tutta evidenza la prontezza, l'operatività e la serietà con cui il Governo si pone rispetto ai problemi atavici e alle grandi questioni che investono il Paese. Infatti, durante l'esame del precedente decreto era emersa l'esigenza di intervenire per consentire la prosecuzione dell'attività produttiva in particolari circostanze, con riferimento allo stabilimento di Priolo. Oggi ci troviamo di fronte al decreto-legge n. 2 del 2023, che non soltanto affronta i problemi urgenti del polo siderurgico di Taranto, ma permette anche di dare risposte ad altre crisi aziendali riferite ad impianti nazionali strategici. Da pugliese, da donna che da sempre fa politica sul territorio, prima ancora che da senatore della Repubblica, non posso che soffermarmi su quanto questo provvedimento entri finalmente nel merito della questione ex Ilva. Finalmente, sì, perché nel corso degli ultimi anni si sono susseguiti decreti a decreti, promesse a promesse, impegni presi con i cittadini tarantini e con quelli dell'intera Puglia da parte del Governo a maggioranza MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico senza che però nulla fosse realmente fatto in concreto. Questo decreto, invece, e non solo per il caso dell'ex gruppo Ilva, ma per tutte le imprese di interesse strategico, vuole reintrodurre le condizioni per la sostenibilità dell'investimento, stabilendo che le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità continuità dell'attività svolta. Questa è l'unica scelta di buon senso se davvero si vogliono porre in essere fatti concreti, in grado di traghettare la nazione verso una seria e credibile ripresa economica. È il momento di accantonare le chiacchiere - e troppe ce ne sono state nel corso dell'ultima legislatura - per passare ad azioni mirate, in grado di apportare un contributo fattivo e determinante per il rilancio, non solo dell'economia, ma anche del Per quanto riguarda gli effetti che il decreto ha su Acciaierie d'Italia, il provvedimento dà la possibilità che vengano attuati e definiti gli accordi tra Invitalia e ArcelorMittal, sancendo la possibilità di una modifica dei patti parasociali, che incideranno su aspetti cruciali quali la partecipazione azionaria e la futura *governance*. Ancora, oltre a tutto questo, l'intervento del Governo di centrodestra dà corpo a una serie di impegni sottoscritti dai soci: rilancio del sito produttivo; garanzie occupazionali, fissando un *target* di produzione superiore a quelli conseguiti da Acciaierie d'Italia nell'ultimo biennio; riconversione industriale per un impianto risanamento ambientale con il completamento dell'AIA nei tempi previsti; investimenti legati allo sviluppo industriale e al polo di Taranto; iniziative di economia circolare; attivazioni di impianti di desalinizzazione tramite il recupero delle acque dolci dei fiumi Tara e Sinni; lo sviluppo del porto tramite impianto di degassificazione. azioni concrete, che segnano un netto cambio di passo rispetto a quanto hanno invece fatto i Governi di sinistra, i quali, per quanto riguarda in particolare la questione dell'ex Ilva, sono rimasti schiacciati da un falso ambientalismo dall'impronta tutta ideologica, che, oltre a non determinare alcun aiuto in termini economici, non ha contribuito in alcun modo, neanche sulla sostenibilità ambientale dell'acciaieria. Il tutto senza contare i danni arrecati a uno degli *asset* fondamentali del sistema Paese e il dramma occupazionale che ha investito Taranto, la sua Provincia e l'intera Regione Puglia. Questo decreto guarda invece ad aspetti concreti, cui si vuole rispondere con azioni necessarie a far sì che possa prendere corpo una strategia e che sul tavolo non rimangano, come troppo spesso accaduto in questi anni, soprattutto per il caso ex Ilva, solo delle buone intenzioni. Chi governa e chi legifera deve avere non solo delle buone intenzioni, delle buone idee, e soprattutto il coraggio di trasformare in azioni ciò che promette agli elettori, e deve possedere le capacità di tradurre le parole in fatti tangibili. Tutti ricorderanno - anche i non addetti ai lavori - che da Monti, quindi nel 2012, a Draghi, il Governo che ha preceduto l'Esecutivo Meloni, non c'è stato Esecutivo negli ultimi dieci anni che non si sia occupato dell'Ilva di Taranto, la più grande acciaieria europea, nata nel 1965, proprio per dare ricchezza a un territorio e a tutto il Mezzogiorno. Il quarto centro siderurgico di Taranto, che fu inaugurato dall'allora presidente della Repubblica Saragat, dopo soli cinque anni dalla sua attivazione, sfornava, già nel 1970, il 41 per cento produzione totale di Italsider; percentuale che nel 1980, anno in cui lo stabilimento ricevette nuovamente la visita dell'allora presidente della Repubblica Sandro Pertini, raggiunse addirittura il 79 per cento Nel 2005 sono 188 le imprese pugliesi dell'indotto Ilva che fatturavano in totale 310 milioni di euro. Taranto, la Puglia e il Mezzogiorno rappresentavano un'eccellenza dell'industria, il motore dell'economia italiana. Meno di vent'anni dopo, alla luce di una gestione ottusa e populista, qualcuno è riuscito a cambiare in peggio la storia economica del nostro Paese. Purtroppo, l'attenzione del Governo italiano si è resa necessaria dal sequestro degli impianti nel luglio 2012 per gravi reati ambientali ed è via via proseguita con una serie di decreti-legge chiamati a dare risposta alle emergenze che di volta in volta si presentavano. Questo certamente ha generato un danno economico, ma la tragedia umana che hanno vissuto i cittadini di Taranto è più di tutto lo stimolo a fare presto e a risolvere definitivamente il problema ambientale. La prima cosa da fare, su un problema così complesso come quello dell'Ilva, è mettere da parte demagogia e populismo e affrontare il tema in chiave di politica industriale. Per questo, più avanti elencherò quello che di buono - molto poco, in realtà - è stato finora fatto, oltretutto in modo decisamente intempestivo. infatti, in questi anni dove ci ha portato una simile conduzione del problema. I 5 Stelle hanno illuso e massacrato un territorio, senza dare alcun apporto oggettivo alla risoluzione del problema. Nessun risultato è stato raggiunto, nessuna promessa si è trasformata in realtà; semmai, la questione si è complicata ulteriormente. È chiaro che Acciaierie d'Italia è un valore aggiunto per il Mezzogiorno tutto, e che Taranto e la Puglia non possono fare a meno di una presenza industriale così importante. Dentro e fuori dai confini nazionali l'acciaio alimenta catene e filiere dell'economia nazionale, ma i pugliesi non possono continuare a pagare il costo economico e sociale della mancata sostenibilità ambientale dell'impianto. Ora che lo Stato è parte di Acciaierie d'Italia l'attenzione deve fortemente concentrarsi sulla soluzione, sugli incentivi e gli aiuti concreti. Per questo discutiamo oggi di questo decreto-legge perché, con il Governo Meloni, lo Stato fa lo Stato e non si nasconde dietro a demagogia e populismo. Il Governo fa il Governo e non una sterile e perpetua propaganda politica. La maggioranza fa la maggioranza e lavora per gli interessi della Nazione e per gli italiani. Le priorità sono la sostenibilità ambientale, la sicurezza, la competitività dell'impresa, a maggior ragione visto il nuovo scenario energetico internazionale. È sulla scorta di queste

vadano assolutamente nella direzione giusta, nonché nella consapevolezza che questo Governo ha tutte le carte in regola per riuscire a determinare le migliori condizioni economico-sociali e che la nostra Nazione, come è sempre stata, è una grande Nazione, annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia *(Applausi)*, perché dal voto di oggi in quest'Aula sono certa che si potrà iniziare a scrivere un nuovo capitolo in grado di proiettare l'ex Ilva, la città di Taranto, la Regione Puglia e l'intera Italia nel futuro.

Presidente, la ringrazio e mi scuso per aver raggiunto l'Aula in ritardo, ma questo è avvenuto per una ragione indipendente dalla mia volontà. la Commissione affari costituzionali, ha dovuto interrompere i lavori allo allo scoccare delle 15,30, senza aver nemmeno potuto iniziare a esaminare e votare i singoli emendamenti. Quindi la prima osservazione che mi corre l'obbligo di fare, dato che stiamo discutendo di una questione pregiudiziale avanzata dal Gruppo Partito Democratico e da altri Gruppi ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del Regolamento, è che uno dei motivi per cui sarebbe bene non proseguire l'esame di questo provvedimento è che si tratta di un provvedimento molto importante, contenente a nostro avviso disposizioni molto gravi e rilevanti, che il Senato della Repubblica non ha avuto tempo a sufficienza per esaminare. La nostra Commissione si è potuta occupare di questo provvedimento, che ha effetti così rilevanti, per pochissime ore. C'è una ragione per cui questo è avvenuto? A noi sfugge. Il decreto-legge n. 1 del 2023 è stato promulgato il 2 gennaio del presente anno, è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* in pari data ed è entrato in vigore il 3 gennaio 2023. Questo significa che il Senato poteva utilizzare questa settimana per tutti gli approfondimenti necessari e opportuni, in quanto avrebbe potuto benissimo passare alla votazione degli emendamenti e al voto finale sul provvedimento la prossima Per quale ragione la Conferenza dei Capigruppo abbia assunto una determinazione diversa, ledendo le prerogative di tutta la 1a Commissione e in particolare dei Gruppi di opposizione, che non hanno potuto nemmeno iniziare a votare i loro emendamenti uno per uno, noi lo ignoriamo e non possiamo, in sede di discussione della questione pregiudiziale, non sottolinearlo. Quindi il primo motivo per cui, a nostro avviso, non bisognerebbe continuare ad esaminare questo provvedimento è che non si può affrontare, con questa leggerezza, con questa fretta e con questa mancanza di spiegazioni sulla fretta, un provvedimento di tale importanza. Poi è un provvedimento ingannevole, tragicamente ingannevole. Il titolo di questo decreto è: «Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori». Ma non si ravvisa, all'interno del provvedimento, niente che assomigli a una volontà di gestione dei flussi migratori. Il titolo del decreto avrebbe dovuto essere: «Misure non urgenti per la strumentalizzazione politica dei flussi migratori». Questo sarebbe stato il titolo corretto e appropriato. *(Applausi)*. Quindi anche la natura ingannevole del provvedimento ci spinge a dire che non dovremmo La gestione manca, la confusione c'è tutta; è una norma manifesto, una norma propaganda. I primi a sapere che non produrrà nessuno degli effetti voluti da chi l'ha proposta sono coloro che l'hanno elaborata. Vengono dichiarati degli obiettivi, che possono essere più o meno condivisibili - e per noi non lo sono - ma gli strumenti approntati all'interno della norma per raggiungere quegli obiettivi sono palesemente inadeguati. Ci sono poi altre ragioni e ne cito due, perché il tempo corre velocemente. Si tratta di una norma che va in palese contrasto con alcune disposizioni fondamentali della nostra Costituzione e, quel che è più importante, con norme consolidate che fanno parte di convenzioni e trattati internazionali. Abbiamo ricevuto tirate di orecchi, rimproveri e critiche molto forti da organizzazioni internazionali importanti - penso, per esempio, alla commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, un'organizzazione che comprende 46 Paesi

Soprattutto, c'è una disattenzione e un'indifferenza ad alcuni diritti umani fondamentali. Quando si fa una norma di questo tipo, al di là dell'opinione politica che si ha, ci si dovrebbe porre una domanda: con queste norme si aumenta o si diminuisce la sofferenza che si infligge a persone che già molto soffrono per persecuzioni, per guerre, per fame, per tutte le ragioni che le inducono ad abbandonare la loro terra e ad affrontare un viaggio a rischio della vita in mare aperto per un sogno di vita migliore altrove? Con queste norme la sofferenza potenziale che si infligge cresce e già questo le rende irragionevoli e in contrasto con il diritto internazionale. Da questo punto di vista noi potremmo citare

«Sappiatelo, è tutto inutile. Per quanti sforzi facciate, ci sarà sempre la Costituzione sopra di voi». Lo ricordo oggi ai colleghi della maggioranza e al rappresentante del Governo; potrei anche dirvi: sappiatelo, è tutto inutile. Per quanti sforzi facciate di complicare la vita a chi va in mare per salvare vite che sono in pericolo, ci sarà sempre la Costituzione sopra di voi.

le prove di un giudizio di un qualunque tribunale italiano, sono coloro che le norme le hanno scritte. C'è totale indifferenza rispetto al fatto di scrivere norme che si sa in principio che saranno dichiarate illegittime rispetto alla nostra Costituzione e al nostro ordinamento. Come volevasi dimostrare, pochi giorni fa il tribunale di Catania

il risultato politico, quello cioè di aver indicato all'opinione pubblica un bersaglio ideologico contro cui scatenare una guerra, sarà stato raggiunto.

raddoppiare gli sbarchi nel nostro Paese; anzi, se restringiamo il periodo della valutazione dal 1° gennaio al 20 febbraio 2023,

alcuni dei partiti che oggi sono in maggioranza: avremmo avuto proteste sotto i palazzi delle istituzioni e alte grida. Oggi, invece, tutti zitti: il problema sembra sparito dall'orizzonte della discussione pubblica. Servirebbe ben altro: servirebbero intese a livello europeo; servirebbero scelte condivise. Ma rispetto a tutto ciò state facendo l'esperienza che fanno tutti i sovranisti di tutto il mondo. Anche il Governo più tostamente sovranista incontra sempre un Governo più sovranista di esso che lo spiazza, e questo sta succedendo anche a voi.

non solo perché, ancora una volta, viene scelta la strada della decretazione d'urgenza su un tema che avrebbe dovuto essere contenuto in un disegno di legge ordinario. Non è vero che esso contiene disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, ma c'è soltanto il tentativo, che dal mio punto di vista è vergognoso, di rendere più complicate e meno efficaci le operazioni di soccorso. Inoltre, proprio per il suo configurarsi come un incentivo all'omissione di soccorso, si configura come un decreto costitutivamente e intrinsecamente anticostituzionale, che contrasta tutti gli obblighi di soccorso contenuti nelle leggi. Ancora una volta avete scelto di dar vita ad una vera e propria norma bandiera, una norma ideologica, cinica, che ha un obiettivo chiaro anche se non dichiarato, cioè rendere più difficili, se non impraticabili, i soccorsi in mare. Voi partite, come spesso avete fatto in questi anni, da un assunto che però è falso, una bugia che avete alimentato con continue operazioni di propaganda, quella tesi secondo la quale le ONG che operano nel Mediterraneo centrale e che svolgono salvataggio in mare sarebbero funzionali all'immigrazione clandestina. Questa è una bugia, una tesi mai dimostrata da nessun tribunale e smentita anche da un recente rapporto delle Nazioni Unite, che certifica peraltro come le cause della migrazione degli esseri umani siano da ricercare certamente non in questo fattore, le ONG, ma nelle cause che tutti conosciamo benissimo da anni, come le guerre innanzitutto e, da un po' di anni a questa parte, anche nelle conseguenze catastrofiche dei cambiamenti climatici. Quello stesso cambiamento climatico - lo dico al Governo e alle forze di maggioranza - che avete negato per decenni, riempendovi la bocca di quella ipocrita formula che dice di "aiutarli a casa loro", mentre tutte le vostre politiche andavano in una direzione opposta, come come avete fatto anche nell'ultima legge di bilancio quando avete tagliato i fondi per la cooperazione internazionale. Differentemente da quello che voi affermate, nessun rapporto illecito è emerso tra le ONG e i trafficanti: è ampiamente dimostrato come non sia la presenza delle navi delle ONG nel Mediterraneo a determinare le partenze dalla Libia. Allora, anziché supportare le ONG, che peraltro solo lo scorso anno hanno salvato la vita a 14.000 naufraghi e a oltre 200.000 nel corso dell'ultimo decennio, voi le criminalizzate. Con questo decreto varate disposizioni che non faranno ovviamente cessare i gravi motivi che inducono le persone a fuggire, né le operazioni di soccorso umanitario imposte dal diritto internazionale. Le uniche disposizioni di urgenza che questo Parlamento dovrebbe affrontare dovrebbero riguardare non la limitazione della presenza delle ONG in mare, ma una riforma - quella sì urgente e necessaria - del sistema di accesso e accoglienza, che ponga finalmente al centro il rispetto dei diritti umani e la tutela della vita delle persone. criminalizzate le ONG, chiamate dispregiativamente sistematico il loro lavoro di ricerca e soccorso, che peraltro è sistematico perché diventa sistematico, perché nel Mediterraneo centrale

liberare quell'area dalla loro presenza, volete che non ci sia più nessuno che svolga questa preziosissima funzione. Anche il Consiglio d'Europa vi ha detto che il testo che state proponendo non è conforme agli obblighi in materia di diritti umani e neanche agli obblighi di diritto internazionale che il nostro Paese ha contratto. L'idea di mandare una nave in un luogo lontano centinaia di chilometri non è conforme né all'idea di porto sicuro, né naturalmente all'etica e all'etica e alla dignità che un Parlamento e un Governo dovrebbero avere. Allo stesso modo, i trattati internazionali non prevedono il bisogno di raggiungere tempestivamente un porto, ma solo quello di prestare soccorso. Voi volete impedire l'approdo in Italia delle persone salvate dai naufragi e, conseguentemente, impedire che l'Italia diventi lo Stato competente all'esame delle domande di protezione internazionale. Infatti, non a caso, pretendete, in uno degli articoli più discutibili di questo provvedimento, una sorta di qualificazione giuridica soggettiva di ognuna di quelle persone, quando l'obbligo di soccorso in mare in condizioni di pericolo oggettivamente ne prescinde, come ricorda peraltro in maniera categorica la Corte di cassazione nel famoso caso Rackete - che ovviamente tutti ricordiamo, perché fu oggetto di cronaca nel corso degli anni passati - quando afferma che le operazioni relative alle domande di protezione internazionale devono essere svolte in terra, solo una volta che i naufraghi siano stati messi in salvo. Ancora, Sottosegretario, violate i trattati internazionali, quando dite che il porto di sbarco deve essere raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso, lasciando intendere un divieto di salvataggi multipli, pretesa che peraltro non avverrà mai, perché ogni capitano, qualunque capitano al mondo che ha già prestato opera di primo soccorso, qualora dovesse venire a conoscenza di un'altra e nuova situazione di pericolo, naturalmente dovrà sempre prestare assistenza

La realtà che vi rifiutate di vedere è che queste navi di soccorso stanno riempiendo un vuoto che gli Stati europei hanno deliberatamente lasciato con l'interruzione delle proprie operazioni di soccorso. gliel'ho detto anche poco fa in Commissione: se volete impedire che i privati si sostituiscano all'autorità pubblica, come ha detto recentemente - sciaguratamente secondo me - il ministro Piantedosi, c'è solo un modo e io vi dico fin da subito che sarei d'accordo se lo faceste: ripristinare Mare nostrum. Ripristinatela! Quella missione, come qualcuno ricorderà, nacque in seguito a una delle più grandi tragedie che purtroppo ha riguardato il nostro Paese e il mar Mediterraneo: il naufragio di Lampedusa,

Ripristinate quella missione; anzi, se ci riuscite, fatelo come Europa e non semplicemente come Italia. Convincete gli altri Governi europei; convincete i vostri alleati degli altri Paesi europei, quelli che in Europa si oppongono a tutte le forme di redistribuzione e di cooperazione collettiva. Fatelo se ci riuscite. Noi di Alleanza Verdi e Sinistra vi invitiamo a non convertire in legge questo decreto-legge vergognoso e in ogni caso, signor Sottosegretario, Ministro, forze di maggioranza, sappiate che non lo farete in nostro nome. State violando la Costituzione, le leggi e i trattati internazionali. Per parte nostra, ci riconosciamo nelle parole della commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa: ritirate questo decreto-legge - ha detto - e assicurate che un nuovo testo sia pienamente conforme agli obblighi del Paese in materia di diritti umani e di diritto internazionale.

la volontà di creare una seria politica dei flussi migratori, cioè di gestire un fenomeno epocale, che contraddistingue la nostra epoca e che certamente non riusciremo a fermare con le mani.

che molti Paesi guardano al fenomeno migratorio anche con interesse perché tra i migranti ci sono persone che sono portatrici di competenze tecnico-professionali che sarebbero di grande interesse per il nostro Paese. Avremmo bisogno di lavorare con i Paesi rivieraschi; avremmo bisogno di lavorare tantissimo con i Paesi del resto d'Europa, di convincere l'Unione a lavorare in modo costruttivo per la ridistribuzione di coloro che arrivano nell'Unione europea, perché è evidente che oggi si arriva a Lampedusa come i nostri antenati arrivavano ad Ellis Island: non si arriva a Lampedusa perché è in Italia, così come non si arrivava a Ellis Island perché era nello stato di New York; si arriva a Lampedusa perché è nell'Unione europea. Purtroppo, però, il Governo non lavora nell'Unione europea per stabilire rapporti di collaborazione che possano sostenerci in questo sforzo;

alle esigenze italiane e che, anzi, ogni qualvolta si sia proposta una redistribuzione dei migranti, hanno girato il pollice verso il basso, facendo esattamente il contrario dell'interesse italiano, proprio perché noi siamo in una posizione anche geografica che ovviamente ci pone in una luce e in una prospettiva particolare rispetto ai flussi migratori. Oggi, però, non siamo qui a discutere del merito di questo provvedimento. Avremo modo di votare gli emendamenti e di fare le dichiarazioni di voto. Oggi parliamo in particolare del del fatto che, a nostro avviso, c'è una patente e manifesta incostituzionalità di questo decreto. Io credo non ci sia molto da dire dal punto di vista tecnico. Io ho ascoltato molti colleghi approfondire le varie questioni per le quali questo decreto si pone in violazione del diritto internazionale e della Costituzione. A me, però, basta dire una cosa molto semplice. Vi è una legge, Vi è una legge, che non è soltanto la legge del mare, la legge dei trattati e la legge delle convenzioni internazionali, ma è la legge dell'umanità. Essa dice che, di fronte ad una persona in difficoltà in mare, c'è da fare una e una sola cosa:

la legge morale dentro di noi e il cielo stellato sopra di noi, come diceva qualcuno più importante di me. Basterebbe dire questo. Ed è la stessa anima del nostro Paese che lo prevede. Signor Sottosegretario, questo decreto, di fatto, serve soltanto a complicare la vita a chi risponde a quella legge morale. È una sorta di salto ad ostacoli che viene posto posto davanti a chi fa il comandante di una nave e si trova ad aiutare delle persone. Succedono cose per cui a chi ha salvato 95 persone nel Mediterraneo viene detto che il porto al quale si devono dirigere

e portata a Foggia, a 750 chilometri di distanza e undici ore di viaggio in autobus. Ciò indica le intenzioni di questo decreto. È un decreto che non regolamenterà nessun flusso; è un decreto che creerà una serie di problemi burocratici, minacciando sanzioni irrogate dai prefetti senza un giudice terzo, sanzioni i cui presupposti amministrativi sono indeterminati. Insomma, sappiamo qual è la vostra tecnica legislativa. L'abbiamo imparata nel Governo Conte 1,

per prima cosa si salva chi è in difficoltà e che pone una serie di ostacoli pratici a chi quella legge dovrebbe applicare è certamente decreto anticostituzionale, incostituzionale e sicuramente questo sarà rilevato dall'alta Corte. Oltre, appunto, alla violazione delle convenzioni e dei trattati, c'è evidentemente un tradimento dello spirito della nostra Carta costituzionale, che è uno spirito solidaristico, che è lo spirito di chi dice che chiunque non possa godere delle libertà democratiche

signor Sottosegretario, ripeto che, indipendentemente da quelli che sono gli aspetti tecnici, esistono questioni morali, cui la nostra Carta costituzionale è ispirata, che sono evidentemente violate, tra l'altro, come qualche collega diceva, anche in modo inutile. I numeri parlano chiaro: quest'anno, tra il 1° gennaio e il 21 febbraio 2023, abbiamo avuto 12.372 sbarchi rispetto ai 4.701 dell'anno prima. per quanto vi diate da fare e cerchiate di fermare la storia con le mani, ciò non è possibile. Ciò che dovremmo fare è ribaltare questo tipo di approccio e fare ciò che è doveroso: da un lato, aiutare chi è in difficoltà. Questa è la prima cosa che va fatta. Io sono stato orgogliosamente componente di un Governo che, non è soltanto andato a salvare chi annegava nel Mediterraneo, ma è andato addirittura a dare sepoltura a chi era morto. E lo abbiamo fatto perché questa è la nostra cultura, perché noi siamo la cultura di Antigone. Noi diamo sepoltura ai morti e aiutiamo le persone che sono in difficoltà, e questo è fuori discussione; è il punto di partenza che dovrebbe accomunarci tutti. Partiti da lì, stabilito questo, l'accordo su questo punto su quale, secondo me, non dovrebbe neanche esserci discussione, perché dovrebbe appartenere a tutti, dovremmo poi provare ad avere un approccio razionale al fenomeno migratorio: le quote, gli accordi con i Paesi rivieraschi e quant'altro. Arrivare qui - ripeto - con un decreto-legge che abbiamo potuto esaminare soltanto molto rapidamente, che sembra voler esclusivamente penalizzare le ONG,

pregiudiziale presentata dal Partito Democratico e a dichiarare ufficialmente che questo provvedimento di legge non ha nulla a che vedere né con la lettera né con lo spirito della Carta costituzionale democratica e repubblicana che ci lega tutti.

di costituzionalità, che legittimamente è stata posta. Voglio dire che stiamo discutendo di questo provvedimento, peraltro, con una calendarizzazione fissata a questa settimana - scadendo il decreto-legge marzo - proprio perché, anticipando la discussione in termini assolutamente fisiologici, ci sarebbe lo spazio anche per eventuali modifiche che dovessero essere riesaminate dalla Camera. Quando si discute l'ultimo giorno, invece, c'è un effetto tagliola; quindi, secondo me, anche la calendarizzazione è ancora più rispettosa della possibilità di confronto. Per quanto riguarda il tema che viene affrontato, voglio richiamare l'Assemblea su un *vulnus* che abbiamo subito mesi fa. Era la scorsa legislatura; io ero Presidente della Giunta delle elezioni che si è occupata di alcuni casi riguardanti l'immigrazione. Ricorderà anche il presidente Centinaio che molte questioni riguardavano l'allora Ministro dell'interno del Governo dell'inizio dell'altra legislatura, che era il Ministro Salvini. Per tre volte ci sono state delle accuse: una volta il Senato le ha respinte, anche con il voto dell'Assemblea; altre volte ci sono state valutazioni diverse; è in corso un processo a Palermo. Dopodiché, abbiamo appreso che la Marina italiana aveva fornito a ben sette procure notizie notizie rilevanti ai fini del voto che l'Assemblea espresse, e che - lo posso dire da relatore di quella vicenda - nell'incartamento non abbiamo mai ricevuto. Colgo l'occasione per dire che, se c'è qualcosa di incostituzionale, non è nei decreti-legge del Governo, ma nelle condotte di alcune procure della Repubblica italiana, che non hanno informato il Parlamento di ciò che sapevano. *(Applausi)*. Questo è molto grave, ragion per cui colgo questa occasione per dirlo. Di che cosa parlo? Del fatto che, a suo tempo, un sommergibile della nostra Marina aveva controllato l'operato di alcune imbarcazioni delle ONG e aveva intercettato

questi materiali. Il sommergibile e altri mezzi militari hanno intercettato il dialogo ONG-trafficanti e lo hanno mandato a sette procure della Repubblica;

più di sette - avevano questi materiali e quando il Parlamento ha ricevuto gli incartamenti per prendere le decisioni proprie, se Salvini avesse agito in qualità di Ministro, nel rispetto dei principi costituzionali o meno, questo materiale non è pervenuto al Parlamento. La magistratura di queste città ha sottratto al Parlamento materiali essenziali per le nostre decisioni. Questa è violazione della Costituzione, perpetrata da sette procure della Repubblica. sì, lei fa questi gesti, senatore Nicita, ma è una violazione; lei non era senatore. Noi abbiamo deciso senza conoscere gli atti che sono stati nascosti al Parlamento, questo è un attentato a organi costituzionali da parte di sette procure della Repubblica. alle quali, qualche settimana fa, apprese queste notizie che non conoscevo (ero relatore e Presidente della Giunta e non conoscevo questi atti, abbiamo lavorato sugli atti che ci sono stati rimessi dalle procure)

una procura su sette. Da quest'Aula dico: vergogna, procuratori che non rispondete al Parlamento delle omissioni che avete fatto! Vergogna, vergogna e vergogna! Le ho citate, le procure, perché non temo nessuna ritorsione da parte di nessuno. Questo, colleghi, per dire che la violazione della Costituzione è quella che fanno alcune toghe, che hanno impedito al Parlamento di decidere con informazioni complete e l'operato di alcune ONG è quello che queste intercettazioni hanno rivelato, il *pull factor*: vanno lì, si mettono d'accordo, i trafficanti mettono natanti pericolosissimi in mare e si moltiplicano le tragedie. Perché la verità è che il cimitero Mediterraneo diventa tale in maniera più grave se si moltiplicano certi viaggi e le attività degli scafisti.

(vedo che ci sono senatori che lo ricordano) e alcuni vennero con atteggiamento timoroso e non volevano venire (come gli spagnoli), ma comunque vennero e accertammo una serie di questioni. Si arrivò al codice di regolamentazione delle ONG, il codice Minniti, e conteneva una serie di direttive sostanzialmente simili al contenuto di questo decreto. Grazie, quindi, al ministro Piantedosi, che non dovete insultare, perché insieme al Governo ha assunto una decisione coerente con l'attività conoscitiva conoscitiva del Senato e del Parlamento, con l'azione che anche il ministro Minniti svolse, cercando di contenere queste attività che andavano oltre le richieste. Per quanto riguarda la questione dei salvataggi, potrei citare - ma il tempo si sta esaurendo le accuse fatte a Casarini, uno di quelli che hanno fatto i centri sociali del mare. Secondo alcune accuse, la sua ONG avrebbe preso addirittura dei soldi per prelevare delle persone.

un'azione comune. Noi siamo in mezzo al Mediterraneo, siamo il primo approdo, ma non possiamo essere l'unico punto di arrivo della disperazione dell'Africa, che va affrontata con il piano Mattei, con un piano Marshall, con politiche internazionali di aiuti per mitigare la miseria, le difficoltà, i cambiamenti climatici, tutte le cose di cui parliamo ma che non sono un problema che solo l'Italia può affrontare. Qualcuno disse al momento sono quattro le Nazioni più esposte nel Mediterraneo: Cipro, Grecia, Italia e Spagna e che ogni Governo europeo dovrebbe mettersi d'accordo su quanti migranti può ricevere, che la politica sui migranti dovrebbe essere consensuale tra i Paesi europei, secondo il principio di collaborazione, non è possibile abbandonare a loro stesse le quattro Nazioni più esposte geograficamente, con tutti i migranti che arrivano sulle loro spiagge. Sapete chi l'ha detto? Il Santo Padre, Papa Francesco. Noi, quindi, non solo siamo nel solco della Costituzione, ma nel solco di una solidarietà possibile che deve avere dei limiti, delle condivisioni, delle collaborazioni, che anche il Santo Padre, sensibile a questi temi, ha più volte richiamato. Cari colleghi, noi riteniamo che sia legittimo esporre gli argomenti che sono stati qui illustrati da altri colleghi, sia legittimo da parte nostra e, quindi, anche del Gruppo Forza Italia, ritenere non fondate le eccezioni di costituzionalità. La normativa - ne discuteremo quando poi affronteremo il merito nelle prossime sedute - è assolutamente coerente con la necessità di una solidarietà possibile, ma di una sicurezza necessaria nel mitigare politiche demagogiche anche di Paesi che danno le bandiere dei loro Stati alle navi delle ONG, ma poi non gli rispondono quando portano i clandestini. Se dai la bandiera, ti devi caricare anche la responsabilità morale e materiale di coloro che arrivano. Non è possibile infatti che la bandiera conti per certi aspetti, ma poi non conti quando è il momento dei doveri, della solidarietà e degli oneri e materiali. Siamo perciò d'accordo con quello che il centrodestra ha detto in Italia e in Europa, siamo d'accordo con quello che accertò il Senato in altre legislature e che altri Governi, con Ministri di schieramenti diversi distanti dal nostro, fecero. Riteniamo che contenere questi viaggi e questa azione

una discussione non facile, di difficile soluzione, ma doverosa. L'Italia ha fatto e fa molto in termini di solidarietà, ha tutto il diritto di fare tanto in termini di sicurezza. di sicurezza. Questo vuol dire rispettare la Costituzione, non come quelle sette procure che hanno omesso la comunicazione al Parlamento di atti doverosi ed è questo un motivo di riflessione che fa capire quanto sia necessario riformare la giustizia e imporre il rispetto della sovranità popolare che viene rappresentata dal Parlamento e non dalle procure della Repubblica.

non è così, sa che nell'*hotspot* di Lampedusa vi sono 2.700 migranti arrivati con mezzi propri, sa che sono arrivati solo in questo fine settimana 400 migranti su 60 barchini. Il punto è non demonizzare per deviare l'attenzione da un problema che, come è stato detto prima di me, è molto grande, che certamente ti strappa dalla retorica della propaganda elettorale. Però avete Però avete vinto le elezioni, avete vinto le elezioni politiche e le regionali, le avete vinte in maniera netta, chiara e questo vi dà il titolo per governare e legiferare.

potete tagliare tutto, ma non potete passare sopra la Costituzione. *(Applausi)*. Questo non potete farlo perché viviamo all'interno di un ordinamento giuridico generale che addirittura poi va ad estendersi all'interno di un diritto internazionale, che deve fare i conti con il diritto della navigazione e potete fare tutto con i voti che avete anche in quest'Aula, ma una cosa non potete farla: non potete contrastare l'omissione di soccorso in mare. Questo infatti ve lo impediscono la Costituzione e il diritto. E non sto parlando di etica, non sto parlando di morale, non sto parlando di quei valori universali di cui hanno parlato egregiamente i colleghi che mi hanno preceduto: il valore della solidarietà, il valore del mutuo soccorso, il valore della condivisione, Non sto parlando di etica; sto parlando di legge. E allora, che questo decreto sia un mostro legislativo inapplicabile nella pratica non ve lo stiamo dicendo solo noi; ve l'ha già detto il Consiglio d'Europa, ve l'hanno già detto le Nazioni Unite e ve l'ha detto anche la sentenza di un tribunale, di quei cattivi magistrati che ce l'hanno con voi e che non vedono l'ora, ogni volta, di nascondervi i documenti, di modificarli e di manipolarli. Sono magistrati cattivi, va bene. Ma c'è una cosa che vi deve far sentire l'obbligo di frenarvi: la Carta costituzionale, i principi e i valori della Costituzione. E questo è un decreto che viola i dettami della Carta costituzionale. Ho concluso.

sostanzialmente preso il codice di condotta che portò avanti il ministro Minniti nel 2017 e lo ha trasformato in una norma di legge, la domanda è: come mai tutte queste pregiudiziali di costituzionalità, legge del mare, trattati internazionali, Consiglio d'Europa, tutto quello che ho sentito in quest'Aula in questo scorcio di pomeriggio ai tempi nessuno osò portare avanti? *(Applausi)*. È solo una domanda, vorrei capire come mai. Dalla risposta comprendiamo perché tanti cittadini e tanti elettori siano un po' disgustati dalla politica e non vadano a votare.

a molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che ogni straniero è nemico. Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi come una infezione latente. Si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati e non sta all'origine di un sistema di pensiero. Ma, quando questo avviene, quando il dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora, al termine della catena, sta il *lager*. Esso è il prodotto di una concezione del mondo portata alle sue conseguenze con rigorosa coerenza. «Finché la concezione sussiste, le conseguenze ci minacciano»: sono parole di Primo Levi, straordinarie per la loro chiarezza e terribili per il loro contenuto; parole che ricordai in occasione dell'approvazione dei cosiddetti decreti Salvini, poi dichiarati in più parti incostituzionali. Sono parole che ho voluto riprendere oggi, perché sollecitano alla prudenza, alla necessità di mitigare e ricondurre a ragionevolezza le paure e le pulsioni all'intolleranza che albergano in ciascun essere umano. Parole di saggezza, di umanità e di esperienza, che credo siano state dal Governo nuovamente trascurate, perché è del tutto irragionevole e di dubbia legittimità - come ha ben spiegato il senatore Parrini - ostacolare le operazioni di soccorso, obbligando ad esempio le navi delle ONG, dopo un'operazione di salvataggio, a raggiungere senza ritardo il porto assegnato per lo sbarco, impedendo così che esse compiano salvataggi multipli. È del tutto irragionevole assegnare alle imbarcazioni un porto di sbarco molto lontano dall'area in cui è avvenuta l'operazione di soccorso. infatti del tutto irragionevole e contrario alla consolidata giurisprudenza considerare adempiuto il dovere di soccorso con il solo salvataggio dei naufraghi a bordo delle imbarcazioni, senza che vi sia altresì lo sbarco degli stessi in un luogo sicuro, cioè in un luogo nel quale le operazioni di soccorso si considerano concluse, la sicurezza dei sopravvissuti e la loro vita non è più minacciata, le necessità umane primarie come cibo, alloggio e cure mediche possono essere soddisfatti e può essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale.

oltre ad essere in balìa degli eventi meteorologici avversi, non consente il rispetto dei diritti fondamentali delle persone migranti soccorse, fra i quali va incluso il diritto a presentare domanda di protezione internazionale. che senso abbia, quale giustificazione giuridica e prima ancora politica e umana possa avere costringere le navi delle ONG a percorrere lunghi tratti di navigazione per condurre a terra le persone salvate e, al tempo stesso, costringere le ONG a ignorare ulteriori richieste di soccorso nelle vicinanze, nel caso in cui abbiano già a bordo persone tratte in salvo, anche quando avrebbero ancora la capacità di effettuare un altro salvataggio. Il Governo non sembra però aver prestato alcuna attenzione all'ammonimento di Primo Levi, anche perché non ha reso possibile che di queste considerazioni di merito e di altre preoccupazioni sollevate da moltissime associazioni si discutesse e lo si facesse in maniera adeguata. Il ricorso alla decretazione d'urgenza - e vedremo se fra poco verrà apposta la fiducia - ha infatti mortificato il confronto parlamentare e tolto ogni spazio alla forza degli argomenti. Per queste ragioni vi diciamo di fermarvi; avviamo un confronto pubblico vero, aperto, nell'interesse del Paese, della legalità e di una convivenza rispettosa dei principi costituzionali e del diritto internazionale, a partire dal fondamentale diritto alla vita, che deve essere garantito a ogni essere umano, quale che sia la sua cittadinanza.

Vediamola allora questa pregiudiziale per come è stata presentata dai colleghi del Partito Democratico, appoggiati anche dagli altri colleghi della minoranza. Essa si incentra fondamentalmente su alcuni aspetti:

Penso di poter dire tranquillamente, a nome di Fratelli d'Italia, che tutti questi punti sono da noi assolutamente rigettati, perché non hanno nessuna compatibilità con quanto viene detto.

e, quando ho sostenuto l'esame di diritto pubblico, già al tempo la dottrina diceva che c'era una esagerazione di decreti-legge con cui il Governo legiferava sostanzialmente al posto del Parlamento: stiamo parlando della fine degli anni '80.

condannava l'eccessivo uso dei decreti-legge. Sono andato allora a vedere chi governava nel 2007: Governo Prodi, con ministro D'Alema. Parliamo di Governi di centrosinistra, che abusavano dei decreti-legge

ancora una volta qualcosa. Oggi, ancora una volta, ripeto, c'è qualcuno da quei banchi che viene a fare la morale perché Fratelli d'Italia e il Governo di centrodestra usano il decreto-legge per legiferare una materia che invece è assolutamente di necessità ed urgenza. Vediamo il merito di quello che dite. Si fa riferimento in particolare al comma 2-*bis*, per cui per cui il decreto-legge prevede le «iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità». Che senso ha scrivere questo quando un simile elemento è già stato superato? superato? È stato ampiamente detto e dimostrato che tali attività non sostituiscono le procedure europee, nel senso che l'informativa a bordo non preclude la possibilità di presentare la domanda a terra e che la raccolta di dati rilevanti non è l'identificazione, che compete ad autorità diverse.

deve essere raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso. E qui entra in scena il vostro supereroe, la commissaria dei diritti umani del Consiglio d'Europa: se c'è qualcuno che in giro per il mondo parla male dell'Italia, voi lo assumete subito come vostro riferimento immediato.

Peccato che non scrivete che il ministro Piantedosi abbia prontamente risposto su questo elemento che la commissaria sottolinea, dicendo che le condizioni previste da questo aspetto sull'immediata richiesta del porto sicuro e il suo raggiungimento senza ritardo non impediscono alle ONG di effettuare interventi multipli in mare e a provvedere ad eventuali ulteriori richieste di soccorso nell'area, anche qualora abbiano già preso a bordo delle persone. Ma allora di che cosa stiamo parlando? *(Applausi)*. Abbiamo già risposto su questo ed è già tutto chiaro, a meno che non sia un elemento surreale pensare che una nave prenda a bordo delle persone che sono in difficoltà e stia lì a navigare tranquillamente come se queste persone non avessero bisogno di aiuto, in attesa che forse qualcuno telefoni, come qualcuno ha ricordato prima, perché ci sono altre persone da prendere a bordo. un tema risolto e già chiaro, non c'è bisogno di dire altro. Voi parlate del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite perché non potete parlare di un'altra istituzione che invece è rimasta silenziosa, l'Unione europea, che su questo non ha detto niente. Il commissario dell'Unione europea su questo tema non ha fatto nessun rilievo al decreto-legge del nostro Governo. Guarda caso, parlate solo di alcuni enti, mentre di altre istituzioni, che potrebbero davvero entrare nella nostra legislazione e che potrebbero fare dei rilievi l'Unione europea non ne

sbarcandole in situazioni di caos? Perché dobbiamo riempire Lampedusa, la Sicilia, la Calabria, quando sappiamo che quegli *hot spot* e quei luoghi sono già al collasso e che quindi è normale, giusto e doveroso anche nei confronti di queste persone portarle in altri porti dove possono essere assistite meglio? che forse, al di là della solidarietà che pontificate in maniera astratta, avete paura che queste persone rovinino le vostre spiagge *radical chic* di Capalbio e di altri luoghi *(Commenti)*, dove invece queste persone non le volete assolutamente incontrare.

nel quale c'è solo il tentativo di mettere in pratica il buon senso e di superare davvero ogni pregiudizio, questo sì, di carattere ideologico.

Grazie,

per riferire sui lavori della 1a Commissione. Il disegno di legge di conversione n. 553 è stato esaminato nella giornata di ieri e nella giornata di oggi.

Questo provvedimento - ripeto - è stato esaminato nella giornata di ieri e nella giornata di oggi. Tuttavia, non siamo riusciti come Commissione a concludere l'esame e la votazione Grazie, cui abbiamo dedicato pochi minuti, e poi abbiamo dovuto interrompere per venire in Aula. Quindi, non abbiamo un relatore e non abbiamo concluso i nostri lavori. Tuttavia, se mi permette, vorrei fare una precisazione in merito a quanto ha detto il senatore Parrini, perché i tempi per esaminare e concludere questo provvedimento in Commissione ci sarebbero stati, soltanto che ieri nel corso della discussione generale il Gruppo PD, che pure ha quattro rappresentanti in 1a Commissione, non si è presentato. A quel punto, per garbo istituzionale, ho ritenuto di non dichiarare chiusa la discussione generale in Commissione, come avrei potuto fare, visto che altri Gruppi avevano chiesto la parola e nessuno più la richiedeva,

generale. Oggi il Gruppo PD si è presentato al completo, ha impegnato tutto il tempo a sua disposizione nella discussione generale

In sostanza, le due ore che oggi avremmo potuto impegnare, secondo le nostre previsioni, nell'esame degli emendamenti, sono stati impegnati (per una scelta legittima - sia ben chiaro - delle opposizioni) nella discussione generale.

a questo punto, però, non mi sembra nemmeno logico che la stessa opposizione, dopo aver fatto tale scelta legittima

che ci fosse più tempo a nostra disposizione, perché due giornate per un provvedimento così importante e anche così divisivo, su cui

e che la Conferenza dei Capigruppo impone di esaminare con tempi irragionevolmente ristretti, non è stata una gentile concessione, ma un suo preciso dovere e mi aspetto che lo assolva nello stesso modo se dovesse ripresentarsi questa occasione. *(Applausi)*. Spero che ci siamo intesi. In secondo secondo luogo, credo di sapere qualcosa di come si conduce la Commissione: l'ho fatto per due anni e nessuno ha fatto mai un intervento in Aula come quello che io sto facendo contro il mio modo di condurre la Commissione.

tante sono le falle, le irragionevolezze e le norme contrarie alla Costituzione. Come il presidente Balboni ben sa, sul complesso degli emendamenti ciascuno dei presentatori può intervenire per cinque minuti, articolo per articolo, sugli emendamenti che ha presentato a quell'articolo; le due ore e mezzo le avremmo quasi quasi esaurite per illustrare il complesso degli emendamenti e ben poco sarebbe rimasto per votare i singoli emendamenti, su ognuno dei quali è possibile intervenire per cinque minuti per motivare il voto. Questo intervento, peraltro, non è senz'altro ostruzionismo: si chiama semplice esercizio di un diritto di democrazia previsto dal nostro Regolamento. *(Applausi)*. Mi dispiace molto aver dovuto prendere la parola, ma noi diciamo alla maggioranza che è suo diritto presentare il decreto-legge

e se ne assume la responsabilità. Noi non lo abbiamo condiviso ed io, quando sono intervenuto in sede d'illustrazione della questione pregiudiziale, ho evitato, per tutta la delicatezza e per il tatto che bisogna avere in Parlamento e che il presidente Balboni ha dimostrato di non avere, di dire per quale ragione la maggioranza ha imposto tempi irragionevolmente ristretti alla discussione di questo decreto-legge. Ci dicano come mai non era possibile esaminare il decreto-legge la prossima settimana, ma abbiamo dovuto farlo in questa, anche se il provvedimento scade il 3 marzo. Lo sappiamo: non è stato possibile perché in Conferenza dei Capigruppo è stato detto che ci sono Gruppi che devono partecipare a una riunione di partito di là dall'oceano, in Florida. Vi auguro che ci siano il sole e grandi occasioni di crescita civile e culturale, ma in questo caso i diritti dell'opposizione sono stati gravemente lesi, non abbiamo avuto il tempo di esaminare l'argomento e nessuna ricostruzione faziosa può alterare questa realtà. apre una nuova finestra"). Ricordo al senatore Balboni, come a tutti i colleghi senatori, che la decisione in Conferenza dei Capigruppo è stata presa all'unanimità e di conseguenza non c'è stato nessuno che si sia opposto

è l'ultima volta che ci sarà. Da oggi in poi voteremo sempre in Aula il calendario dei lavori e finirà così anche questa modalità di lavoro, visto che i fatti vengono riportati all'opposto di come si sono determinati. vorrei intervenire brevemente per precisare due aspetti. Il senatore Parrini ha detto che nella scorsa legislatura non vi sono mai stati interventi in Aula come quello che lui stava per fare. Questo può anche voler dire che, forse, chi era all'opposizione nella scorsa legislatura ha pensato di gestire le cose in Commissione non sempre con piena soddisfazione. Do atto della correttezza generale del senatore Parrini, Presidente della Commissione affari costituzionali nella scorsa legislatura, ma il fatto che abbia fatto una protesta in Aula

Quanto alla questione che è stata sollevata in seguito, è stato menzionato, tra le ragioni per votare questa settimana, per trasparenza, che c'è una riunione che non è precisamente un raduno balneare, ma una riunione a livello internazionale di partiti che appartengono a una coalizione internazionale. Non si svolge in Florida - questo è stato un mio errore, perché ce n'era stata una analoga che si era svolta lì - ma nella più severa Washington. Non cambia nulla a mio parere, però mi dispiace di averla indotta a fare gli auguri per le spiagge, che a Washington mancano; ma questo perché avevo citato una città diversa. Quanto ai tempi, ricordo che il decreto-legge scade il 3 marzo,

tendiamo a non voler apportare modifiche per evitare problemi in un ulteriore passaggio alla Camera, ma, ove mai delle modifiche fossero fatte - tante sono state proposte dall'opposizione - bisogna avere il tempo per un eventuale ulteriore passaggio, che comunque ritengo non ci sarà, ma che l'opposizione chiede che ci sia.

finestra"). Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Balboni, il disegno di legge n. 553, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento. Dichiaro aperta la discussione

vorrei interpretare le parole dell'ultimo intervento del senatore Malan come il fatto che il Governo non si appresta a mettere la fiducia e che noi dalle dalle prossime ore cominceremo l'esame emendamento per emendamento in quest'Aula per decidere di questo provvedimento. Se così non fosse, trovo la discussione che c'è stata finora un dibattito fatto a non dirci come stanno le cose e come

pensiamo sia anticostituzionale. In realtà, non è che lo pensiamo; vediamo le caratteristiche di violazione della Costituzione, anche se voi

il Ministro ha affermato che una delle ragioni per cui bisognerebbe evitare che ci sia l'arrivo di migranti e di rifugiati attraverso la via del Mediterraneo è quella che poi non avranno una collocazione, rimarranno marginali e si faranno sfruttare. Non c'è dubbio che nel nostro Paese si sfruttino i migranti; ne abbiamo ampia documentazione e ampi processi. Questo Parlamento, non moltissimo tempo fa, ha dovuto approvare una legge sul caporalato esattamente per intervenire contro questi processi. Ciò che appare un po' strano, però, è che siano le persone a farsi sfruttare, non che ci siano degli sfruttatori. È esattamente questo rovesciamento della logica che non fa vedere il perché continueranno a esserci persone sfruttate se non utilizziamo la parte propositiva, e cioè come concretamente si costruiscono i processi di integrazione. Di questo ha bisogno il nostro Paese, salvo che voi non continuiate a pensare una cosa che non trova alcuna ragione nella storia del mondo, ovvero che ci siano un modo o una possibilità di fermare i flussi migratori.

direi che poi si fa fatica a dire che si è persone, che si è umani e che si hanno delle ragioni. In questo caso, non c'è neanche bisogno di scomodare la Costituzione. Voi dite spesso - l'avete detto anche poco fa in quest'Aula che dovremmo essere preoccupati, se importanti istituzioni del resto del mondo parlassero male dell'Italia. Io sono molto preoccupata, soprattutto se lo fanno il Commissario delle Nazioni Unite a proposito della Convenzione sui diritti umani o il Commissario europeo sui diritti umani, perché nelle loro parole sento che si dice a questo Paese che non ha il coraggio, la capacità e la voglia di allungare una mano e dare una risposta a chi è in grande difficoltà.

temo che siamo noi a non riuscire a mostrare un volto dell'Italia in grado di affrontare i problemi che ha dando le risposte giuste e necessarie. *(Applausi)*. Quando si ha paura dei complotti, si fanno sempre grandi disastri nell'analisi di ciò che succede intorno a noi. Vengo a un'altra affermazione che ho sentito sempre nelle trasmissioni di questa mattina: poiché i blocchi navali - per fortuna - non si possono fare e quindi a quelli avete rinunciato,

vorrei usare le parole che sono state usate anche in quest'Aula: non in mio nome. Mi bastano gli accordi che sono stati fatti con la Libia, quelli che determinano che l'Italia è il Paese finanziatore delle torture, dei *lager* e dell'impossibilità per quei migranti di raggiungere il nostro Paese o i Paesi europei in condizioni sane. *(Applausi)*. La Turchia riceve molti soldi dall'Europa, anche dal nostro Paese, perché l'Europa ha pensato che in questo modo non ci sarebbe stato l'arrivo in particolare dei siriani, il cui Paese, com'è noto, è in guerra da dodici anni e che in questo momento sta affrontando anche quella piccola cosa che è un tremendo terremoto e fa fatica a ricevere gli aiuti, perché per darglieli bisogna togliere le sanzioni che abbiamo messo nei confronti di quel Paese e devo dire che per fortuna gli Stati Uniti l'hanno fatto. trovano in campi, spesso sono stati visitati da commissari europei e da delegazioni europee che non ci hanno raccontato della migliore delle soluzioni e delle ospitalità possibili. Non solo, ma da qualche tempo, nell'indifferenza totale, anche nostra, progressivamente quelle popolazioni siriane che sono nei campi vengono spostate nelle terre curde, da cui vengono cacciate attraverso i bombardamenti i legittimi abitanti. Ebbene, io non farei mai un paragone e non direi mai che potremmo affrontare il tema dei flussi migratori continuando ad alimentare accordi monetari che allontanano da noi il problema, ma creano ulteriori rifugiati e ulteriori persone bisognose di protezione

il resto del mondo si è aperto a noi, perché se Paesi vicini a noi - penso alla Gran Bretagna - avessero la stessa opinione rispetto ai giovani italiani, saremmo in grande difficoltà, perché ci sarebbe qualche centinaio di migliaia di nostri concittadini senza le soluzioni di lavoro e di integrazione che invece in quel Paese gli vengono offerte. Rammento a tutti voi che, quando si discuteva la Brexit, il sottofondo di quella discussione era la necessità di salvaguardare le condizioni dei nostri concittadini, perché non avremmo voluto trovarci di fronte al fatto che venissero considerati come stranieri o clandestini. Infine, concludendo, vorrei proporvi la necessità di riflettere su un altro aspetto; abbiamo parametri un po' vecchi, con i quali definiamo chi è un migrante, chi un rifugiato, chi un richiedente protezione e così via. di parametri un po' vecchi perché le ragioni per cambiare Paese e per allontanarsi da un territorio cambiano nel tempo. Qualche volta perché non le vediamo in ragione della politica, come quando non vediamo i bombardamenti in Yemen; qualche volta perché non ci rendiamo conto che i cambiamenti climatici sono molto più veloci di quello che ci immaginiamo. Una delle ragioni però per cui potremmo invece provare a capire queste cose è non fare quello che avete fatto con la legge di bilancio, non decidere cioè che non ci sia il personale addetto alle questure, alle prefetture o al Ministero dell'interno che si occupa della protezione umanitaria. infatti questo strano *record* per cui vorremmo che andassero nel porto più lontano, che poi si trasferissero in autobus, che poi si mettessero in coda alle questure e che poi non ottenessero comunque risposte, perché non c'è il personale. A me pare più una persecuzione che una scelta di risposte positive.

provvedimento che oggi siamo chiamati a trasformare in legge sottende allo scopo e all'intento di ricondurre l'attività di soccorso delle navi ONG nelle maglie del diritto internazionale, coniugando il dovere di assicurare l'incolumità delle persone recuperate in mare con l'esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. Ciò perché negli ultimi anni si è alimentata una situazione di totale illegalità ed è ora di dire basta. Non si può permettere che le navi ONG pattuglino il Mediterraneo per giorni con centinaia di persone a bordo, per dirigersi in porto solo una volta raggiunta la capienza massima. Non si può permettere che una nave ONG effettui fino a sette interventi in settantadue ore senza alcun coordinamento con il soccorso italiano, com'è capitato alla Geo Barents lo scorso novembre prima di approdare a Catania con ben 572 migranti a bordo. È palese che la Geo Barents non si è imbattuta in situazioni di pericolo, ma è andata in cerca di migranti da trasferire sulla propria imbarcazione. Le nuove norme vogliono regolamentare proprio la questione dei salvataggi multipli, uno degli aspetti più controversi dell'operato delle ONG, le quali, anziché intervenire su una singola situazione di rischio, restano in mare per giorni, effettuando diversi trasferimenti prima di condurre i migranti in un porto sicuro, comportandosi di fatto come veri e propri traghetti che fanno la spola da una sponda all'altra del Mediterraneo. Che cosa dicono queste nuove norme? Dicono che nell'immediatezza dell'evento di soccorso la nave ONG deve richiedere l'assegnazione del porto di sbarco che dovrà essere raggiunto senza ritardo. Mi sembra normale e intuitivo, visto che parliamo di soccorso in mare, che normalmente viene offerto ai naufraghi. Naufrago ha un significato ben preciso: è il superstite di un naufragio,

Senatore Nicita, per favore, lasci intervenire la collega e porti rispetto per quello che sta dicendo. Scusi,

la collega si prende la responsabilità di quello che dice, ma chiedo di non parlarle sopra. È una questione di rispetto e di educazione. Altro argomento: non si può pretendere che il porto più sicuro sia necessariamente anche quello più vicino. Intanto, occorre fare chiarezza: il porto più sicuro è, per definizione, quello in cui si considerano terminate le operazioni di salvataggio, cioè quel luogo in cui, nel caso dei sopravvissuti, questi non si trovano più esposti a un rischio per le loro vite; nel caso dei migranti, è il luogo dove questi ultimi possono accedere a tutte le procedure per ottenere un passaggio verso la destinazione finale. Per cui, considerato che, una volta intervenuto il soccorso, i migranti presenti sulle navi ONG non sono più in condizioni di pericolo per la propria incolumità e considerato che quelle delle ONG sono spesso navi di grande cabotaggio, che dunque possono affrontare serenamente tratte di navigazione considerevoli in assoluta sicurezza (come ricordo è avvenuto per la Ocean Viking), non si capisce perché il Governo italiano non possa decidere quale sia il luogo più adeguato per far sbarcare i migranti ed evitare che si creino situazioni emergenziali e indecorose come quella di Lampedusa, in cronico sovraffollamento. perché no a porti come Ravenna, Ancona, Genova o Livorno? Vogliamo essere solidali con le Regioni del Sud, costrette a farsi carico dei continui arrivi, oppure no? Nel 2022 sono arrivati 105.140 stranieri irregolari, per la stragrande maggioranza migranti economici, provenienti da Egitto, Tunisia e Bangladesh, non da Siria e Afghanistan, dove sono in corso crisi ed emergenze sanitarie. Dei 105.140 stranieri arrivati, 11.892 sono stati condotti a terra dalle ONG, ossia l'11 per cento del totale. Certo, non sono numeri trascurabili in termini assoluti, però non bastano a giustificare la narrazione degli attivisti che descrivono le ONG come gli unici occhi che vedono cosa succede nel Mediterraneo. Infatti, la stragrande maggioranza dei soccorsi viene operata dalla Guardia di finanza, dalla Guardia costiera e dalle navi della Marina, a cui va sempre il nostro ringraziamento. Per cui, voler regolamentare le attività di queste organizzazioni nel Mediterraneo non significa mettere a repentaglio la vita dei migranti o far crescere il numero dei morti in mare; significa contribuire a disincentivare le partenze irregolari, considerato che - come ha rilevato anche Frontex il pattugliamento delle navi umanitarie davanti alle coste della Tripolitania è stato identificato più volte come un fattore di attrazione per i migranti. Delle 11.892 persone condotte in Italia dalle ONG, 11.076 provengono dalla Tripolitania, cioè il 93,2 per cento È del tutto chiaro che l'attività delle ONG è concentrata su quella rotta e che la loro presenza abbia un effetto incentivante sulle partenze da quell'area. Con queste nuove disposizioni viene finalmente regolamentata una situazione lasciata a sé stessa, in cui

e vanno rispettati anche i migranti, perché chi sta rischiando la vita ha diritto a essere salvato. Cosa diversa, invece, è farsi utilizzare dalla tratta degli esseri umani del terzo millennio e continuare a far fare miliardi di euro agli scafisti. Con queste norme il Governo pone un primo tassello per contrastare l'immigrazione illegale e interrompere il *business* dei trafficanti, perché migranti e profughi sono due cose diverse e si gestiscono in maniera diversa.

ha riconosciuto l'immigrazione come un problema europeo che necessita di un approccio globale; piccoli ma importanti passi per trovare soluzioni efficaci a temi sui quali fino a oggi soluzioni efficaci non ne sono state trovate, perché l'approccio è sempre stato ideologico, quando ideologico non dev'essere. Concludo. La crisi energetica offre un'occasione all'Europa di tornare a essere presente in Africa, dove, avendo indietreggiato negli anni precedenti, lo spazio vuoto è stato riempito da Cina, Russia e Turchia. L'Italia può diventare Nazione capofila nella creazione di un modello virtuoso di collaborazione e di crescita tra l'Unione europea e le Nazioni africane; un modello basato su un approccio collaborativo, che garantisca sviluppo, dignità e lavoro, nonché il sacrosanto diritto di non dover emigrare, perché - come diceva Papa Benedetto - prima di garantire il diritto di emigrare, bisogna garantire il diritto di non doverlo fare.

il decreto-legge oggi in conversione segna un preoccupante e significativo arretramento in materia di protezione dei diritti umani fondamentali e colloca con le sue scelte l'Italia in una posizione molto difficile e molto complicata nei confronti della comunità europea e di tutta la comunità internazionale. I limiti penetranti che questo decreto impone alle imbarcazioni che svolgono operazioni di soccorso in mare nel Mediterraneo centrale violano molteplici obblighi internazionali e contravvengono a un elementare principio di civiltà umana, che quegli stessi obblighi incarnano: in mare si soccorre chi è in difficoltà e lo si conduce con semplicità nel porto più vicino. Il Governo dall'autunno scorso ha reso difficile, se non impossibile, il rispetto di questo essenziale principio: imbarcazioni costrette a navigare per giorni, con il loro carico di sofferenza e di dolore, per raggiungere porti lontani come La Spezia o Ancona; uomini, donne e minori costretti a vivere e a rivivere il trauma del viaggio in mare e del naufragio, talvolta in condizioni metereologiche davvero complicate, e, una volta sbarcati, costretti a nuovi e lunghi viaggi via terra per raggiungere i centri di accoglienza. È così accaduto che persone - talvolta tanti minori - salvate di fronte alle coste della Sicilia e sbarcate a La Spezia abbiano poi addirittura dovuto percorrere 700 chilometri in un autobus per raggiungere Foggia.

Lo ha affermato la Commissione per i diritti umani del Consiglio d'Europa, che il 26 gennaio ha invitato il Governo a ritirare il decreto o quanto meno a modificarlo per assicurare il pieno rispetto degli obblighi internazionali e dei diritti umani. Lo ha osservato anche l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, che il 16 febbraio ha rivolto un analogo appello al Governo, denunciando che più persone in difficoltà soffriranno e saranno a rischio più vite in assenza di un aiuto tempestivo, se questa legge verrà approvata e, ancora, che anche vittime di tortura, violenza sessuale e altre violazioni dei diritti umani saranno costrette a ulteriori ritardi nell'accesso a cure mediche e riabilitazioni adeguate. Questo è il quadro, colleghi e colleghe, ed è per questo che come Partito Democratico abbiamo avuto e manteniamo una posizione di ferma ostilità e contrarietà questo provvedimento, chiedendone fin da subito il ritiro. Un'altra delle aberranti conseguenze di questo provvedimento è la norma che impone all'equipaggio delle imbarcazioni che abbiano effettuato le operazioni di soccorso di avviare tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, e, in caso di interesse, a raccogliere dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità, ponendola addirittura come condizione di legittimità dell'ingresso e del transito nelle acque territoriali. Una norma semplicemente sbagliata, che viola il diritto dell'Unione europea e affida compiti delicatissimi a persone non formate per svolgerli, mettendo così a rischio l'effettività del diritto di asilo. Si tratta di una norma che ignora due fondamentali disposizioni, per esempio, della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e, in particolare, gli articoli 60 e 61. L'articolo 61 dispone il divieto di respingimento delle donne vittime di violenza; l'articolo 60 obbliga gli Stati firmatari a sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di concessione dello *status* di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale. Queste norme andrebbero rispettate nel momento in cui si avviano le procedure finalizzate alla richiesta di protezione internazionale. Il provvedimento in esame semplicemente lo impedirà. Come se non bastasse, vi è un ulteriore profilo grave e preoccupante del provvedimento, il fatto cioè che le restrizioni che esso pone non violano soltanto gli inderogabili obblighi internazionali in materia di soccorso in mare, ma aggravano in maniera intollerabile le diverse situazioni di vulnerabilità che le persone migranti già si trovano a vivere. Questo è il caso soprattutto di minori e di donne vittime di violenza, donne che fuggono dai loro Paesi di origine a causa di situazioni di grave dolore e di grave sofferenza legate a guerre, situazioni politiche, economiche, ambientali, che colpiscono sempre di più le donne in modo diverso e in maniera sempre più dolorosa, intrecciandosi con squilibri, evidentemente di genere, già esistenti o con vere e proprie situazioni di disuguaglianza strutturale e violenza sistemica nei confronti delle donne. Le donne fuggono da violenze ambientali e culturali, quando non familiari, e anche dai rischi di tratta. Queste donne molto spesso nel loro stesso viaggio - ricordiamolo - sono vittime di ulteriori violenze, anche sessuali. Le donne sfuggono insomma alla categoria del migrante economico e del migrante politico, e per questo è necessario

protezione garantito alle mamme. Noi troviamo davvero assurdo tutto questo. Il diritto all'immigrazione non può rimanere insensibile alle specificità personali, non può rimanere cieco rispetto alla condizione di vita e alla peculiare condizione di vulnerabilità delle donne, in modo particolare di quelle migranti. Le donne, come ogni persona migrante, devono poter raggiungere sempre il porto più vicino al luogo di soccorso in condizioni di assoluta sicurezza, e al loro arrivo devono trovare ad accoglierle personale adeguatamente formato soprattutto al contrasto della violenza maschile. Penso in modo particolare a tutti i centri antiviolenza che sono oggi presenti sul nostro territorio nazionale e che fanno già fatica molto spesso a essere presenti nei porti di sbarco. Ecco, di questa specificità e di questa differenza lo ripeto - abbiamo il dovere e l'onere di prenderci cura, perché provvedimenti disumani e contrari a elementari principi di civiltà, come questo provvedimento in conversione, colpiscono in modo duro ogni persona, ma è evidente - ne possiamo essere certi - che si abbattono ancora di più su persone già vulnerabili, in modo particolare sulle donne vittime di violenza. Rispetto a tutto questo credo che sia assurdo tacere.

faccio appello a lei e alla sua sensibilità per rappresentarle un problema che per noi è molto importante.

Signor Presidente, prima di entrare nel merito del mio intervento in discussione generale, mi associo alle parole della collega Zampa, perché anch'io faccio parte della 10a Commissione,

consideriamo questo decreto davvero miope, incostituzionale e disumano. Il Governo dimostra tutta l'incapacità di affrontare il grande tema dell'immigrazione

quindi togliere qualsiasi nota retorica o ideologica, perché serve una discussione seria sul tema. È un problema che c'è e ci sarà, perché il tema ha una dimensione globale, internazionale, dalla crisi climatica alla crisi economica, dalla crisi sociale alla crisi demografica che svuota certamente il nostro contesto italiano ed europeo, ma - come sapete bene - questo problema è esploso nel continente africano. Allora, non basta un decreto-legge e non basta soprattutto questo decreto. Non basta perché il compito della politica è un altro. Il compito delle istituzioni istituzioni è governare i processi storici, indirizzarli in una direzione di umanità, di sviluppo e di benessere per le donne e gli uomini che abitano in questo pianeta. Questo è lo sviluppo che abbiamo a cuore: in sostanza è il rispetto della nostra Costituzione, il riconoscimento di quei diritti inviolabili della persona, riconosciuti anche a livello internazionale. C'è quindi un grande tema di gestione globale. Ebbene, come si fa a far fronte a un tema così grande e complesso se non parliamo in Europa di questi temi?

immigrati che chiedevano asilo noi abbiamo litigato con la Francia, che in quel momento concludeva la Presidenza dell'Unione europea, e sotto quella Presidenza il 10 giugno a Lussemburgo firmava un patto di solidarietà, che non è stato firmato dalla Polonia e dall'Ungheria, cioè i Paesi con cui voi vi confrontate è il motivo per cui non è stato firmato. Secondo elemento: si deve gestire la questione della sicurezza e della presa in carico di chi oggi è nei nostri mari e, anche qui, invece di fare un ragionamento complessivo partendo dal Governo Gentiloni e da quello che aveva fatto il ministro Minniti,

perché bisogna trovare un alibi; bisogna che troviate il vostro nemico immaginario, cioè le navi ONG *(Applausi)*, quelle che per voi sono responsabili di una vera e propria invasione, un nemico a cui addossare tutte le responsabilità, invece di affrontare seriamente il problema. Allora, da un lato si sposta la responsabilità sui soggetti sbagliati, dall'altro si affronta la questione con una soluzione impraticabile, inefficace e anche incostituzionale. Il decreto ONG non solo è contestabile nel merito per la sua inefficacia, ma è anche non accettabile nemmeno nella forma, poiché solleva numerosi e palesi dubbi di incostituzionalità, com'è stato ben evidenziato da altri colleghi. La questione non è soltanto formale: qui siamo di fronte a una norma disumana, una norma che dilata oltre ogni logica il concetto di porto sicuro, che costringe ad allungare di giorni il viaggio delle navi che hanno a bordo esseri umani - collega - e non le crociere. crociere. Parliamo di questo: sappiamo di tutte le persone che sono morte, che non ci sono più e dovremmo ricordarle, anche durante la discussione generale di questo decreto-legge. Affrontare il tema con serietà significa provare a riformare il sistema di accoglienza e di integrazione; depotenziare quei decreti-legge sicurezza, quei provvedimenti vergogna, a cominciare per esempio dall'istituzione di un'autorità indipendente per l'immigrazione, che permetta di gestire separatamente il fenomeno della migrazione economica da quella derivante dalle guerre, dalle violazioni dei diritti umani e da altre emergenze umanitarie. Insomma, non si affronta un tema così importante in maniera esclusivamente emergenziale. Bisogna rivedere il sistema dei rimpatri, che ad oggi non è funzionante e allo stesso tempo risulta essere anche molto costoso. Affrontare il tema con serietà significa, ad esempio, codificare in un nuovo testo organico tutte le norme relative all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza. Significa armonizzare la legislazione a norme costituzionali, internazionali ed europee. Ma significa anche rafforzare gli sportelli unici e le ambasciate italiane nei Paesi di partenza,

noi abbiamo cercato, come terzo polo, anche nell'Aula della Camera di parlare di questo, perché abbiamo le idee molto chiare: vogliamo parlare di norme che siano davvero attuabili ed efficaci. Vi chiediamo quindi di convincere,

un grande Paese come l'Italia - primo per volontariato, per solidarietà, per accoglienza, per ospitalità - a parlare bene di quello che stiamo facendo e che vorremmo fare. Per favore, siete ancora in tempo. Dovevo dare una risposta alle senatrici Zampa e Sbrollini. L'articolo 29, comma 8, del Regolamento prevede che i Presidenti possano convocare le Commissioni qualora non ci siano votazioni in Aula. Di conseguenza, la convocazione è regolare. Come da vostra richiesta, lo abbiamo chiesto al Presidente della Commissione e la stessa è stata riconvocata al termine della discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Ternullo.

La prima legge organica sul tema, la cosiddetta legge Martelli, è del 1990: essa ha posto le basi per l'accoglienza e l'integrazione degli immigrati in Italia, segnando anche un confine tra immigrazione legale e illegale. Per anni l'immigrazione è stata altresì regolata dai cosiddetti decreti flussi, che avevano l'obiettivo condivisibile di far incontrare la domanda di lavoro con l'offerta che veniva dalle imprese, soprattutto riferita ai lavori stagionali. Poi le cosiddette primavere arabe, che avrebbero dovuto accompagnare la democrazia, hanno portato negli ultimi anni a nuovi flussi di immigrati non regolamentati, che oggi è difficile controllare. Il provvedimento in esame tenta di porre rimedio alle attività delle navi delle organizzazioni non governative, che spesso risultano essere fattore attrattivo per i mercanti di migranti. Regolamentando e limitando il dinamismo in mare nel Mediterraneo, ci si attende un numero minore di arrivi sulle nostre coste, ma gli arrivi ormai avvengono anche con i cosiddetti barchini e in maniera autonoma, anche dalla Tunisia, soprattutto sulle coste della nostra vicinissima Sicilia. Le norme in esame, che valutiamo positivamente, non hanno visto diminuire i flussi negli ultimi due mesi di quest'anno, posto che il decreto è del 2 gennaio, e hanno evidenziato che questa non è la soluzione definitiva. Più di 12.000 arrivi per mare a gennaio e febbraio 2023 rispetto ai 4.700 nello stesso periodo del 2022: sono numeri più alti perfino di quelli dello stesso periodo del 2018, e cioè prima dei cosiddetti decreti Salvini. Certamente nel periodo in cui Salvini è stato Ministro dell'interno i numeri degli arrivi diminuirono sensibilmente: ovviamente, parlano i dati ufficiali. Così come gli arrivi sono tornati a crescere dopo che il Governo Conte 2 ha depotenziato i decreti che portano il nome del *leader* della Lega. Buona parte dei flussi che proviene dal Mediterraneo proviene ancora dalla Libia, cioè da uno Stato dove è stata creata un'instabilità politica che ormai dura dal 2011; ma non solo dalla Libia, anche da altre sponde mediterranee. Con i due Governi che controllano i territori di uno stesso Stato, la Tripolitania e la Cirenaica, e con la difficoltà di trovare degli interlocutori credibili con cui dialogare, certamente tutto si fa più difficile. Quei bombardamenti e il rovesciamento della guida di Gheddafi hanno vanificato un lavoro diplomatico enorme, voluto e tessuto personalmente dal presidente Berlusconi con grande capacità e lungimiranza politica. Così come dal presidente Berlusconi venne la straordinaria intuizione di chiamare al vertice di Pratica di Mare del 2002 la Russia e farla sedere al tavolo con i principali Paesi del mondo, inclusi quelli dell'Alleanza atlantica. Putin che stringe la mano di Bush *junior* è una immagine indimenticabile, un capolavoro diplomatico dovuto a un uomo capace e pragmatico come l'allora Capo del Governo e *leader* di Forza Italia. invece, l'attuale Presidente americano e quello russo - sempre lo stesso di Pratica di Mare, Vladimir Putin - non solo non si parlano, ma si confrontano militarmente sul territorio ucraino, dopo essersi confrontati militarmente in altri territori a Oriente, come Siria, Afghanistan, Yemen e altri. Questa instabilità geopolitica che ancora si registra in Oriente ha fatto aumentare le fughe dal proprio Paese di origine di migliaia di profughi, che spesso sono anche migranti economici. Le loro storie sono molto simili e il loro tragitto finisce per raggiungere il Mediterraneo e poi l'Italia. Cosa bisogna fare per fermare gli arrivi? Bisogna tornare a fare accordi seri con chiunque abbia il controllo dei territori dove vivono i migranti e fare in modo che sia più attraente restare che migrare. Oggi la diplomazia sembra essere diventata incapace di intessere accordi di pace e di creare benessere per i popoli. Un altro dato che deve guidare il nostro ragionamento è l'attribuzione del permesso di soggiorno, posto che i dati del Viminale ci dicono che il permesso viene negato a sei richiedenti ogni quattro. Fare arrivare nuovi immigrati significa creare nuove sacche di clandestinità, perché chi non ha un permesso di soggiorno rimane comunque in Italia in modo illegale. Quindi, chi ha titolo dovrebbe arrivare in Italia attraverso appositi corridoi umanitari, senza rischiare la propria vita. Ovviamente, il nostro pensiero non può non andare alle migliaia di morti inghiottiti dalle onde del mare. Dopo gli arrivi degli ultimi anni, il numero dei clandestini in Italia è stimato in più di 600.000 unità, cioè la popolazione di un'intera città come Palermo, che, senza alcun titolo, vediamo sparsa sull'intero territorio italiano.

il disagio di questi stranieri che vivono alle periferie della città spesso si somma a quello degli abitanti, ponendoli di fronte al degrado sempre più ampio delle periferie. I costi che paga tutta la nostra società sono enormi. I costi che paga la mia Sicilia sono giganteschi, sia perché gli approdi sono continui sia perché la gestione di flussi così ingenti comporta problemi quotidiani per i miei stessi concittadini. In termini di bilancio dello Stato, parliamo di oltre 2 miliardi appostati per il 2023 per affrontare il fenomeno dell'immigrazione e dell'accoglienza degli stranieri che giungono in Italia. Un dato, però, va evidenziato: nei Paesi africani in cui sono cresciuti gli investimenti esteri, dove sono state create infrastrutture moderne, sono aumentati gli insediamenti produttivi e i posti di lavoro; da quei Paesi gli esodi sono diminuiti. Il più grande investitore in Africa negli ultimi quindici anni è la Cina, arrivata a più di 250 miliardi di euro di scambi commerciali nell'ultimo anno. Un analogo livello di investimenti dovrebbe essere messo in campo dall'Unione europea, che, però, appare priva di una direzione concreta in politica estera. estera. La questione migranti dell'Africa ma anche dell'Asia va affrontata soprattutto a livello europeo. L'Europa, quindi, deve farsi carico del problema degli arrivi, ma soprattutto deve farsi carico di firmare accordi che evitino le partenze. La gestione degli arrivi e dei permessi deve essere distribuita omogeneamente su tutti i Paesi europei; allora, anche le norme di questo decreto-legge diventerebbero meno cogenti in quanto crollerebbe il numero reale degli arrivi in Italia. Italia. Soprattutto va messo in campo un piano europeo per cambiare il paradigma che ha visto i Paesi europei come colonizzatori e farli diventare finalmente Paesi investitori. *(Applausi)*.

vorrei partire da una considerazione che ho condiviso oggi pomeriggio anche con i colleghi della Commissione affari costituzionali, che è un rilievo che faccio principalmente sotto il profilo giuridico, che riguarda le tecniche di normazione che sono state adottate dal Governo per questo decreto-legge. Sapete che quando si concepisce una norma giuridica, questa va a inserirsi nel contesto di un quadro normativo complessivo; va a inserirsi in un ordinamento giuridico e deve necessariamente tenere conto di tutto il complesso di norme che è non soltanto italiano, ma anche internazionale. Parliamo per il momento di ciò che ci impongono norme che sono alla base della nostra Repubblica italiana. Parliamo delle norme costituzionali; ne sono state citate a tante dai colleghi, ma io vorrei focalizzare l'attenzione su una di queste che ritengo fondamentale e prioritaria: l'articolo 2 della nostra Costituzione. È un articolo che vuole difendere i diritti umani: la Repubblica italiana difende e garantisce i diritti umani, e - Presidente - il primo dei diritti umani è il diritto alla vita e all'incolumità personale; diritto alla vita che questo provvedimento mette in discussione perché va a inserire un sistema di iperburocratizzazione nella gestione di un momento di emergenza. Signor Presidente, non basta che una norma si inserisca in un contesto normativo: una norma giuridica deve inserirsi anche in un contesto sociale, all'interno di un contesto culturale, e io sono convinto che non risiede nella cultura italiana e che non fa parte del DNA degli italiani una cultura dell'intolleranza, del disprezzo. Anche quando abbiamo studiato le fonti del diritto, Presidente, la prima fonte del diritto non è certo il diritto naturale che prevede la prevaricazione del più forte sul più debole, e non esiste neppure una fonte di diritto divino che stabilisce e ci detta quali sono le regole. Pensiamoci bene: quando l'uomo per la prima volta ha iniziato a scrivere le sue regole ha attinto innanzitutto al suo mondo interno, alla sensibilità. Esiste prima di tutto un sentimento di giustizia, quel sentimento che risiede nelle corde più profonde della nostra anima; quel sentimento che consente anche a un bambino di capire se un fatto è giusto o meno.

Qualunque problema può avere una soluzione, ma ciò che è fondamentale è dare innanzitutto una risposta umana, una risposta degna di una società civile.

però, su un secondo elemento, che non è semplicemente formale, Presidente, ma travalica la forma ed è alle basi della nostra democrazia: la scelta della decretazione d'urgenza. È vero: si torna spesso su questo problema, ma in questo caso abbiamo un problema costituzionale, ovvero l'articolo 77 vieta al Governo di adottare decreti che abbiano valore di legge. Sono scorciatoie normative che la Costituzione non consente e sono consentite soltanto se c'è una delega delle Camere - in questo caso non c'è - oppure quando ci sono casi di straordinaria necessità e urgenza. qual è la necessità e quale l'urgenza di affrontare un tema che esiste da anni, senza che vi sia alcun tipo di elemento di novità per giustificare la compressione dei diritti democratici e di un confronto democratico parlamentare. Probabilmente pensiamo che sia soltanto un problema di forma, perché tutto sommato siamo qui anche a discutere, nonostante si tratti di un decreto. Ma chi ben conosce quali sono le norme e le procedure in ambito parlamentare sa bene che un decreto pone dei limiti fondamentali, che sono limiti temporali, ed ecco che il dibattito viene precluso. Presidente, di fatto il Senato in questo provvedimento non può mettere bocca. Ne possiamo parlare, ma non abbiamo alcuna possibilità di intervenire come richiederebbe, invece, un provvedimento così delicato che riguarda il tema dell'immigrazione. Non è un problema secondario, Presidente, e non coinvolge soltanto un ramo del Parlamento, perché la scelta della normazione dell'emergenza ha precluso anche all'altro ramo del Parlamento di poter fare un completo lavoro emendativo. ora nel merito del provvedimento, anche se quella che ho appena menzionato è una questione non di forma, ma di rispetto della democrazia e della popolazione che su questo tema può mostrarsi giustamente divisa e che va degnamente rappresentata. Con questo provvedimento, stiamo inserendo un sistema di iperburocratizzazione del salvataggio di emergenza. Stiamo inserendo una burocrazia che rischia di uccidere. Ricorderete Rigopiano e quanto allora la burocrazia è riuscita a rallentare la gestione di un'emergenza, quando strumenti fondamentali di monitoraggio sono rimasti bloccati per ore alla dogana perché non bastavano le telefonate ma era necessario un fax. Dobbiamo sapere che ogni volta che noi associamo la parola burocrazia all'emergenza stiamo commettendo un errore imperdonabile di cui dobbiamo assumerci la piena responsabilità. C'è un altro elemento che riguarda la tecnica normativa, ma che non può essere sottovalutato: avrete notato che ci sono state tantissime diverse interpretazioni che sono nate da questa norma, con la preoccupazione - da un lato - che ci fosse il divieto del doppio salvataggio, che poi qualcuno ha messo in discussione. Noi accusiamo spesso il popolo italiano di essere litigioso, di riempire i tribunali di contenzioso, ma nella vita faccio l'avvocato e so che non è vero; so che noi ci ostiniamo e continuiamo a produrre normative che non sono chiare, che lasciano troppo spazio all'interpretazione e minano quell'esigenza fondamentale di certezza del diritto. Non è colpa degli italiani: è colpa di un legislatore che è poco attento a dettare norme che, se da un lato devono essere generali e astratte, dall'altro non possono generare incertezze e divergenze che creano problemi a chi poi nel concreto le deve applicare. Un problema di questa portata andava affrontato dal Parlamento con i tempi necessari, richiesti da una legge ordinaria. Attenzione, vorrei usare un'immagine freudiana: quando abbiamo un fiume in piena, dobbiamo non interrogarci sulla potenza delle sue acque, ma chiederci per quale motivo ci sono ostacoli, per quale motivo ci sono degli argini che l'hanno ingabbiato. Noi stiamo sempre pensando di risolvere il problema una volta che esso ci sta precipitando addosso. Cosa ha proposto sempre il MoVimento 5 Stelle per risolvere il problema dell'immigrazione? In primo luogo, ha proposto la cooperazione internazionale che non va depotenziata, ma deve essere incrementata, una gestione europea dell'immigrazione. Vorrei raccontarvi una piccola storia - spero di averne il tempo - che riguarda un esempio che va attribuito purtroppo non allo Stato, ma a un'associazione privata, dove la cooperazione internazionale aveva portato i suoi frutti, purtroppo successivamente distrutti da uno scellerato intervento militare. Parlo di un piccolo villaggio dell'Etiopia, di un piccolo villaggio dell'Etiopia, dove un'associazione di volontari ha realizzato un ospedale e una scuola. Bene, quel piccolo villaggio, nell'arco di poco tempo, è diventato una cittadina di 70.000 abitanti,

di sopravvivenza, di avere un ospedale e di non morire per la puntura di una zanzara; avere la possibilità di dare un futuro ai propri figli grazie alla possibilità di ricevere un'istruzione. recuperare il senso delle cose e cominciare a pensare che i problemi vanno sistemati alla loro radice e che dobbiamo arrivare all'inizio ai problemi. Ma soprattutto dobbiamo recuperare la capacità di legiferare in modo umano, recuperare la dimensione umana del sistema normativo.

il decreto flussi migratori rappresenta un primo passo verso il riordino della gestione migratoria. Parlo di riordino perché già un po' di ordine con Matteo Salvini, Ministro dell'interno, lo avevamo messo, così come inteso da questo Governo. Basta guardare i dati sull'immigrazione nel nostro Paese per vedere in modo molto chiaro che avevamo ragione. Quando eravamo al Governo, ed erano in vigore le regole dei decreti sicurezza di Salvini, nel 2019 gli sbarchi erano 11.000; con le nuove regole e, poi, nel corso del 2020, sono stati 33.000; nel 2021 sono stati 63.000; nel 2022 siamo addirittura arrivati a superare i 100.000; un incremento quasi del 60 per cento. Sono numeri che sono ritornati a essere esorbitanti e preoccupanti. Modificare quei decreti ha comportato un aumento incontrollato dell'immigrazione clandestina nel nostro Paese. Gli italiani però questo lo hanno capito e hanno capito che la linea politica della sinistra è quella dell'invasione incontrollata, e questo è uno dei motivi per cui abbiamo vinto le elezioni. Questo provvedimento che riguarda nello specifico il tema del soccorso in mare, quindi le ONG, rappresenta un primo tassello nella giusta direzione da parte di un Governo che si è rapidamente attivato per tornare a controllare i flussi migratori.

che, con chiaro disinteresse nei confronti delle attuali leggi, e quindi delle leggi italiane, avrebbero intensificato la loro attività in barba alle leggi per portare ancora più immigrati in Italia? È una chiara sfida ideologica a quello che invece rappresenta un problema serio, che richiede un approccio altrettanto serio e pragmatico. Se le ONG dichiarano apertamente che vogliono violare la legge italiana e se 65 parlamentari stranieri tentano di dire al Parlamento italiano cosa fare, non siamo certo noi a fare una battaglia politica come qualcuno ci accusa sono proprio loro a fare una battaglia politica contro il Governo e soprattutto contro l'interesse della nostra Nazione e degli italiani. La nostra è una proposta concreta per la risoluzione del problema. La parte che trattiamo oggi riguarda, quindi, quella parte del decreto Lamorgese sullo stravolgimento delle norme sul divieto di ingresso, di transito e di sosta nelle acque territoriali italiane, la riduzione delle multe, la cancellazione del blocco amministrativo delle navi, rendendo possibili multe e sanzioni amministrative soltanto dopo un procedimento penale. Ciò significa di fatto - come tutti noi abbiamo potuto appurare - renderle assolutamente inefficaci. Oggi le azioni di questo Governo sono in perfetta conformità di pensiero con il decreto di cui stiamo trattando e con le ripetute critiche che apertamente abbiamo sempre espresso nei confronti della normativa dell'ex ministro Lamorgese. Quello di oggi è un intervento necessario, finalizzato al riordino di un ambito che è stato lasciato al caso, in un clima che sembra ormai un *far west* e che palesa una netta soggezione nei confronti dell'Europa. L'Italia e il nostro Mezzogiorno non possono e non devono diventare - come vorrebbe qualcuno - un unico campo di accoglienza senza controllo. È evidente che il problema esiste e va affrontato nel modo giusto. Entrando nel merito delle modifiche, questo decreto fissa norme di sicurezza per chi fa attività di salvataggio, ma soprattutto per chi viene salvato. Esso prevede la conformità della nave alle certificazioni e alla documentazione richieste dallo Stato di bandiera e prevede che la richiesta di assegnazione del porto sicuro debba avvenire immediatamente dopo il salvataggio. Prevede inoltre la collaborazione con le autorità nazionali per fornire informazioni sulle operazioni di salvataggio; viene richiesto di non creare situazioni di pericolo e di arrivare tempestivamente al porto assegnato. Oltretutto il comandante ha l'obbligo di rendere un'informativa al migrante recuperato sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale. Questo è importante a fronte delle regole del Trattato di Dublino. Sappiamo bene che chi oggi arriva in Italia come richiedente asilo deve restare qui e che l'Italia in questo caso deve farsi carico di esperire tutte le pratiche. È quindi evidente che c'è chi ha interesse ad affrontare il tema dell'immigrazione assecondando l'illegalità. Occorre invece difendere i confini nazionali e creare flussi di immigrazione legali, ponendo regole serie, come quelle che stiamo affrontando oggi in quest'Aula. Questa maggioranza e questo Esecutivo continueranno senza sosta la battaglia contro l'immigrazione clandestina. Chi pensa oggi di opporsi per puro idealismo, pensando di fare un torto a questo Governo, sta di fatto facendo un grave danno agli italiani e al nostro Paese. Questo Governo ha voluto dare da subito dei segnali concreti anche all'amministrazione di Lampedusa, che ha sempre avuto contatti contatti continui e costanti direttamente con il ministro Salvini. Quando si parla di Lampedusa, è qualcosa che non ha colore politico, ma che trasversalmente dovrebbe interessare e dovrebbe stare a cuore a tutti. Ma purtroppo è chiaro che non è così. Nei pochi mesi di Governo, con il decreto milleproroghe abbiamo già previsto un contributo straordinario di due milioni e mezzo di euro in considerazione degli sbarchi degli immigrati. Abbiamo previsto inoltre il ripristino della norma sulla moratoria fiscale e, quindi, la proroga dei tributi già introdotta da un Governo di centrodestra nel 2011, poi abrogata un paio di anni fa da un Governo di centrosinistra. ancora la norma per consentire al Comune di Lampedusa di assumere personale a tempo determinato in deroga alle norme sui bilanci di previsione. Si tratta di provvedimenti fortemente voluti dalla Lega, che ha sempre confermato la sua grande attenzione per l'isola. Oggi vogliamo ringraziare tutto il Governo Meloni per quello che fin qui è stato fatto e per questo provvedimento il ministro dell'interno Piantedosi e il nostro sottosegretario Nicola Molteni perché approcciarsi a un sistema di immigrazione corretto significa tutelare la sicurezza dei cittadini. E questo è prioritario nell'interesse non soltanto della Sicilia, ma dell'Italia e dell'Europa tutta.

Abbiamo opinioni molto diverse in materia, ma soprattutto penso che possiamo partire cercando di evitare di dire le cose che sono state già dette in questa sede, cioè che c'è una sinistra che vuole l'immigrazione clandestina e che vuole favorire l'invasione. Usciamo da qui, per favore. Non stiamo facendo comizi elettorali e non siamo alla ricerca di voti. Le campagne elettorali sono finite e siamo tutti impegnati per avere un'immigrazione regolare, dignitosa, seria. Siamo impegnati a far la guerra ai trafficanti di armi e ad avere finalmente una politica dell'immigrazione che sia degna di un grande Paese occidentale. Fa un po' tristezza sentire in quest'Aula ancora ripetere che noi siamo a favore dell'invasione dei nostri quartieri, che vogliamo creare insicurezza. Ho sentito parole non credere alle mie orecchie, sinceramente, signor Sottosegretario. Credo che anche lei, che comunque è una persona ragionevole e seria, possa avere qualche dubbio. Certe parole possono essere pronunciate durante la festa della birra di qualche partito, ma non in un'Aula parlamentare. Per dimostrarle che questo mio intervento vuole essere un contributo e non vogliamo essere arroganti sull'argomento, che sappiamo quanto sia complesso, dico che apprezziamo il suo sforzo e quello del ministro Piantedosi, perché crediamo siate seriamente impegnati. Mi consenta, è stato detto - sulla decretazione d'urgenza usata inutilmente, e le abbiamo avute con i nostri Governi. In questo caso crediamo che voi ne abbiate abusato in maniera nel senso che una decretazione d'urgenza su un argomento che non è in alcun caso e per nessun motivo attribuibile a situazioni di emergenza è veramente molto oltre quello che persino noi abbiamo osato fare. Abbiamo colpe comuni

e arrivasse una richiesta di soccorso, pensate che le decine e centinaia di navi mercantili che transitano in Italia non dovrebbero salvare quei migranti? Lo stanno già facendo. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma di cosa state parlando? Che cosa c'entrano le ONG? Sapete benissimo che la gran parte dei migranti arriverebbe comunque sulle navi mercantili che sono vincolate a leggi internazionali, non a leggi locali, Presidente. Spero che il Sottosegretario riesca ad ascoltare con l'altro orecchio.

detto da tutti i Capi di Governo che l'immigrazione è un problema europeo. Certamente sarebbe necessario che anche le altre Nazioni, come la nostra, condividessero perlomeno la revisione del Regolamento di Dublino, cioè l'onere che arriva sulle nostre coste; cosa che abbiamo ripetutamente chiesto con tutti i Governi dal 2013 in poi e che ci è stata

una cosa che, a differenza di quello che ha detto il collega Romeo, non c'entra proprio un bel niente con il codice di condotta delle ONG. Ricordo benissimo quel codice di condotta, perché fu impostato dalla dalla Guardia costiera italiana e fu assunto dal ministro Minniti che lo fece poi firmare alle ONG. Quel codice di condotta stabiliva delle regole molto chiare, molto semplici, pattizie: il fatto che non bisognasse fare trasbordo di migranti; il fatto che non bisognasse mai spegnere gli apparati radio; il fatto il fatto che bisognasse avvertire e coordinarsi continuamente con l'autorità preposta per il centro di coordinamento e soccorso. Inoltre mi chiedo: se bastava il codice di condotta, perché abbiamo fatto un decreto-legge?

questo in realtà non è un decreto-legge flussi contro l'immigrazione clandestina; non è un provvedimento per governare i flussi regolari; non è un provvedimento per disciplinare meglio i salvataggi in mare, che sono già disciplinati dalle Convenzioni del 1974 e del 1979, con le revisioni SAR e SOLAS del 2004. non c'entra proprio niente con tutto ciò. Si tratta semplicemente di un modo per continuare a dichiarare guerra alle ONG. Sapete quali sono i nomi delle ONG che ci fanno tanta paura? Medici senza frontiere, Emergency: questi sono i nemici della Repubblica. *(Applausi)*. Oggi scopriamo che l'emergenza del Paese è combattere contro Emergency e Medici senza frontiere,

giustamente obbligate, perché è un segno di civiltà e il Mediterraneo dovrebbe essere un mare di civiltà e non di morte, un mare dove si riafferma l'indiscutibile sacralità della vita umana. *(Applausi)*. Ogni vita che perdiamo è una sconfitta: sono sicuro che condividiate questo e non mi permetterei mai di dire che fate questa cosa per affogare più gente nel Mediterraneo. Non mi permetterei mai, perché penso che siate animati da buoni propositi; purtroppo non siete animati da buona sapienza amministrativa, perché tutta questa roba non c'entra proprio un bel niente. La guerra alle ONG - me lo si permetta - è la guerra ai migranti. Li

Avete mai visto scendere i bambini dalle navi delle ONG? Avete mai visto le facce delle donne e degli uomini che sono stati settimane in mare o stuprati nei campi della Libia? *(Applausi)*. Li avete mai visti in faccia per dire che sono minicrociere? Ma è una vergogna! Non si può sentire che sono minicrociere. *(Applausi)*. Siamo indignati per questo. Non penso che vogliate fare del male a nessuno, ma non potete dire cose del genere. che si fanno centinaia di chilometri perché ci si diverte nel Mediterraneo. Ma li avete mai visti negli occhi, magri, impauriti, che tentano di suicidarsi dalle navi? navi? Questo è quello che succede. Dopo discutiamo su come fare meglio, ma non diciamo stupidaggini e non facciamo provvedimenti impegnando lo Stato e il Governo, facendo la guerra a Emergency e a dei migranti impauriti che scappano dalla guerra e dalla fame. Presidente, per questo motivo siamo delusi anche oggi, perché speravamo che il Governo cominciasse finalmente a fare meglio le cose che anche noi magari potevamo fare molto meglio. Invece, ancora una volta, siamo qui a vedere sventolare una bandiera inutile e dannosa per il nostro Paese.

onorevoli colleghi e colleghe, componenti del Governo, ritengo doveroso prendere la parola quest'oggi quest'oggi per spiegare i motivi che spingono Fratelli d'Italia ad essere convintamente a sostegno di questo decreto, ma anche per rispedire al mittente alcune accuse gravi, molto gravi, che sono state fatte a questa parte politica.

discussione, ci siamo sentiti dire che noi saremmo quelli che vogliono impedire i soccorsi, quelli che vogliono ledere il diritto alla vita

nostro esame è esattamente il contrario di quello che continuate a gridare nelle piazze. All'interno di questo decreto ci sono delle norme che cercano di tutelare e difendere i diritti dei migranti e se qualcuno prima di parlare avesse il buon gusto di leggerlo scevro da qualsiasi condizionamento ideologico, si accorgerebbe che al suo interno ci sono semplicemente delle norme di buon senso che cercherò di spiegare. Riteniamo che sia una norma di buon senso quella che prevede che il porto di sbarco debba essere raggiunto senza ritardo, dopo che sia stato effettuato il salvataggio. mi spiegate come fate ad essere contrari a questa norma? I soccorsi, da che mondo è mondo, sono caratterizzati dalla tempestività e dalla velocità dell'intervento. Voi trovate umano che persone salvate in mare, dopo giorni di navigazione su imbarcazioni di fortuna, una volta sulle navi siano costrette a rimanervi ore, se non giorni, fino a quando non venga raggiunto il pieno carico? Questa è una clausola che francamente ho trovato soltanto nei *tour operator*, laddove è scritto: attenzione: il viaggio si farà solo se verrà raggiunto il massimo dei partecipanti. Le operazioni di soccorso non sono sono viaggi organizzati, vero? *(Applausi)*. Siamo d'accordo almeno su questo? Allora, lasciamoli portare rapidamente a terra i migranti, il che non esclude - com'è stato anche chiarito dall'intervento del senatore Scurria - che sia possibile fare altri salvataggi durante la rotta che conduce al porto assegnato. Un'altra norma di buon senso è quella che prevede che nelle operazioni di soccorso ci sia un raccordo con le autorità italiane. Anche questa mi sembra una cosa scontata, si verifica in qualsiasi operazione di soccorso: un coordinamento tra tutti gli attori che intervengono nelle attività di soccorso. A proposito di autorità, consentitemi di ringraziare tutti gli uomini e tutte le donne della Guardia costiera, della Guardia di finanza, della Marina militare che, con le loro imbarcazioni, salvano

modo è una norma di buon senso la previsione per cui la richiesta di assegnazione del porto di sbarco da parte delle ONG avvenga nell'immediatezza del salvataggio e soprattutto che siano le autorità italiane a decidere dove effettuare lo sbarco e non le ONG. Anche questa è una scelta assolutamente giusta. Forse sfugge che ci sono dei centri di accoglienza, come per

negli stessi porti dove ci sono centri sovraffollati, andando a creare anche problemi di ordine pubblico. A questo

vi chiedo se queste previsioni sono contro o a tutela dei migranti, ma la risposta è una sola: tutte queste norme sono assolutamente di buon senso. Che si

perché i veri nemici dei migranti sono tutti coloro che fanno finta di non capire che dietro questo costante flusso c'è la criminalità organizzata, ci sono i trafficanti di vite umane! *(Applausi)*. È contro i migranti chi non vuole capire che per fermare le morti in mare bisogna fermare le partenze e per farlo bisogna affermare il principio che in Italia si entra solo regolarmente.

Noi, dunque, vogliamo accogliere i profughi e garantire loro la massima protezione e contestualmente vogliamo creare le condizioni di sviluppo sociale ed economico

Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire nella giornata di domani, anche alla luce degli emendamenti che sono stati appena presentati, per fare un'analisi più attenta degli stessi.

a nostro avviso, violazione di principi costituzionali e di norme inequivoche del diritto internazionale, chiediamo appunto, ai sensi dell'articolo 96, di non passare all'esame degli articoli, ma di rinviare il provvedimento in Commissione, in modo da poter svolgere in tale sede quel confronto, quella discussione, quell'approfondimento che non è stato possibile effettuare. prevede che questa richiesta possa essere messa in votazione dopo le repliche del Governo.

non si ritrovasse, fra pochi giorni, ad avere un testo di cui non potremo certo andare fieri. Ho sentito che il Governo ha dato un barlume di spiegazione, ma limitandosi a dire che si riserva di valutare gli emendamenti e di Ma la replica a ciò che abbiamo detto, la replica alle considerazioni che abbiamo fatto, la replica alla discussione generale che si è svolta,

fondati, così tanto difficili da controbattere, allora il Governo potrebbe dire che va alla ricerca di qualche ragione per provare a spiegare perché, ad esempio, si possa affrontare il tema dell'immigrazione ostacolando il lavoro delle ONG; o spiegare perché ad esempio si debba prevedere il divieto di soccorso multiplo. Ecco, se il Governo ha bisogno di trovare una qualche ragione per spiegare, a noi e al Paese, il perché di questo provvedimento, forse potrebbe prendere la parola e dire

visto che, come ha precisato il senatore Giorgis, si tratta di repliche. In italiano, si replica a qualcosa che si è ascoltato. Non c'entrano niente gli emendamenti, di cui parleremo domani. La replica è riferita agli interventi che abbiamo ascoltato in Aula

cui il dibattito che si è sviluppato, non solo nelle due Aule del Parlamento, ma anche abbondantemente sui *media* e nell'opinione pubblica del Paese, è a mio avviso maturo. Ripeto, secondo me, secondo me, le questioni sono state evidenziate con grande nettezza e mi sembrano molto chiare; le abbiamo enucleate dal punto di vista della conformità al diritto internazionale e alla nostra Costituzione, e abbiamo avuto elementi puntuativi su alcune questioni tecniche. Abbiamo sottolineato in molti modi quali sono gli ostacoli che vengono posti in capo a chi sta svolgendo un'attività di salvataggio in mare: elementi di aumentata burocrazia e accresciuta responsabilità,

per l'informazione dell'opinione pubblica del Paese, sarebbe utile poter apprendere direttamente dal sottosegretario Molteni come mai un salvataggio che avviene presso la Sicilia viene poi indirizzato verso il porto di La Spezia e perché le persone salvate a La Spezia vengono caricate su un autobus e portate a Foggia. Se ci fosse una logica in tutto questo, credo che l'immagine del Governo ovviamente ne beneficerebbe, ma ne beneficerebbe altresì anche la consapevolezza dell'intero Paese sulla visione e la strategia in relazione a un elemento così importante per la nostra opinione pubblica nazionale. Sarebbe utile anche comprendere, per esempio, quali siano le attività che si vogliono immaginare per migliorare l'efficacia del lavoro all'interno dell'Unione europea, dove, appunto, la vicinanza a Governi che tradizionalmente si oppongono alla ridistribuzione dei naufraghi creano un problema. tutta una serie di questioni - sorvolo sulle crociere di cui oggi abbiamo dovuto, purtroppo, sentir parlare - però, se almeno potessimo utilizzare anche il tempo che abbiamo a disposizione fino alle 20 per comprendere meglio quella che appare una strategia completamente erratica posta in essere dal Governo, inspiegabile al buon padre di famiglia rispetto al sano buonsenso, penso che questo farebbe bene al dibattito pubblico nazionale. Quindi, anche da parte nostra, l'invito al sottosegretario Molteni è di approfittare del tempo che abbiamo per illuminarci quanto a questa oscura strategia posta in essere dal Governo e quindi aiutare non soltanto il dibattito parlamentare nell'approvazione di questo importante decreto-legge, ma anche la consapevolezza del Paese rispetto a un tema che - ripeto - credo sia vicino al cuore di tutti gli italiani. *(Applausi)*.

del sottosegretario Molteni. Capisco che ci sia un po' di disorientamento in quest'Aula che per troppo tempo è stata abituata sempre al voto di fiducia e al fatto che il Parlamento non possa minimamente intervenire. di costituzionalità, si è messo in evidenza che il Parlamento assolutamente non viene mai chiamato a esprimersi e adesso addirittura il Governo dice

Signor Presidente, evidentemente ci deve essere un caso di omonimia, ci deve essere un altro Massimiliano Romeo che è stato al Governo per quasi tutta la scorsa legislatura.

la decisione di non apporre la fiducia su questo provvedimento e quindi di consentire il voto degli emendamenti, che peraltro non sono neanche eccessivamente numerosi (circa 168). Gli Gli emendamenti sono gli stessi che erano già stati depositati in Commissione, quindi anche dire che c'è una necessità per il Governo di analizzarli e di studiarli per capire di che cosa si tratta può andare bene per chi al di fuori non conosce lo svolgimento dei lavori e quello che è già successo, quindi è chiaro che per noi questa motivazione non è valida. Vorrei però sottolineare un'altra cosa, Presidente.

la discrezionalità che autorizza il Governo a decidere quando svolgere le repliche o meno? Inviterei il Governo a replicare, così si può andare avanti e procedere nei lavori come democraticamente è dovuto a questa Assemblea. Senatrice Maiorino, la questione è in questi termini: è pervenuta alla Presidenza una richiesta di non passaggio all'esame degli articoli ai sensi dell'articolo dell'articolo 96 del Regolamento, regolarmente sottoscritta e firmata, e il Governo, interpellato sulla replica, ha inteso dichiarare che intende svolgerla domani mattina, questo anche avendo apprezzato le circostanze, se la Presidenza interpreta correttamente,

l'argomento su cui ho chiesto la parola per un intervento di fine seduta forse avrebbe meritato un'altra collocazione, ma come Gruppo Partito Democratico, rappresentando la volontà di un largo numero di cittadini, noi abbiamo la necessità di sollevare la questione in maniera urgente. Mi riferisco al pestaggio squadrista avvenuto nel Comune di Firenze davanti al liceo «Michelangiolo» sabato scorso, di cui hanno riferito ampiamente i quotidiani locali e nazionali. Sono in corso indagini delle Forze dell'ordine e di altre autorità inquirenti. C'è una città, il capoluogo toscano, che è stata letteralmente scioccata da quanto è avvenuto, perché noi condanniamo sempre le violenze e ce ne dissociamo ogni qualvolta le vediamo avvenire e sempre quando riguardano la nostra parte e anche altre parti. Assolutamente non crediamo possibile che ci sia sottovalutazione, ambiguità e silenzio quando succedono cose come quelle che sono accadute sabato. C'è stata un'aggressione organizzata; sei persone che paiono, a giudicare dalle immagini, molto ben allenate nel ruolo di picchiatori, se la sono presa con degli studenti per ragioni su cui le Forze dell'ordine stanno indagando, ma lo hanno fatto in una maniera che ricorda tempi bui della nostra storia e che assolutamente non può essere accolta né con comprensione, né con mistificazioni, né soprattutto può essere accolta con il silenzio. con il silenzio. Ci sono in questo momento sei persone indagate, tre maggiorenni, tre minorenni, tre dalla procura della Repubblica ordinaria, tre dalla procura per i minori, per violenza privata aggravata e per manifestazione non autorizzata, tutti e sei appartenenti ad Azione studentesca. Voglio soffermarmi su un aspetto, altrimenti non si capisce Azione studentesca, nella città di Firenze, è un'organizzazione giovanile legata molto fortemente al partito di maggioranza relativa, a Fratelli d'Italia, fino al punto di avere la propria sede in Via Frusa 37, nello stesso stabile dove c'è una sede di Fratelli d'Italia e una di Casaggì. Ora noi non intendiamo minimamente estendere la responsabilità dell'aggressione al partito Fratelli d'Italia, anzi noi pensiamo che ci sia profondo imbarazzo e anche che ci sia la volontà di non riconoscersi assolutamente in queste gesta, anche se vengono da un'organizzazione vicina. Da giorni però chiediamo inutilmente alla Presidente del Consiglio, che di Azione studentesca è stata presidente nazionale nel 1996 e al ministro dell'interno Piantedosi *(Applausi)* di dire una parola una parola di condanna e di presa di distanza da questo pestaggio squadrista e fascista, che ha provocato ieri a Firenze una manifestazione con migliaia di studenti in corteo! Una parola! Una! Non è arrivata una parola e questo è molto grave perché noi, tutte le volte che una minaccia riguarda la Presidente del Consiglio, abbiamo senatori e deputati del Partito Democratico che fanno comunicati stampa per dissociarsi e io tutte le volte che avviene qualcosa che sa di violenza contro una carica dello Stato, dico che non va bene, prendo la parola e non mi permetto mai né il silenzio né l'ambiguità. Sono passate novantasei ore, quattro giorni da quel pestaggio, ci sono sei persone di Azione studentesca indagate. Azione studentesca è un'organizzazione vicinissima a Fratelli d'Italia e il Presidente del Consiglio di Fratelli d'Italia non può più tacere e il suo Ministro dell'interno deve venire in Parlamento a dire quali iniziative intenda intraprendere! A dire come intende reagire! Non possono avvenire le aggressioni davanti alle scuole, davanti ai licei, e tutto questo nel silenzio del Governo. E poi c'è anche un presidente di Regione, il presidente dell'Abruzzo Marsilio, che ha fatto il commento più geniale, dicendo che quella non è stata un'aggressione fascista, ma una rissa. Ha parificato le responsabilità. Il presidente Marsilio ha qualche difficoltà nella lettura dei video, oppure vede i video sbagliati oppure ha perso un'occasione per tacere.

ieri nella mia città, a Genova, un uomo di trentasette anni, un operaio di Ansaldo Energia, ha subito un gravissimo infortunio sul lavoro, che lo costringe in queste ore a lottare tra la vita e la morte all'ospedale San Martino di Genova. Istat raccontano che nel 2022 abbiamo avuto il 30 per cento di denunce in più per infortuni sul lavoro, e si parla di mille morti sul lavoro nel 2022. Io penso che questo problema vada affrontato in modo serio. Vorrei dire che il Gruppo MoVimento 5 Stelle è al fianco dei lavoratori di Ansaldo Energia, che questa mattina giustamente a Genova hanno scioperato e hanno manifestato per questo fatto gravissimo. All'interno di Ansaldo Energia, a quanto leggiamo e a quanto pare, si lavora su macchine vecchie di quarant'anni. Vorrei dire che ci stringiamo attorno alla famiglia di questo ragazzo, di quest'uomo, e speriamo che possa vincere la battaglia che in queste ore sta combattendo. andare a lavorare e non sapere se tornerai a casa, morire o rischiare di morire nel 2023 credo che sia qualcosa di assolutamente inaccettabile e insopportabile. In questi primi mesi questo Governo si è occupato molto spesso e prevalentemente di finte emergenze. Noi speriamo sentitamente che nei prossimi mesi voglia occuparsi di un'emergenza vera, quella della sicurezza sul lavoro.

si sono espressi già il nostro Capogruppo alla Camera, condannando ogni forma di violenza e quella violenza, il nostro Capogruppo al Senato e il Capogruppo in Regione Toscana. Devo sommessamente evidenziare che la veemenza con la quale è stato proposto di fronte all'opinione pubblica questo episodio e invece e invece l'eccessivo silenzio che viene riservato ai tanti episodi di violenza che vengono perpetrati dalla sinistra nei confronti dei ragazzi di centrodestra *(Applausi)* non corrisponde a quello che ha detto il collega Parrini, ovvero che condannano tutti gli episodi di violenza. Vi dico che oggi, in questi giorni, la procura della Repubblica di Bologna sta notificando un avviso di 415-*bis* a dodici persone che si sono incontrate

di ragazzi di Azione universitaria, tra i quali c'era anche il Capogruppo di Fratelli d'Italia in Comune a Bologna. Sono indagati e ad oggi imputati per rapina, violenza privata, lesioni e minacce (erano in trenta). Non ho visto una riga a livello nazionale, quando sette mesi fa questi episodi sono accaduti. *(Applausi)*. Non ho sentito una parola su questa violenza dei collettivi di sinistra nei confronti dei ragazzi di destra. Rispetto a quell'episodio tutta Fratelli d'Italia ha espresso solidarietà e condanna ferma nei confronti di ogni forma di violenza, come fa sempre. Dopodiché, proprio come ricordava il collega, diciamo anche che, quando ci sono le indagini della magistratura, le sentenze non si traggono prima, ma si aspetta l'esito dell'indagine e si condanna sempre e soltanto la violenza, quando c'è, però da tutte le parti. Attendiamo l'esito delle indagini. Crediamo che il Presidente del Consiglio abbia anche tanto altro da fare e probabilmente era impegnata in questi giorni; nel momento in cui le massime cariche di Fratelli d'Italia si esprimono e condannano ogni forma di violenza, credo che sia sufficiente. Aspettiamo la condanna degli episodi e delle violenze di sinistra, altrettanto squadriste.